questa legge di bilancio è nata sotto una cattiva stella. Ci sono volute le opposizioni per rendere più digeribile il testo. Il voto alla manovra, però, resta gravemente insufficiente. Ma perché ho detto che è nata sotto una cattiva stella? L'intemerata o, per meglio dire, la velata minaccia che la Presidente del Consiglio ha rivolto nei confronti della propria maggioranza al fine di precludere la possibilità di presentazione degli emendamenti, è qualcosa di inedito nella storia della Repubblica. È qualcosa che si contrappone fortemente al corretto esercizio del mandato parlamentare come garantito dall'articolo 67 della Costituzione. Secondo questa fine strategia politica, si sarebbe dovuto approvare il testo della legge di bilancio senza alcuna difficoltà in via definitiva molto prima di Natale, almeno così si leggeva sui quotidiani. Nulla di più lontano dalla realtà. Figuriamoci cosa sarebbe successo se anche i componenti della maggioranza avessero potuto presentare emendamenti. È vero, senatore Lotito? Brucia più la sconfitta con l'Inter o la mancata approvazione dell'emendamento relativo al rientro dei cervelli, comprensivo anche dei calciatori? E ancora, saremmo stati curiosi di verificare la spaccatura della maggioranza sul voto su di un emendamento sul superbonus. Forza Italia era favorevole, ripensateci, non voltate le spalle a milioni di italiani che hanno ancora progetti *in itinere.* Molti in quota alla maggioranza ne hanno usufruito: date anche agli italiani quantomeno la possibilità di ultimare i lavori in avanzato stato. È stato approvato un emendamento unitario delle opposizioni relativo alla violenza di genere, giustamente la norma più evidenziata dall'informazione. tolto questo, la maggioranza cosa aveva previsto? Cosa c'era nel testo a favore delle donne vittime di violenza? Il buio. A parole tutti bravi, poi quando si tratta di stanziare somme per le donne, la coperta risulta sempre troppo corta. Invece, quando si parla del Ponte sullo Stretto si saccheggia, ahimè, il Fondo per lo sviluppo e la coesione e conseguentemente si sottraggono ingenti somme alle Regioni Calabria e Sicilia, le quali avrebbero sicuramente investito i soldi in maniera differente.

Sui giornali leggo con stupore di continui dissidi nella maggioranza: staremo con i popcorn a osservare le diatribe del centrodestra all'approssimarci delle elezioni europee, ad iniziare dalla scelta di campo relativa a quale delle grandi famiglie europee vorranno appartenere. Siamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento; poteva essere fatto di più; di certo poteva essere fatto meglio; visti i tempi, però, siamo soddisfatti del risultato. Certo è che se la maggioranza non avesse proposto emendamenti iperlocalistici, magari avrebbe potuto convergere sull'emendamento e investire somme superiori rispetto a 40 milioni. Sulla giustizia, invece, non è stato fatto niente. Abbiamo proposto un complesso pacchetto emendativo sul tema, direi forse anche troppo per la maggioranza, perché non è stato compreso. l'assunzione di 250 magistrati subito e non legati alla scellerata riforma proposta dal ministro Nordio, che prevede sì l'assunzione di 250 magistrati, ma la lega al nuovo procedimento cautelare che si trasforma in collegiale. Se questa riforma dovesse vedere la luce, servirebbero non 250 ma 2.500 magistrati in più per far fronte all'incompatibilità che da questa norma deriverebbe. le assunzioni del comparto di polizia penitenziaria, di funzionari al Ministero della giustizia, dei mediatori culturali e funzionari giuridico-pedagogici sono state assolutamente ignorate da questa maggioranza. Sul PNRR siamo in ritardo con il *timing* perché manca il personale. Noi proponiamo assunzioni e voi le ignorate perché preferite modificare la prescrizione, la normativa relativa al *trojan*, alleggerire la normativa di contrasto ai delitti dei cosiddetti colletti bianchi (leggasi abolizione dell'abuso di ufficio), prevedete un'udienza partecipata per l'esame del contenuto dei cellulari, con serio pericolo di *disclosure* e quindi di violazione del segreto istruttorio; declassate i delitti contro la pubblica amministrazione nell'esercizio dell'azione penale; ostacolate le proroghe nelle intercettazioni. Tassello dopo tassello state demolendo il codice di procedura penale? *(Applausi)*. disegno di legge di bilancio non ci ha assolutamente convinti, come del resto nessuna delle politiche finora espresse da questa maggioranza di destra,

la prima è che sarà approvata con un voto di fiducia e la seconda è che rappresenta una dimostrazione ulteriore che a questo Governo interessa poco investire sulla promozione dell'Italia nel mondo e sulle sue comunità all'estero. Questo poco interesse il Governo l'ha dimostrato con il decreto *made in Italy* e lo ribadisce in legge di bilancio. Purtroppo, non ritiene importante investire per permettere all'Italia di costruirsi una posizione di sempre maggior prestigio a livello mondiale. Non è una priorità. Avevamo presentato emendamenti che costituivano un'occasione di investimento, ma il Governo, come ha fatto fino ad oggi, ha preferito andare avanti senza considerare proposte sulle quali imbastire anche un discorso comune per risolvere problematiche che vanno al di là dei partiti e degli schieramenti e che rappresentano le esigenze vere del Paese. Per esempio, non è stato minimamente considerato l'impatto che gli investimenti in lingua e cultura all'estero possono avere sul futuro imprenditoriale ed economico del nostro Paese.

Immaginate il potenziale che per il nostro Paese ha ogni singolo studente che studia l'italiano all'estero; pensate a quanto frutta ogni singolo euro investito per insegnare la lingua e la cultura italiana a livello primario e secondario e a quanto le conoscenze culturali acquisite da questo studente a scuola coinvolgano la famiglia e ne cambino o amplino lo stile di vita e di acquisto. Sembra che questo Governo non riesca a capire che a livello mondiale sono lingua e cultura che contribuiscono a creare quell'immagine del *made in Italy* e dell'*italian style* che si riverbera poi in ciò che si acquisterà o nel luogo in cui si trascorreranno le vacanze. Il Governo non riesce a valutare come lo sviluppo di lingua e cultura contribuisca a diffondere l'italianità, per esempio tramite il risveglio delle origini degli oltre 80 milioni di discendenti italiani che vivono nel mondo, che poi sono quelli che spesso arrivano qui e investono ingenti capitali anche in aree del Paese giudicate meno appetibili. Si continua ad ignorare il contributo che nella promozione culturale e linguistica giocano gli enti gestori e le nostre comunità all'estero. Eppure, nei nostri emendamenti avevamo cercato di porre rimedio a queste mancanze. Avevamo tentato di accendere i riflettori sui punti essenziali che riteniamo una base di partenza per programmare il futuro, evitando che si continuasse con la scure dei tagli,

Abbiamo solo ottenuto in legge di bilancio che si cercasse di porre rimedio alla situazione del personale a contratto dei consolati e delle sedi diplomatiche nel mondo: almeno su questo, anche se solo in parte, ci avete ascoltati; è un piccolo intervento, che certamente aiuta, ma non risolve il problema. La nostra rete diplomatica è quella addetta a offrire servizi ai cittadini, siano essi temporaneamente residenti all'estero, discendenti di italiani, turisti intenti a visitare l'Italia o imprenditori che vogliono investire nel nostro Paese ed è impensabile che non sia messa nelle condizioni di lavorare o che i suoi dipendenti in alcuni Paesi percepiscano salari non adeguati al costo della vita e per la professionalità richiesta. Ormai la mancanza di personale in alcuni consolati ha portato le attese per i servizi di cittadinanza oltre ogni tempo ragionevole e anche questo, signor Presidente, influenza l'opinione sull'Italia e sul *made in Italy* nel mondo. Non possiamo più permetterci quest'incapacità di offrire servizi ai cittadini e a chi è interessato all'Italia: non è degno di un grande Paese come il nostro, che soprattutto ambisce a primeggiare nei mercati mondiali. Nel futuro, come dicevo prima, dobbiamo trovare una soluzione strutturale a questo problema. La legge di bilancio poteva anche essere un'occasione per dare risposte su alcuni temi di giustizia sociale, per l'equiparazione dei diritti dei cittadini italiani residenti in Italia e di quelli residenti all'estero. Casa, sanità, tasse: ci sono oggi sperequazioni che potevano essere colmate attraverso la ricezione di alcuni dei nostri emendamenti e che invece si è deciso di non considerare, perdendo un'altra occasione importante. Una per tutte: l'impossibilità per gli italiani iscritti all'AIRE di usufruire del sistema sanitario nazionale quando tornano temporaneamente in Italia, cosa che invece è concessa ai cittadini stranieri provenienti da Stati europei ed extraeuropei (ma non ai cittadini italiani). Avevamo anche segnalato questioni relative a enti istituzionali, come i Comites e il CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), per far sì che avessero l'opportunità di adempiere ai propri ruoli, contando su un bilancio che, per quanto ristretto, potesse comunque contribuire alla promozione della lingua e della cultura italiana e alle iniziative di sostegno alle comunità locali. In altre parole, permettere a questi due organi istituzionali eletti organi istituzionali eletti dalle comunità italiane all'estero di essere parte integrante ed effettiva del sistema Italia; ma anche in questo caso abbiamo riscontrato la chiusura totale della maggioranza. In sintesi, signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato a questa legge di bilancio avevano lo scopo quantomeno di ripristinare i tagli di oltre due milioni di euro che il Governo ha apportato a tutte le voci connesse con gli italiani e l'Italia all'estero; tagli che continuano a dimostrare una scarsa visione strategica per l'Italia. Il futuro del nostro Paese non può non includere uno sviluppo dell'Italia connesso a questa grande opportunità rappresentata dalle sue comunità nel mondo, rappresentano (rappresentiamo) di per sé un mercato di 80 milioni di persone, che comprano italiano senza bisogno di essere convinte o raggiunte da chissà quale strategia di *marketing*; 80 milioni di persone di discendenza italiana nel mondo, che costituiscono gli avamposti del *made in Italy*, i suoi ambasciatori più proficui, che influenzano, con la loro italianità, le comunità non italiane con cui vivono a contatto stretto e che ricoprono cariche importanti nei centri decisionali dei Paesi in cui vivono. Non si può, signor Presidente, continuare a ragionare pensando che l'Italia sia solo ciò che è racchiuso all'interno dei confini dello stivale. L'Italia è ormai nel mondo, con la sua gente, le sue imprese, la sua cultura il suo *know how*, e una visione strategica è ciò che una legge di bilancio dovrebbe avere per definizione intrinseca. Non può essere miope di fronte a questa realtà e non pensare di strutturare quanto già esiste per amplificarne i risultati già spontaneamente ottenuti. Questa legge di bilancio, il disegno di legge *made in Italy*, il decreto per la riduzione dei benefici fiscali per i rimpatriati secondo noi sono provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata, ovvero quella della chiusura dell'Italia verso le comunità italiane nel mondo e della totale mancanza di considerazione nei loro confronti. In conclusione, signor Presidente, potrei dire che il Governo e le forze di maggioranza hanno perso un'altra buona occasione. Purtroppo questa occasione non l'hanno persa solo le forze di maggioranza e il Governo, ma l'abbiamo persa noi tutti, l'ha persa l'Italia.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi in Aula credo sia necessario, dopo

e dalle mistificazioni, che consenta agli italiani, sempre nel pieno rispetto degli equilibri democratici, di giudicare il lavoro che è stato svolto dal Governo Meloni sulla legge di bilancio e sui provvedimenti che ad essa sono collegati.

io ne faccio parte e posso confermare la qualità del lavoro che è stato svolto, in un clima assolutamente concreto e pratico

surreali. Se da una parte è chiaro a tutti che quando si fa politica bisogna confrontarsi anche con quello che è il consenso popolare ed elettorale, non bisogna però distorcere e ribaltare completamente la realtà, ma bisognerebbe fermarsi al confine dell'etica e della morale, o almeno - dico io - della decenza. decenza. Ringrazio il presidente Calandrini per aver gestito in modo ordinato - l'hanno detto ieri anche i colleghi - i lavori in Commissione, che ci hanno visti impegnati in una maratona non certo dovuta al caos, come ha sostenuto qualcuno dai banchi dell'opposizione, ma più che altro all'attenzione che è stata riposta su ogni proposta emendativa e ogni sollecitazione che è venuta da parte dei vari portatori di interessi. Anche quest'anno si arriva ad approvare una legge di bilancio nei tempi giusti, con buona pace di tutti i gufi e di chi tifa contro l'Italia. Arriviamo ad una manovra che è prudente, responsabile e realistica, ma non per questo una manovra rinunciataria. I ringraziamenti vanno ai nostri relatori, al nostro capogruppo Liris, ma anche ai colleghi Testor e Damiani. È proprio dai loro interventi e dalla loro relazione che voglio prendere spunto, perché non possiamo non porre l'attenzione sui numeri complessivi: parliamo di 24 miliardi di euro, di cui come noto - 16 miliardi di extra-*deficit* e 8 miliardi che derivano da una riduzione di spese che è stata attuata dai vari Ministeri, che è pari a circa il 5 per cento di tutte le voci discrezionali. Qualcuno ha detto che è mancato il coraggio e che siamo tornati all'*austerity*: a questo qualcuno voglio rispondere che andrebbe ricordato che nel 2024 l'Italia avrà circa 13 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito da pagare in forza

100 miliardi di buco creati dalla più grande truffa della storia italiana. *(Applausi)*. Allora, più che il coraggio, semmai, sono mancate le risorse, che sono state gettate dalla finestra dai signori del gratis; quindi più che l'*austerity*, diciamo che è tornata la serietà. Qualcuno ha aggiunto, nel commentare questa manovra, che mancano gli interventi sul caro vita e sul caro carburante. Allora mi chiedo - e vi chiedo - se i 10 miliardi sulla conferma del taglio del cuneo fiscale e gli otto miliardi per il rinnovo dei contratti del 2022-2024 del pubblico impiego, della sanità e delle Forze dell'ordine in testa non siano un intervento a difesa del potere di acquisto e contro il caro vita. Allora, i 18 miliardi su 24, che sono impiegati per tutto questo, non sono forse un aiuto agli italiani? Dobbiamo dedurre che per le opposizioni un intervento che mette in busta paga ben 100 euro al mese a circa 18 milioni di lavoratori sia un fatto trascurabile. Per noi non lo è. Dobbiamo desumere che per le opposizioni, quelli che si stracciano le vesti per il salario minimo a nove euro l'ora, non sia importante evitare che un agente di polizia guadagni sei euro l'ora durante gli straordinari. E così ancora ricordiamo il tetto del *fringe benefit* che è stato portato a 2.000 euro per i lavoratori con figli e a 1.000 euro per tutti gli altri. Anche questi questi provvedimenti, a nostro giudizio, non sono fatti assolutamente trascurabili. Capisco che sia poco interessante per chi è passato dalle 5 Stelle nel simbolo alle 5 stelle di Cortina, ma io vi assicuro che per molti italiani 100 euro in più in busta paga non saranno affatto una questione trascurabile. Parliamo degli stessi che non comprendevano gli interventi del Governo Meloni sul caro carburante e che ora, visto invece il repentino calo dei prezzi, hanno perso la loro loquacità. Qualcuno ha detto che c'è poco o nulla per le famiglie, per le imprese e che c'è zero crescita. Andiamo per punti: abbiamo introdotto il principio del più assumi e meno paghi, una super deduzione del costo del lavoro per i nuovi contratti a tempo determinato, un 120 per cento che arriva fino a 130 per per chi assume mamme, *under* 30 percettori del reddito di cittadinanza e persone con invalidità. C'è la nuova Sabatini, ulteriormente finanziata con 30 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni di euro annui per gli anni che vanno dal 2024 al 2026. Si tratta di una misura cruciale per le micro, piccole e medie imprese, che facilita l'acquisto o il *leasing* di beni strumentali materiali e immateriali, come i macchinari, le attrezzature e i *software*. C'è poi la recente revisione del PNRR, un grande successo per il Governo Meloni, grazie a cui avremo di fatto una seconda manovra finanziaria incentrata sulla crescita e sulla competitività del sistema produttivo; ben 12,4 miliardi in più per le imprese, risorse aggiuntive rispetto ai 19,6 miliardi in dotazione e ai 7,7 miliardi del fondo complementare. un totale di 37 miliardi di euro. Cito una misura su tutte: la Transizione 5.0 con 6,3 miliardi di euro per per sostenere la transizione verde e digitale delle imprese, compresa l'autoproduzione di energia rinnovabile. poi l'esonero totale dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri con due o più figli, il potenziamento del *bonus* asilo, con un incremento progressivo dell'autorizzazione di spesa annuale, partendo da 240 milioni nel 2024 fino a raggiungere 306 milioni annui a partire dal 2029. Qualcuno ha osato dire che i tagli del Governo colpiscono la sanità. Basterebbe ricordare che i 37,5 miliardi di euro che sono stati tagliati dal 2010 al 2019 oppure la favola del 7,4 del PIL investito in sanità nel 2020 sono solo uno dei miracoli del presidente Conte, dovuto al crollo del PIL italiano durante la pandemia. Noi invece dovremmo richiamare e ricordare i 136 miliardi previsti *(Applausi)*, il più alto stanziamento di sempre, e i fondi che sono stati indirizzati in modo specifico per il contrasto alle liste di attesa.

Sono tanti gli interventi che sono stati fatti dal Governo. In tutto questo vogliamo dire che la nostra manovra merita la dovuta attenzione e nei confronti di chi critica una manovra seria, coerente e responsabile, di chi agita la bacchetta magica millantando di avere tutte le soluzioni per quella stessa Italia che in realtà ha messo in ginocchio, noi non invochiamo il giurì d'onore, non è il caso: a darvi la sentenza di sfratto ci hanno già pensato gli italiani e per noi questa è l'unica cosa che conta.

della NADEF, che riportava un'incidenza negativa sulle capacità di spesa dovute al ribasso delle previsioni di crescita del PIL, ma soprattutto ai 20 miliardi di debito creati dal superbonus che ci porteremo dietro per anni e al debito creato dal reddito di cittadinanza. Nonostante questi problemi, il Governo ha creato una legge di bilancio con diverse risposte per gli italiani, le imprese e le famiglie, in particolare: il taglio del cuneo fiscale per circa 10 miliardi per il rinnovo dello stesso nel 2024, ossia il 7 per cento per i redditi fino a 25.000 euro, 6 per cento per i redditi fino a 35.000 euro;

altre misure a sostegno delle famiglie e della natalità per 1 miliardo di euro, tra cui anche il rifinanziamento del Fondo prima casa, soprattutto per i giovani. Sulla sanità mi voglio soffermare più approfonditamente, perché tanto si è detto in quest'Aula, sui giornali, in televisione, a discapito degli investimenti che questo Governo fa. Parlo di investimenti perché la sanità non è un costo, ma un investimento che lo Stato fa sulla salute dei cittadini e un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Ebbene, siamo passati dai 115 miliardi stanziati prima del Covid nel 2019 ai 134,1 miliardi in questa manovra nel 2024, fino ad arrivare a 136 miliardi miliardi nel 2026: nessun Governo aveva mai investito così tanto fino ad ora nel sistema sanitario nazionale. In un periodo come quello attuale, caratterizzato da scarsità di risorse cui attingere, da crisi internazionali, da situazioni economiche e sociali flagellate dall'aumento dei prezzi sull'onda dell'inflazione e dell'aumento dei costi energetici, il Governo ha ritenuto di tutelare appunto il diritto alla salute sancito dalla Costituzione, incrementando gli stanziamenti di oltre 3 miliardi per il 2024, fino ad arrivare a 4,2 miliardi fino al 2026. fronte di questi numeri, non mi sembra che questo Governo abbia fatto tagli alla sanità pubblica. Vorrei anche spiegare meglio l'uso distorto e strumentale dell'incidenza percentuale sul PIL della spesa sanitaria, perché questo è un indicatore ambiguo sostanziandosi in un rapporto che dipende anche dall'andamento del PIL. Inutili quindi le proposte delle Regioni, come per esempio

Dobbiamo quindi guardare i veri numeri in dettaglio, stabiliti dalla legge di bilancio. Scendendo nel dettaglio delle misure, voglio sottolinearne alcune poiché particolarmente significative: l'incremento *record* di circa 2,4 miliardi delle risorse a valere sul Fondo sanitario nazionale per il rinnovo dei contratti del personale sanitario, al fine di affrontare la carenza del personale medico e del comparto, di ridurre le liste d'attesa e l'utilizzo delle esternalizzazione; l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e infermieristico; ulteriori misure per il rifinanziamento dei piani operativi per l'abbattimento delle liste d'attesa, estendendo anche per l'anno 2024 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare le strutture private accreditate; l'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, e ciò permetterà ai sistemi sanitari regionali e delle Province autonome di poter garantire a tutta la popolazione nazionale i nuovi livelli LEA, anche ricorrendo al privato accreditato. In tema di spesa farmaceutica, una prima proposta normativa prevede la rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dal 2024 e, conseguentemente, la spesa farmaceutica convenzionata rideterminata nel valore del 6,8 Una seconda proposta, davvero rivoluzionaria, mira a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate del Servizio sanitario nazionale e ai malati cronici di avere direttamente a disposizione i farmaci nelle farmacie territoriali. Questa soprattutto è una misura importante per gli anziani, per avere a disposizione i farmaci sul

a fronte anche di una proposta della Lega, che è in realtà una proposta di maggioranza, perché poi è stata sottoscritta da tutti i partiti. Si tratta del disegno di legge n. 224. In questa legge di bilancio si è deciso di investire 250 milioni per il 2025, 350 milioni per il 2026 per il personale dipendente e dieci milioni di euro per il per il Fondo per le cure palliative e terapie del dolore. Questa è una misura molto importante. *(Applausi)*. Infine, abbiamo anche ascoltato le opposizioni. Io faccio parte dell'Intergruppo per l'Alzheimer e le demenze. L'opposizione ha presentato un emendamento, che è diventato l'articolo 50-*bis*, votato all'unanimità. Questo mostra la capacità di ascolto del Governo di questa maggioranza anche delle proposte che nascono dall'Intergruppo. Un Fondo per l'Alzheimer e per le demenze, dunque, stabilito per 4,9 milioni per il 2024 e per 15 milioni per il 2025 e per il 2026. 2026. Signor Presidente, nei collegati fiscali collegati alla manovra, oltre alla riorganizzazione e al potenziamento del sistema territoriale, vi è anche la delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati del Ministero della salute. Sono due punti importanti che, oltre a tutti gli altri collegati a questa manovra di bilancio, dovremo

per il lavoro importante che è stato svolto per raggiungere questo obiettivo. Tanto lavoro ci aspetta nei prossimi anni, proprio per portare avanti quanto abbiamo promesso in questa legge di bilancio e soprattutto per riorganizzare e rinnovare il nostro sistema sanitario nazionale.

ora più che altre volte in cui ho avuto il privilegio di intervenire in quest'Aula, provo un senso di profonda amarezza. Nel gioco delle parti, che è proprio quello della politica, nell'alternanza di Governo che è propria della nostra democrazia, è normale e legittimo che una volta si sia all'opposizione e una volta invece si sia chiamati ad avere responsabilità di Governo. Siccome qui stiamo discutendo della legge più importante che il Parlamento è chiamato ad approvare, nessuno si nasconde dietro ipocrisie: la maggioranza fa la maggioranza e l'opposizione altrettanto. Vi sono, però, questioni, tuttavia, sulle quali non può esistere una spaccatura e rispetto alle quali invece sarebbe doverosa una certa trasversalità e una visione comune, rispetto alla cultura della legalità, alla lotta alle mafie e alla corruzione. sono quei casi in cui le nostre azioni, i nostri provvedimenti, ciò che noi facciamo in queste Aule, rappresentano una difesa del nostro Stato di diritto, della qualità della nostra democrazia, delle istituzioni che rappresentiamo, del profondo senso di giustizia su cui esse si fondano. Per far comprendere l'amarezza che provo nell'intervenire oggi in Aula, vorrei raccontare qualche storia, che forse molti di voi conoscono. La prima è la storia di un testimone di giustizia, la storia di chi, di fronte alla mafia, ha deciso di fare la cosa più difficile, difendere la verità e scrivere una pagina di giustizia, anche a costo di sacrificare la propria vita. Sì, perché quando Piero Nava, il 21 settembre del 1990, vide con i propri occhi l'esecuzione del giudice Rosario Livatino, avvenuta per mano della mafia, con una vera e propria esecuzione sulla superstrada tra Canicattì ed Agrigento, non esitò un istante a raccontare ciò che aveva visto alla polizia. Le sue parole furono fondamentali, perché permisero di individuare gli esecutori del delitto del giudice Livatino. Con quella testimonianza Nava divenne il primo testimone di giustizia, una figura che non va confusa con il collaboratore di giustizia, che è notoriamente colui che da affiliato, da complice della mafia, decide di collaborare con lo Stato. La scelta del testimone di giustizia Nava ha cambiato radicalmente la sua stessa vita: dopo quella scelta di coraggio, pagherà il suo gesto perdendo il lavoro e i propri affetti, finendo nel più assoluto isolamento, costretto a cambiare più volte residenza ed emigrare all'estero. Ma nonostante tutto, Nava non ha smesso un giorno di credere allo Stato, non si è mai pentito della scelta, al contrario si è fatto carico di un compito ancora più gravoso, ovvero raccontare la sua storia e il suo gesto ai ragazzi, agli studenti, nelle università, nelle scuole, nei luoghi della cultura. Ebbene, per Piero Nava lo Stato ha previsto un'indennità che non potrà mai e poi mai ripagare l'enorme sacrificio che ha rappresentato il suo gesto ed è la ragione per cui avevamo presentato un emendamento che permettesse a Nava di rendere reversibile, secondo le regole dei trattamenti pensionistici, l'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese. Questo Governo risponde con un impegno vago, un ordine del giorno, un'azione minuscola se paragonata all'enorme coraggio di Piero Nava e dei tanti altri testimoni che ne potrebbero usufruire. Credo che non serva aggiungere ulteriori commenti. L'altra storia è quella di tante donne che si rifiutano di ritenere quella mafiosa l'unica organizzazione sociale possibile, donne che hanno deciso di infrangere codici millenari fondati sulla violenza, sulla minaccia e sul rispetto timoroso di un ruolo subordinato. Chiedono una mano per fuggire dalle mafie con i loro figli. Per loro fuggire dalle mafie significa essere in pericolo di vita, perché la famiglia mafiosa, per ripristinare il potere, le deve uccidere. Non mi dilungo sulle tante donne uccise solo perché avevano denunciato i loro mariti, padri, fratelli; Lea Garofalo è quella che forse più di tutti conosciamo; la sua ribellione alla 'ndrangheta l'ha pagata con la vita. Queste donne, grazie al progetto «Liberi di scegliere», tra l'altro sottoscritto da alcuni Ministeri, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, dalla procura per i minorenni, dalla Procura nazionale antimafia, dall'Associazione Libera e dalla Conferenza episcopale italiana, è uno strumento per uscire dal circuito mafioso. Avevamo presentato un emendamento perché anche a loro lo Stato riconoscesse la possibilità di un reddito di libertà. Parliamo di donne molto spesso vittime della violenza mafiosa, costrette a subire quella concezione di possesso tipico della società patriarcale su cui la mafia trova radici. Voglio riportarvi la testimonianza di una di loro, forse conoscendo e ascoltando le parole dirette delle persone che le vivono, sentiamo una maggiore responsabilità. non si aspettavano che saremmo andati via. Ci sono riuscita fingendo anche di essere pazza perché era un modo di non farmi più tenere in considerazione. Era il 2008 e per due anni avevo provato a partire chiedendo aiuto. Purtroppo nessuno ci è stato di aiuto. Nel 2010 però ho conosciuto don Luigi Ciotti, ho conosciuto Libera che ci ha supportato in tutto, nella nostra partenza e nella nostra riabilitazione, aiutandoci a rieducarci nella civiltà. Oggi viviamo, anzi sopravviviamo, ci nascondiamo, non abbiamo la nostra identità e questo ci impedisce di farci sentire persone, ci nega il riconoscimento. Quello che chiedo, quindi, è il diritto alla vita, per me e i miei figli. Vogliamo vivere. Anche su questo, signor Presidente, avevamo presentato un emendamento perché si desse loro la possibilità di uscire da questa condizione, di affermare la forza dello Stato su quella della mafia. Questo emendamento non ha meritato alcuna attenzione, nonostante un impegno sul tema dovuto in larga parte all'azione dell'opposizione. Era anche un segnale importante per tante altre donne che vivono in contesti mafiosi e hanno paura. Noi abbiamo il dovere istituzionale di dare loro voce e strumenti per liberare la loro libertà, il loro coraggio. *(Applausi)*. La loro forza dipende da quello che noi sappiamo fare. Per loro non avete fatto nulla. Potrei andare avanti e citare in questa manovra l'assenza dei fondi per i beni confiscati, gli stessi distratti dal ministro Fitto e che sarebbero dovuti arrivare da provvedimenti di cui ancora non c'è traccia, oppure l'assenza di volontà di rifinanziare il fondo per i progetti sulla legalità nelle università. Anche questo emendamento non ha incontrato alcun pensiero. Potrei andare oltre, ma non ho tempo a disposizione. Mi auguro che un giorno su legalità e difesa dello Stato questo Governo faccia qualcosa di concreto, che la politica possa lavorare unita. Prendo atto, però, con amarezza che non è questo il giorno. La *premier* Meloni in ogni suo intervento sul tema delle mafie parla spesso del giudice Paolo Borsellino: la strage di via D'Amelio è stata lo stimolo - dice - per il suo impegno. Forse però la Presidente del Consiglio e tutto il Governo dimenticano il significato profondo delle parole di Paolo Borsellino quando diceva che per togliere il consenso alle mafie dobbiamo lavorare sì sulla repressione (e questo lo fanno le Forze dell'ordine, la migliore magistratura che abbiamo in questo Paese e, ancora, la migliore legislazione antimafia), è più importante seminare la cultura della legalità e della responsabilità. Servono tanti maestri. *(Applausi)*.Con queste scelte il Governo non va in questa direzione; fa solo proclami e interventi *spot*.

Presidente, onorevoli colleghi, lo dico senza giri di parole: parole: piuttosto che un disegno di legge di bilancio, questa è un'orazione alla disperazione e al sacrificio di 60 milioni di italiani. È un monumento all'indifferenza che certifica l'egemonia dell'egoismo. Questa è la manovra del siamo pronti, siamo pronti a mettervi il bavaglio, non solo alle opposizioni, ma alla stessa maggioranza. È una manovra orizzontale, anzi prona ai poteri forti. Di certo, se una *premier* verticale, così come è stata definita da esponenti della maggioranza, partorisce una manovra così orizzontale, non c'è da stare allegri per il futuro del Paese. In un contesto storico caratterizzato dall'aumento dei costi delle materie prime, da un'inflazione galoppante, da un Covid che ha rialzato la testa e dalle conseguenze di guerre, questa manovra finanziaria lacrime e sangue, miope e mediocre è un atto di disprezzo verso milioni di cittadini, un attacco diretto contro i più basilari diritti costituzionalmente garantiti, dalla sanità, all'istruzione, alla giustizia (grande assente di questa manovra), ma soprattutto al lavoro, al diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti. Eppure non ora, ma già nei mesi scorsi avevate il dovere di adottare misure concrete per favorire la lotta all'evasione, invece avete aumentato la soglia del contante. Dovevate occuparvi della questione meridionale ed invece con la vostra autonomia differenziata aumenteranno le asimmetrie tra Nord, Sud, Centro e periferie. Dovevate adottare misure di contrasto alla povertà, invece da subito avete attaccato i poveri, modificando il reddito di cittadinanza favorendo il lavoro sottopagato, trasformando una misura universale in una misura categoriale. A proposito di questa misura, ricordo a tutti gli italiani che dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza sarà abrogato e verrà sostituito da una nuova misura che di inclusione porta solo il nome, perché di fatto depennerà dalla Costituzione parole come solidarietà, dignità, coesione, discriminando milioni di italiani che non riusciranno nemmeno più a mettere un piatto a tavola. vorrei dire a tutti i colleghi della maggioranza che sono orgoglioso di aver presentato in questa

innalzato i salari, perché gli imprenditori non avevano più la possibilità di utilizzare degli schiavi disposti a lavorare per una paga da fame. Eppure questo reddito di cittadinanza, il nostro reddito di cittadinanza, aveva avuto l'appoggio anche della Banca d'Italia, che aveva scritto che l'introduzione del reddito di cittadinanza è stata una tappa significativa dell'ammodernamento del *welfare* del nostro Paese e ha contribuito a evitare un milione di poveri in più. La CEI addirittura si era espressa sul reddito di cittadinanza favorevolmente e invece, onorevoli colleghi, in un momento in cui la solidarietà e la coesione sociale sono più importanti che mai, questa maggioranza sta compiendo un atto di segregazione segregazione sociale, creando ulteriori divisioni tra coloro che hanno e coloro che non hanno. Questa non è soltanto una questione economica, ma di giustizia sociale e di equità. La vostra idea di far cassa sui poveri in un momento così delicato è moralmente ripugnante e politicamente irresponsabile: ebbene, era dovere nostro, del Movimento 5 Stelle, opporci con forza a questa manovra di bilancio e lavorare per un'alternativa equa, sostenibile e orientata al benessere di tutti i cittadini, con l'obiettivo di investire maggiori fondi a sostegno dell'istruzione, della sanità, della cultura, dei trasporti, delle infrastrutture (di tutte, non di un'unica) e dell'ambiente, così da garantire che ogni individuo abbia accesso ai servizi di qualità, indipendentemente dal proprio stato sociale ed economico. Onorevoli colleghi, c'è però una cosa che non possiamo accettare, cioè il vostro accanimento contro i più fragili, e non parlo solo della vostra lotta personale contro i poveri, ma anche contro gli italiani con gravi problemi di salute. Lo dimostra il fatto che, subito dopo aver bocciato il mio emendamento sul ripristino del reddito cittadinanza, avete anche respinto e bocciato l'incremento di due milioni del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare.

malattie rare. E ancora, avete bocciato un emendamento per rendere i farmaci di fascia C - sempre per le malattie rare - indispensabili, in alcuni casi, come viene prescritto dai protocolli diagnostici, terapeutici e assistenziali, ma non solo. Non avete neanche

Che prudenza c'è nel dichiarare guerra ai lavoratori fragili, che sono in trincea per sostenere i nostri servizi essenziali pensando bene di bocciare in tronco un mio emendamento che prevedeva la proroga dello *smart working* per i dipendenti pubblici fragili fino al 30 gennaio 2024? Lo chiedo a lei, signor Presidente, e, per il suo tramite, alla maggioranza: è prudente questo atteggiamento nei confronti dei lavoratori fragili della pubblica amministrazione? Lo è? Il Governo Meloni, retto per tutta evidenza da una maggioranza di no vax e negazionisti del Covid, ha così remato contro milioni di italiani che lavorano quotidianamente mettendo a rischio la propria incolumità. Lo dimostra anche il fatto che avete respinto un altro emendamento,

all'interno delle aziende ospedaliere collocate in zone disagiate, quali i territori montani, le aree interne e le isole minori, date le loro particolari condizioni di lavoro. Ricordo, ad esempio, che solo quattro isole possono contare su presidi ospedalieri, mentre nelle altre ci si affida all'operato dei medici di base. Onorevoli colleghi, questa maggioranza sta riuscendo nell'impresa di scatenare scioperi e proteste di piazza. Ieri sono stato con i lavoratori della UIL che hanno gettato una luce sulla decisione vergognosa di aumentare l'IVA sui prodotti alimentari per l'infanzia. Da una *Premier* che - a chiacchiere, evidentemente - si professava attenta all'esigenza di incrementare il tasso di natalità del nostro Paese ci aspettavamo una diminuzione dell'IVA sui prodotti di prima necessità, non certo una sua riduzione sugli alcolici, sui tartufi o sui prodotti estetici.

Il MoVimento 5 Stelle, di fronte allo scempio vergognoso di questa manovra di bilancio, non arretrerà di un millimetro, continuando a presidiare ogni centimetro di democrazia, perché è quando si crede di non avere più motivi per combattere che occorre trovare nuovi motivi per continuare la lotta. E continueremo la nostra lotta. il confronto che abbiamo avuto in Senato sul disegno di legge di bilancio non ha cambiato il nostro giudizio, il giudizio del Partito Democratico sulla manovra; semmai lo ha peggiorato. di legge di bilancio e i provvedimenti connessi definiscono una manovra molto fragile, perché basata su previsioni di crescita largamente sovrastimate e perché finanziata per due terzi a *deficit*. È una manovra di corto respiro quella che ci apprestiamo a votare: quasi tutte le misure più significative sono finanziate solo per il 2024. Vale solo per il 2024 la proroga del taglio del cuneo contributivo; vale solo per il 2024 - ed è un fatto assolutamente inedito - quella che voi chiamate avvio di riforma IRPEF, ma che è un intervento complessivamente modesto e transitorio; vale solo per il 2024 persino l'intervento sul canone Rai, piuttosto che quello sul *welfare* aziendale. Non c'è un euro dal 2025 in avanti. In compenso, c'è una pesantissima ipoteca sul futuro, con oltre 15 miliardi di euro che dovranno essere trovati, dal 2025 in avanti, per confermare queste misure. È una manovra iniqua; vale per tutto quello che è stato fatto sulla sanità. È surreale questa discussione se giudicare l'intervento sulla sanità sul valore assoluto delle risorse stanziate. In tutto il mondo le organizzazioni internazionali valutano il rapporto spesa sanitaria-PIL per dare un giudizio se sia adeguato o meno il finanziamento a un sistema sanitario pubblico. E il rapporto spesa sanitaria-PIL, nel triennio di programmazione, scende a un livello inferiore a quello del 2019, che era ritenuto sottofinanziato da molti osservatori. Non avete imparato le lezioni della pandemia e la sanità pubblica è sottofinanziata da una legge di bilancio che apposta poco più delle risorse che servono per il rinnovo del contratto, ma non quello che serve per le liste d'attesa, per assumere i medici e gli infermieri che mancano, per garantire il servizio universalistico scritto nella Costituzione. Non c'è un euro sulla casa e non c'è un euro sul trasporto pubblico. Ci sono in compenso tagli alle pensioni, perché sarà più difficile andare in pensione con Opzione donna, con APE sociale, per chi è interamente nel sistema contributivo, e rimarrà in qualche misura un taglio probabilmente incostituzionale alle pensioni di oltre 700.000 dipendenti pubblici. *Dulcis in fundo* - si fa per dire l'intervento sull'IVA. Il ministro Giorgetti ci ha raccontato che era necessario riportare dal 5 al 10 per cento l'IVA sui prodotti per l'igiene femminile e per l'infanzia (a proposito di Governo amico della famiglia); ma poi, in sede emendativa, avete abbassato l'IVA sugli integratori alimentari e avete esentato la chirurgia estetica. Evidentemente per voi è più importante la chirurgia estetica dei prodotti per le famiglie e dei prodotti per l'igiene femminile. Questa legge di bilancio si basa su un piano di privatizzazioni da 21 miliardi di euro, che è niente per ridurre il debito, lo 0,7 per cento di un debito che si avvia verso i 2.900 miliardi di euro, ma in compenso rischia di indebolire fortemente il ruolo dello Stato nelle politiche industriali, proprio quando ci sarebbe invece bisogno di una presenza forte dello Stato. Guardate, quello che è accaduto ieri sull'Ilva è imbarazzante e sconcertante: quattro Ministri all'incontro con le organizzazioni sindacali per decidere di non decidere, per l'ennesima volta, sul futuro di una realtà essenziale *(Applausi)* per la siderurgia ed essenziale per la vita di migliaia di famiglie che dipendono da quei posti di lavoro. Questa è una manovra di stagnazione, una manovra di austerità ed è una manovra che non rilancerà la crescita di questo Paese. Basta leggere i dati di cinque giorni fa di Banca d'Italia, che ha previsto per il 2024 una crescita dello 0,6 per cento, esattamente la metà di quello che avete programmato nel disegno di legge di bilancio. Ed è una crescita, quella stimata dalla Banca d'Italia, che incorpora quanto voi avete previsto nella manovra di bilancio. È una manovra di stagnazione ed è l'antipasto dell'austerità verso cui voi vi state incamminando, perché il il Governo ha perso la partita sul nuovo Patto di stabilità e crescita. Questo è il risultato vero del negoziato che si è concluso all'Ecofin di ieri in videoconferenza, che secondo il ministro Giorgetti non doveva portare ad una decisione finale. finale. Voi, nei mesi scorsi, avete attaccato a testa bassa il commissario Gentiloni, che aveva lavorato ad una proposta che era un punto di avanzamento vero rispetto al vecchio Patto di stabilità. Lo avete attaccato e accusato di essere contro il nostro Paese, ma ieri la presidente Meloni e il ministro Giorgetti hanno avallato e accettato a testa bassa un accordo che è molto peggio della proposta della Commissione. *(Applausi)*. Questo perché nell'accordo di ieri entrano regole automatiche, pro-cicliche e vincolanti di riduzione annuale del *deficit* e del debito che non c'erano nella proposta della Commissione. Per mesi avete chiesto una *golden rule*, una regola aurea sugli investimenti per l'economia verde, per il digitale e per la difesa. Non c'è traccia della *golden rule* nell'accordo che ieri avete avallato. ieri avete avallato un accordo che, di fatto, è esattamente lo stesso accordo che si profilava nei giorni scorsi, quando - voglio rinfrescare la memoria a chi l'ha corta - la presidente Meloni evocava il veto molti di voi chiedevano il rinvio a gennaio. Non c'è stato alcun rinvio, Francia e Germania hanno deciso anche per noi e voi vi siete accodati. Vi siete accodati sulla cosa più importante, il Patto di stabilità e crescita, mentre oggi vi dividete, in modo incredibile e indecoroso, su una cosa che conta meno, che è significativa, ma non ha la portata del Patto di stabilità, perché quanto sta accadendo alla Camera con Fratelli d'Italia e Lega che stanno dando parere contrario alla ratifica del trattato istitutivo del MES, mentre Forza Italia si asterrà, dà il segno dello stato confusionale in cui versa questa maggioranza che fa la voce grossa sulle cose sbagliate, mentre accetta supinamente accordi penalizzanti per il nostro Paese. *(Applausi)*. Allora, signor Presidente, è evidente la responsabilità del Governo verso queste decisioni che stanno venendo avanti. Dovevate fare fronte comune con Francia e Spagna, non l'avete fatto per ragioni politiche, perché in Francia state con Le Pen e in Spagna state con Abascal, e vi siete ritrovati da soli in Europa sul Patto di stabilità e sul MES state dando lo spettacolo che è sotto gli occhi di tutti. Questo è il quadro: è un quadro molto negativo per l'Italia, sia sulla manovra di bilancio che per le decisioni che stanno venendo avanti in Europa. *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, rappresentanti del Governo,

sicuramente il mio intervento al cuore della manovra e metterlo in evidenza. Innanzitutto, voglio ringraziare il Governo per una manovra coraggiosa in un momento difficile della nostra storia italiana: il quadro internazionale, due guerre, l'aumento del prezzo dei combustibili fossili e le sue variabili vedono ancora gli strascichi della crisi energetica sulla nostra economia. L'aumento dell'inflazione ha costretto la Banca centrale europea a intervenire con decisioni di politica monetaria dure per un Paese con uno *stock* di debito pubblico elevato come quello italiano. I maggiori interessi passivi ammontano a 12,5 miliardi su un totale di quasi 97 miliardi rispetto ad una manovra che ha un valore netto di poco più di 21 miliardi. Le decisioni della BCE sui tassi e sul piano degli acquisti di titoli dei Paesi dell'Europa condizionano i rendimenti dei titoli di Stato, chiaramente italiani. Al contrario, lo *spread* a 167 punti di base, sceso di oltre il 20 per cento dall'inizio del 2023, e i giudizi dell'agenzia di *rating* fotografano una Italia in grado di meritare un *outlook* positivo, cioè la prospettiva di un'economia in crescita. Oltre alle agenzie di *rating*, i dati della bilancia dei pagamenti, che sono di ieri, ci dicono contrariamente, caro Misiani, a quanto da lei detto, che aumenta la fiducia degli investitori internazionali nel nostro Paese. Il Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ha stimato la crescita per il 2024 all'1,2 per cento, cioè circa 24 miliardi di euro. Noi riteniamo che sia un obiettivo raggiungibile e realistico, attivato peraltro da una leva finanziaria in *deficit* di soli 15,7 miliardi di euro. Lo straordinario lavoro fatto dal Governo sul PNRR ha dimostrato anche ai pessimisti che l'Italia sta facendo molto bene. Entro la fine di quest'anno saranno arrivati 102 miliardi di euro in Italia dall'Europa, altri 92,4 miliardi arriveranno tra il 2024 e il 2026. L'impatto degli investimenti del Piano nazionale, cui si unirà quello dei fondi di coesione, sulla crescita del prodotto sarà importante. Le riforme chieste dalla Commissione europea procedono celermente grazie al lavoro proficuo del Parlamento e sono parte integrante delle decisioni di bilancio. In questo quadro di difficoltà, che vede anche un'eredità pesante dei crediti d'imposta edilizi (18 miliardi nel 2023 e 22 miliardi nel 2024), la manovra è molto razionale

La spesa non poteva continuare a crescere senza una precisa ridefinizione delle poste e una revisione di quella improduttiva. La diminuzione di oltre un punto percentuale del rapporto debito-PIL è un ulteriore indicatore di un'azione efficace dell'azione di bilancio. La decisione europea di ieri sul nuovo Patto di stabilità rafforza, caro senatore Misiani, la concretezza e la lungimiranza dell'azione di Governo che si è dato *target* di bilancio sostenibili e raggiungibili. La manovra è realistica perché le norme in esame operano un attento e scrupoloso intervento di riprogrammazione, rifinanziamento e soprattutto definanziamento sulle due sezioni che compongono il disegno di legge di bilancio. Due terzi delle risorse vanno ai redditi medio bassi, al sostegno delle famiglie, ai servizi essenziali per gli italiani; la restante parte contribuisce al sostegno dell'impresa e degli investimenti infrastrutturali. C'è una concreta riduzione della pressione fiscale che avviene attraverso gli otto decreti già approvati della delega fiscale. Allora la dedicammo al presidente Berlusconi, oggi lui andrebbe fiero di un insieme di norme *(Applausi)* che riducono il peso delle tasse e cambiano il rapporto tra il contribuente e il fisco. La manovra conta tante misure di equità verso i bisogni della gente e un'attenzione verso i ceti produttivi, un insieme di norme a cui abbiamo lavorato in lunghi confronti con tutti i componenti della Commissione bilancio, attraverso uno straordinario lavoro di squadra, per rendere questa legge ancor più completa ed equa. A loro e ai tanti funzionari del Senato, che hanno lavorato con noi senza sosta giorno e notte, va il ringraziamento per il grande lavoro svolto. Non riesce a scalfire questa mia grande fiducia neanche l'ironia di chi ha voluto deridere la mia attività di senatore. Rappresento con onore e orgoglio gli interessi di tutti i cittadini, compresi quelli che operano nello sport italiano che, nel complesso, vale circa 80 miliardi di prodotto e 12 di tasse versate. Vado soprattutto orgoglioso di aver guidato in Commissione la squadra dei senatori di Forza Italia che hanno contribuito in modo determinante al conseguimento di importanti risultati nell'interesse esclusivo della Nazione.

all'impronta dell'austerità, poco identitaria; una manovra con tasse occulte. Anche i giornali di centrodestra, quelli che tipicamente supportano la maggioranza così come i diversi giornalisti che vediamo nei *talk show*, danno la stessa opinione. Nessuno dà un'opinione esaltante di questa manovra. Eppure lo scorso anno in quest'Aula avevate detto che la vera manovra sarebbe stata quella del 2024, perché governavate da pochi mesi, mesi, per cui quest'anno avremmo dovuto vedere quei provvedimenti rivoluzionari, da veri patrioti, che invece non vediamo. Oggi vediamo che avete approvato un "pacco di stabilità",

non avranno i fondi per essere rinnovate. Quindi avete messo un cappio al collo al Paese con questo "pacco di stabilità" che

sul cuneo fiscale, perché non avrete i soldi, a meno che non aumentiate le tasse o tagliate la spesa sanitaria. Questo è il futuro. Probabilmente questa manovra così austera in realtà sarà quella meno austera del Governo Meloni, perché probabilmente le prossime saranno peggiori. È questo lo scenario che oggi vediamo con le decisioni che state prendendo in Commissione europea. europea. È vero, viviamo in un'epoca difficile. Noi abbiamo affrontato con il Governo una pandemia mondiale; poi c'è stata la crisi energetica; ci sono state diverse difficoltà. Ma questa è la normalità: oggi siamo in un'epoca purtroppo apocalittica, dove la quotidianità sarà fatta di sconvolgimenti climatici, crisi, guerre. Quindi questa è la normalità. Se dobbiamo affrontare il futuro del nostro Paese, lo dobbiamo fare con misure rivoluzionarie, non con delle misure da zero virgola che non servono a nulla. state solo ritardando la soluzione dei problemi. Noi, a differenza vostra, quando abbiamo governato - ed era sicuramente un periodo peggiore di questo, perché c'era una pandemia mondiale - non ci siamo mai lamentati. Non abbiamo detto che non avevamo i margini di manovra perché,

Dai danni fatti dai Governi di centrodestra abbiamo avuto aumenti di debito pubblico; abbiamo avuto per esempio 5 miliardi in più di debito Alitalia ad Air France. Però non facciamo come fate voi, che parlate solo di banchi a rotelle; ormai è un *must*, non tenendo conto che i banchi a rotelle sono stati scelti dai dirigenti scolastici e non sono stati imposti dal Governo.

una richiesta di tutti i partiti di centrodestra di allargarlo anche alle seconde case unifamiliari, tanto è vero che voi e mezzo Governo l'avete usato per restaurarvi la casa *(Applausi)*. Allora restituite quei soldi oggi, se siete contro il superbonus. Abbiate il coraggio di restituire i soldi che avete preso per restaurare la vostra casa *(Applausi)*, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi che sono pubbliche, e dateli agli esodati del superbonus.

Senatore Trevisi, la prego di rivolgersi alla Presidenza.

miliardi, settanta miliardi sono ritornati nelle casse dello Stato. E questi settanta miliardi dove sono finiti? Cento miliardi sono stati spesi dal Governo Draghi ad oggi per affrontare il caro energia. Quindi, i soldi del superbonus li avete usati per abbattere il costo dell'energia. Il superbonus ha prodotto più incassi, più PIL. Ha prodotto un milione di posti di lavoro. Gente che prendeva i sussidi di disoccupazione ha trovato lavoro. Ha pagato le tasse e versato i contributi. Questo è stato il superbonus: è stata una manovra espansiva che in quell'epoca serviva. L'errore è stato, magari, una volta finita la pandemia,

che ha portato PIL, ricchezza, economia al Paese e che voi oggi utilizzate come scusa, per dire che, se non state riuscendo a mantenere tutte le promesse che avete fatto in campagna elettorale, è perché il superbonus ha pesato.

dei miliardi che Giuseppe Conte ha portato dall'Europa in questo Paese, grazie al PNRR! Con la quinta rata arriveremo a 100 miliardi. Siamo alla quarta e arriveremo a 100 miliardi con la quinta il prossimo anno. Parlate dei costi, che poi sono tutti da dimostrare, e non parlate dei soldi che il Governo Conte ha portato in questo Paese. Anche questa è ipocrisia. Voi trovate solo delle armi di distrazione di massa, perché non avete il coraggio di dire che in campagna elettorale avete sparato un sacco di fesserie e avete ingannato il popolo italiano. Questa è la verità! Voi non avete il coraggio di dire che avete preso in giro gli italiani e oggi trovate queste armi di distrazione di massa! Un Presidente del Consiglio che risponde a un *influencer*: ma non si rende conto che un Presidente del Consiglio dovrebbe stare a un livello più alto? Invece, si abbassa a rispondere a un *influencer*! Evidentemente non avete argomenti. Potete solo continuare a prendere in giro gli italiani, perché non avete scuse e le dovete trovare, ma non dicendo che siete pronti e proponete questo per la soluzione dei problemi. Non avete soluzioni, non avete strategia, non avete nulla. Sapete solo recriminare sul passato e non siete pronti a fare nulla. Siete solo pronti a prendere le valigie e andarvene a casa!

se vogliamo provare a sintetizzare un giudizio, una valutazione su questa manovra di bilancio, io direi che essa rappresenta in modo molto chiaro ed evidente i limiti e l'inadeguatezza di questa maggioranza, sia quanto al metodo sia quanto al merito. Spenderò poche parole sul metodo col quale è stata approvata. In realtà, già in passato, negli ultimi anni - lo sappiamo bene - si era dovuti arrivare a ridosso della fine dell'anno per approvare la manovra, spesso in modo convulso e complicato. Dunque, sotto questo profilo non c'è una grande novità, se non fosse che era stato proclamato con grande enfasi dalla Presidente del Consiglio che questa volta, grazie alla compattezza, alla forza e alla solidità della maggioranza, le cose sarebbero andate diversamente, cioè la manovra sarebbe stata approvata a metà dicembre senza emendamenti. Se questa doveva essere la prova di quella compattezza, di quella solidità e della forza politica della maggioranza, direi che è stato provato l'esatto contrario, visto che anche questa volta verrà approvata a fine anno e dopo un bell'assalto alla diligenza dei Gruppi di maggioranza. *(Applausi)*. Ma non è tanto questo che mi interessa e che interessa agli italiani, quanto ovviamente il contenuto di questa manovra. Molti osservatori hanno parlato di manovra senza anima, grigia, senza slanci, senza grandi prospettive. Io direi che sono giudizi abbastanza generosi. La verità è che si tratta di una legge di bilancio che appare ignorare completamente e banalmente le condizioni del nostro Paese e vorrei anche sperare che sia finita finalmente la stagione della litania della responsabilità dei Governi precedenti. Da una maggioranza che è in sella saldamente al Governo da un anno e mezzo ci si aspetta l'assunzione di una responsabilità finalmente piena e la fine del patetico vittimismo che fa ancora capolino ogni tanto nei discorsi di maggioranza. Parlavo di una miopia, ma vorrei parlare di una cecità di fronte ai problemi e alla realtà in cui si dibatte il Paese e farò tre macroesempi di questi problemi. la crescita economica. L'Italia viene da un periodo di crescita piuttosto sostenuta in uscita dalla pandemia; una crescita che la *premier* Meloni, proprio in quest'Aula, ha ridicolizzato parlando di rimbalzo di un gatto morto, nel senso che anche un gatto morto quando cade rimbalza e sale. Come a dire nessun merito ai Governi precedenti, nessun merito al Governo Draghi che ci ha traghettato fuori dalla pandemia, perché tutti avrebbero potuto ottenere quei risultati dopo il tracollo dovuto al Covid. una simpatica battuta che però, fossi stato nella Meloni, mi sarei risparmiato, perché dopo l'arrivo di questo Governo il gatto giace a terra immobile. La situazione economica attuale del nostro Paese, infatti, è preoccupante e sembra riprecipitarci verso la stagnazione di qualche anno fa. La previsione di crescita di quest'anno è scesa a un modesto +0,7 per cento, cioè meno della Francia e della Spagna. Gli investimenti che avevano trascinato il Paese nel 2021 e nel 2022, crescendo molto di più che negli altri principali Paesi europei, nell'ultimo trimestre mostrano un preoccupante segno meno e la crescita per il 2024 sarà dello 0,5-0,6 per cento, facendoci precipitare al quartultimo posto in Europa. Cosa c'è, allora, in questa finanziaria per stimolare la crescita? crescita? Mi limiterò a riportare a questo riguardo le parole scritte in un documento delle categorie produttive bresciane (parliamo di Brescia, motore economico del Paese). Cosa dicono le categorie produttive in questo documento scritto nero su bianco? legge di bilancio presenta «la sostanziale assenza di misure a sostegno degli investimenti privati e più in generale di una strategia per la crescita e la competitività». Queste sono le parole delle categorie produttive di uno dei motori della crescita del Paese. Tutta la modesta crescita di quest'anno e dell'anno prossimo è basata sul PNNR, quel santo Piano di ripresa e resilienza che Fratelli d'Italia e la sua *leader* Meloni non votarono all'epoca e che oggi, paradossalmente, è la loro ancora di salvezza per garantire al Paese di non precipitare in recessione. Dovrebbe ringraziarci la *Premier* per quanto ottenuto allora contro il suo parere.

sulla giustizia non c'è nulla in questa finanziaria, ma quello che ci preoccupa è che nel piano pluriennale di bilancio è prevista una contrazione del 10 per cento delle risorse assegnate alla giustizia, da 11 miliardi a 10 miliardi di euro, e questo rischia di portare al collasso il sistema. Altro che recupero di efficienza

soprattutto per effetto dell'inflazione molto alta, che ovviamente ha eroso le capacità di reddito, di risparmio e di spesa. Le persone in povertà assoluta son passate dal 9,1 al 9,7 per cento della popolazione italiana, che vuol dire

non c'è nulla per aggredire questo problema; anzi, pochi giorni fa la *Premier* ha rivendicato con orgoglio la misura con la quale è stato abolito il reddito di cittadinanza in favore dell'assegno di inclusione. A prescindere dal giudizio che si volesse dare sul reddito di cittadinanza - anche noi eravamo convinti che avesse bisogno di un robusto tagliando - quella riforma di questa maggioranza si è accompagnata a una riduzione dei fondi destinati al contrasto alla povertà, che ammontavano a circa sette miliardi e sono scesi sotto i sei miliardi. Dunque, aumenta la povertà nel nostro Paese, la *Premier* riduce i fondi per contrastarla e se ne vanta pure. Complimenti! terzo problema di questo Paese riguarda la crisi demografica, di cui si parla tanto. Penso al drammatico calo delle nascite, a cui si accompagna il grande tasso di migrazione dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che rischia di far precipitare il Paese verso un declino economico irreversibile. Sappiamo che questo è dovuto a tanti fattori: i costi eccessivi dell'accesso al *welfare*, dall'istruzione alla sanità, salari bassi e stagnanti. tutte condizioni che rendono sempre più oneroso e difficile per i giovani formare una famiglia, che scoraggiano la filiazione, che incentivano la ricerca altrove, fuori dal nostro Paese, di una promessa di realizzazione che oggi non trovano più e che non viene loro riconosciuta adeguatamente. C'è una sola misura in questa manovra che cerca di affrontare almeno una delle questioni che riguarda il calo demografico, cioè il taglio

Non c'è nulla sulla casa, sul caro affitti, sulla scuola, sugli asili nido, sul costo dei trasporti per gli studenti. C'è poco sulla sanità: come è stato detto, cala la spesa della sanità in rapporto al PIL, con una situazione che rischia di peggiorare nei prossimi anni. Vi abbiamo proposto tanti emendamenti per tentare di invertire questa tendenza. Vi abbiamo proposto misure significative, alcune anche a costo zero per le casse dello Stato, come il famoso salario minimo, che avrebbe potuto dare un orizzonte di speranza, ma non ci avete dato retta. Ci spiegate come intendete invertire questa tendenza al declino se i nostri giovani, i nostri ragazzi, il nostro *welfare,* sono totalmente fuori dalla vostra agenda politica? In conclusione, questa è una manovra che guarda al passato, miope e inadeguata, esattamente come questo Governo.

Signor Presidente, il disegno di legge di bilancio per il 2024 contiene delle misure sicuramente prudenti, responsabili e realistiche. Alla luce delle delicata situazione economica in corso, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi mediorientale, esse sono concentrate sulla riduzione della pressione fiscale, sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, per dare un sostegno vero alle famiglie. Se vogliamo parlare del mondo del lavoro, si conferma il taglio del cuneo fiscale, a cui sono destinati 10 miliardi di euro e che include anche la riforma per l'accorpamento delle aliquote Irpef e l'innalzamento per i dipendenti della *no tax area*. La manovra conferma inoltre la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento, che sono importantissimi, e la soglia fino a 2.000 euro dei *fringe benefit* per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri: si potranno utilizzare anche e soprattutto per pagamento di affitti o mutui prima casa. Insomma, si tratta di misure concrete. Nell'ambito delle attività produttive, è importantissima la previsione di spesa di 190 milioni di euro per il 2024 e di 210 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale, asse portante della nostra economia. Inoltre, il Governo ha rifinanziato con 100 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per la nuova Sabatini, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (il 95 per cento del tessuto imprenditoriale del nostro Paese). Viene incrementata poi la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (110 milioni di euro per il 2024 e 220 milioni per il 2025). Altre risorse importantissime vanno agli incentivi, con meccanismi premiali per le aziende che investono, nonché alle realtà industriali che ritornano a produrre nel nostro Paese, Per le imprese sono stati stanziati circa 1,3 miliardi di euro per le nuove assunzioni e sono previsti incentivi anche per le assunzioni di donne disoccupate.

Numerose e importanti misure poi sono state realizzate per il mondo dell'agricoltura, con le sue 740.000 imprese agricole, ma anche per il mondo della trasformazione, con il rifinanziamento del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti per oltre 600 milioni di euro,

finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro rispettivamente Vengono inoltre ampliati gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a carico del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo che vi rientrino anche quelli compensativi per far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura. Rispetto al passato, il Fondo di solidarietà può

destinati al finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione in campo agricolo, dal punto di vista sia genetico che zootecnico. Per quanto riguarda la famiglia, si interviene con misure in favore della natalità, con la decontribuzione per le madri con due o tre figli strumento Carta Dedicata a te, il cui relativo fondo, dedicato al sostegno delle persone in difficoltà per l'acquisto di beni di prima necessità, è stato anche incrementato. Si è integrato lo stanziamento per il Fondo di garanzia per i mutui sulla prima casa si sono stanziate risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il *bonus* sociale elettricità, per sostenere le fasce più deboli della popolazione anche nel primo trimestre del 2024. Tra le novità,

e non qualche migliaia di persone, con un risparmio a carico delle famiglie italiane di 420 milioni di euro. Il taglio al canone Rai - lo dico senza ombra di dubbio - fortemente voluto dalla Lega, deve essere uno stimolo per un servizio pubblico moderno, competitivo e concorrenziale. Trasformazione digitale e razionalizzazione di reti e direzioni devono essere le parole chiave per la prima azienda culturale del Paese. Il prodotto va differenziato per piattaforme e per genere, che possono anche interagire. La Radiotelevisione italiana non può essere ferma e ancorata a vecchi modelli, deve stare al passo con il progresso e con il mondo che cambia. Stiamo lavorando bene in Commissione di vigilanza Rai in questo periodo, con la Presidente e con tutti i colleghi, e abbiamo visto che c'è una presa di coscienza da parte dei vertici Rai, dell'amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Rossi, ma anche dei direttori dei generi e delle testate. Questo è importante, perché vuol dire un cambiamento, uno stimolo che la Lega ha voluto dare, ma anche un gravare meno sulle famiglie, perché poi agli abbonati corrispondono le famiglie italiane. In definitiva, vorrei ricordare che le misure contenute nel provvedimento hanno un unico obiettivo, in un periodo di grave incertezza costellato da moltissime difficoltà: l'attenzione che deve essere necessariamente rivolta da questo Parlamento e dal Governo sempre ai più deboli della popolazione, alle famiglie, a chi garantisce lavoro. Prima alcuni colleghi hanno esternato dei numeri particolarmente interessanti. Vorrei ricordare a quest'Aula che, tra bonus facciate e superbonus, il costo complessivo che andrà a pagare l'Italia è di 130 miliardi di euro a fine 2023. Dal 2019 ad oggi il reddito di cittadinanza - condivido quanto ha detto prima il collega, e cioè che necessariamente ci voleva un tagliando, ma molto prima di oggi - è costato 30 miliardi di euro. 160 miliardi di euro - non so quale sia il ritorno definitivo, andremo poi a vedere i numeri - che vuol dire sei leggi di bilancio, Presidente. Prendere coscienza di questi dati, per non commettere certi errori in futuro, e avere la responsabilità di accettare gli errori che sono stati fatti dai Governi precedenti

Comincia con l'essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dell'umiltà». Ecco, questa legge di bilancio rappresenta le fondamenta umili, ma efficaci, e tiene conto delle priorità di tutti gli italiani, nessuno escluso. Signor Presidente, vorrei concludere augurando, attraverso la fine di questo mio intervento, buon Natale e buon anno a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per il bene del nostro Paese, compresi tutti i colleghi e le colleghe presenti in quest'Aula, e soprattutto augurando

debole e iniqua, insieme priva di coraggio e di visione. Ci voleva davvero tanta capacità per mettersi contro quasi tutto il Paese. Vi siete messi contro le imprese, che lamentano l'assenza di segni di politica industriale e di sostegno alla crescita degni di questo nome. Tutti i sindacati hanno attaccato la manovra, CGIL e UIL anche con scioperi, nonostante Salvini e il Governo facciano di tutto per colpire questo strumento democratico, mentre la CISL lo ha fatto con altre forme di protesta. I sindacati si battono per le pensioni, per il lavoro, per un salario dignitoso e degno di questo nome, contro la povertà e per la difesa della sanità pubblica. E così ha fatto tutto il mondo delle professioni sanitarie, costretto a scioperare per la dignità del proprio lavoro *(Applausi)*, per il diritto costituzionale dei cittadini a vedere tutelata la propria salute da un servizio pubblico a cui state assestando quotidianamente colpi letali. Ha protestato il mondo della scuola: gli insegnanti e gli studenti che si vedono colpito il diritto allo studio. Un Paese che non investe nella scuola, nella formazione e nella salute, rinuncia al proprio futuro. Avete gestito la vicenda superbonus in maniera irresponsabile, mettendo a repentaglio famiglie e tantissime imprese. Presidente Centinaio, lo dico attraverso lei: presidente Meloni, quando sarete capaci di ascoltare davvero il Paese? Quando vi renderete conto che l'Italia quotidiana è molto diversa dalla bolla propagandistica di Atreju? In questa manovra si danno poi messaggi molto gravi: con i condoni si premia chi non rispetta le regole, chi ha evaso le tasse. Basta: non è giusto che a sostenere il Paese siano solo i lavoratori pubblici e privati *(Applausi)*, i pensionati che hanno le ritenute alla fonte o le tantissime partite IVA e imprese che il loro dovere lo fanno. Questi milioni di persone fanno funzionare i servizi pubblici, mandano avanti il Paese anche per quelli che fanno della furbizia e della violazione di regole la propria prassi quotidiana. Del resto, non ci stupiamo: questo Governo colpisce i *rave*, ma non gli evasori; colpisce gli imbrattatori, ma non chi trucca gli appalti; aumenta pene, carcere per i minori, per le donne incinte o con bambini, ma non colpisce davvero la criminalità organizzata. Di questo purtroppo siamo convinti, altrimenti non avreste tagliato i fondi per la gestione dei beni confiscati; altrimenti non avreste alzato le soglie del contante, con rischi di favorire il riciclaggio; altrimenti non colpireste non colpireste le intercettazioni, ma investireste in tecnologie per contrastare, con strumenti adeguati, mafie sempre più finanziarizzate, globalizzate e tecnologizzate. Lo ricordavano bene, benissimo Enza Rando e Alfredo Bazoli. Avete bocciato tutti gli emendamenti da noi presentati per il contrasto alle mafie, o quelli finalizzati a rendere più efficace la gestione della giustizia italiana, forse perché siete troppo occupati a colpire l'indipendenza della magistratura *(Applausi)* e il pilastro costituzionale della separazione dei poteri. A questo punto voglio dire che è gravissimo anche quanto è accaduto l'altro ieri alla Camera, con un voto che vorrebbe impedire ai giornali di pubblicare fatti e notizie. Questo non è garantismo, che voi praticate solo per i colletti bianchi o per i coinvolti nei casi di corruzione e non lo praticate, invece, per i cittadini colpevoli di reati comuni, o per chi, politici o rappresentanti di ONG, compie il reato di umanità, cercando di salvare persone disperate dall'annegamento in mare. Per questo, anche da qui, vogliamo esprimere solidarietà a parlamentari ed esponenti politici, anche del nostro partito, come Matteo Orfini, Giuditta Pini, Sandro Ruotolo, fatti oggetto di attacchi violenti per questi motivi. *(Applausi)*. Anche noi siamo per le garanzie contro le gogne mediatiche, ma dal vostro provvedimento emana un tanfo che sa di regime, colpisce la libertà d'informazione e rischia perfino di togliere tutele a indagati e imputati. solo una parentesi: permettetemi di protestare, anche come parlamentare dell'Umbria. Oltre ad aver dato l'ennesimo colpo alle speranze degli alluvionati dell'Emilia, a quelli di Ischia e a quelli del terremoto 2016, avete bocciato un nostro emendamento. Era un emendamento semplice: inserire nell'area del cratere 2016 i territori umbri colpiti dal terremoto del 9 marzo scorso.

solidità, semplificazione e velocizzazione alla ricostruzione, ma voi l'avete bocciato. Spero non sia stato perché è firmato da parlamentari di opposizione, ma in ogni caso il colpo l'avete dato non a noi, ma a quei cittadini. Ho concluso, Presidente. Purtroppo voi non siete capaci di fare gli interessi dell'Italia e quello che è avvenuto, per esempio, con l'accordo sul Patto di stabilità o con quello sui migranti a livello europeo lo conferma. Questo Governo mostra i muscoli, ma a livello europeo scontiamo isolamento e paghiamo atteggiamenti e alleanze antieuropeiste. *(Applausi)*. E il pietoso atteggiamento di queste ore sul MES ne è una conferma. Sì, è una manovra piccola

Signor Presidente, io penso che, se qualcuno ci sta ascoltando al di fuori di questa Aula, ha l'impressione che si parli di due Paesi differenti. Da una parte, si dipinge un Paese che va bene, una manovra perfetta che risponde a tutte le esigenze che erano state sollevate - va tutto bene, madama la marchesa - dall'altra parte, critiche aspre e accese. Da che parte sta la verità? Non spetta a me dirlo, anche se io ho un'idea ben chiara e non credo di avere difetti di comprensione quando guardo il Paese. La sanità non va bene, gli stipendi sono al palo, le famiglie sono in difficoltà. Forse qualche critica ve la siete meritata in quest'anno abbondante di Governo, se fuori da qui mille problemi vengono sollevati continuamente e in questa manovra di bilancio non trovano assolutamente alcuna risposta. continuiamo a sentire affermazioni fantasiose da parte di esponenti della maggioranza su banchi su banchi a rotelle, superbonus, fantomatici miliardi di truffe sul superbonus, che non vengono però mai certificati dall'Agenzia delle entrate, che parla di cifre decisamente più contenute e al di sotto di altre manovre. Mi domando se siate affetti da una patologia che vi porta ad essere bugiardi patologici o se siate affetti da analfabetismo funzionale, perché non è possibile che non riusciate a capire neanche quello che dice l'Agenzia delle entrate. Mi soffermerei più sull'idea che siate più inclini alla bugia che alle difficoltà di comprensione. D'altronde membri di questa maggioranza affermarono senza ombra di dubbio che Ruby era la nipote di Mubarak. Veniamo ai contenuti della manovra o meglio a quello che nella manovra non c'è. Non c'è la risposta alle esigenze del Paese, come dicevo prima. Guardiamo per esempio alla sanità. Continuate a dire che non si possono mettere risorse all'infinito nella sanità, che il rapporto rispetto al PIL dà una distorsione, che abbiamo raggiunto cifre mai viste, come ogni anno, sul fondo sanitario nazionale. Se guardiamo dietro di noi, ogni anno c'è sempre stato qualcosa in più dell'anno precedente *(Applausi)*, ma non è abbastanza.

se dobbiamo spendere in sanità, conta la cifra assoluta. Fate pace con voi stessi: o l'una o l'altra. Non può essere l'una quando fa comodo a voi e l'altra quando farebbe comodo ai cittadini italiani.

si è raggiunto un accordo arrivando a definire le spese di difesa come rilevanti spese di investimento da scorporare dal Patto di stabilità.

siano un notevole investimento nella salute dei cittadini italiani che avrà nel futuro un impatto rilevante sui conti del *welfare*, preoccupandoci solo di fucili, cannoni e carri armati. Va bene. liste d'attesa sono il problema più spinoso. Voi che fate? Regalate i soldi al privato, ovvio. Facciamo credere ai cittadini italiani che non c'è altro modo di risolvere questo problema. Facciamo finta di non sapere che in realtà gli altri modi ci sarebbero, come ad l'aumento del personale. Ma no: teniamoci il tetto di spesa, fa così comodo, altrimenti come si fa a fare i favori alla sanità privata e a far credere che la sanità pubblica non funziona e non possa funzionare meglio di così? la quota di privato convenzionato che possono utilizzare le Regioni. Perché invece non usiamo i nostri sanitari e le nostre strutture andando a comprare da noi stessi le prestazioni in *intramoenia*?

con controlli mai fatti e soldi mai incassati rispetto alle prestazioni private fatte dai medici nell'azienda pubblica. In quante altre realtà succede la stessa cosa? Quanti altri soldi i *manager* nominati dalla politica sperperano nella nostra sanità? Volete fare una razionalizzazione? Cominciamo a togliere le nomine alla politica *(Applausi)* e a far fare questo lavoro a chi lo fa obiettivamente, per la sanità pubblica e per i cittadini italiani, invece che favorire sempre i privati. Altro problema italiano: i salari al palo. Non lo diciamo noi, ma lo dice l'INAPP: dal 1992 al 2022, quindi in trent'anni, la crescita dei salari italiani

una quota di contratti collettivi nazionali al di sopra dei 9 euro, ma quelli che stanno al di sotto, quelli che stanno peggio, voi li ignorate sistematicamente. *(Applausi)*. Ce l'avete con i poveri. Ce l'avete con chi è in difficoltà, per fare esclusivamente favori ai potenti, alle banche e alle assicurazioni, in questa legge di bilancio. Questo sapete fare: essere forti con i deboli e deboli con i forti. Questa è la vostra specialità principale. Sempre Inapp ci dice che si è ribaltato il rapporto salari-profitti: da 60-40 a 40-60. Ma questi per voi sono numeri insignificanti. Non riuscite neanche a comprendere per i cittadini italiani che cosa ciò voglia dire. Eppure, vi mettono tutti in guardia sul fatto che questo modello sul lungo periodo sarà insostenibile. Voi state preparando una rivolta sociale e neanche ve ne rendete conto; quella rivolta che era stata neutralizzata grazie all'avvento del MoVimento 5 Stelle, grazie a misure solidaristiche per il Paese come il reddito di cittadinanza, che doveva essere seguito dal salario minimo, accompagnato per dare supporto alle fasce più fragili della popolazione. Invece voi avete affossato tutto e non vi rendete conto di quello che succederà nel Paese nei prossimi anni. Di cose anni. Di cose da dire ce ne sarebbero ancora tantissime, ma i miei colleghi hanno già sottolineato molto. Un'altra misura su cui chiudete sempre gli occhi è

e mai una misura strutturale. Questo è sicuro: alle misure strutturali siete allergici. Anche quando si tratta del supporto psicologico nelle scuole, scuole, non ce la fate a fare quel passo in più verso la risposta alle reali esigenze del Paese. Vediamo tutti i giorni quali sono le richieste dei nostri giovani e voi misure *spot*, come quella fatta dalla Ministra dell'università, che almeno qualcosa fuori dalla tasca ha tirato fuori per queste misure, ma sempre a livello volontario. Mai nulla che dica: si fa così e lo si fa dappertutto, a Pantelleria, a Roma e a Sondrio. No, è sempre un chi vuole può. Davvero grazie. Chi vuole può solo quando pare a voi; poi, quando si tratta di altri generi di volontà, invece no: decidete voi per tutti nella sfera intima delle persone. Dio, patria e famiglia. Questo è il vostro grande *slogan*. Ma quale famiglia? Solo la vostra, ovviamente; per quella di favori ce ne sono tantissimi. Invece, per milioni di famiglie italiane sarà un Natale amaro e un risveglio, l'anno prossimo, ancora peggiore, quando si renderanno conto che le buste paga sono esattamente identiche a quelle dell'anno precedente. Bravi, bravi!

che stiamo varando una legge di bilancio che non porta il Paese verso il futuro. Anzi, è il contrario. Mi sarei aspettata, visto l'andamento dell'economia italiana, una legge di bilancio che innanzitutto puntasse ai fattori della crescita e dello sviluppo nel nostro Paese. Mi sarei aspettata interventi economici importanti, a sostegno della transizione energetica, di quella digitale, delle nostre imprese, con grandi iniezioni economiche rispetto alla formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, per accompagnare, insieme alle imprese, anche la loro trasformazione professionale, il loro aggiornamento. Mi sarei aspettata, vista la stagnazione della nostra economia, di bilancio che innanzitutto puntasse alla ricerca, all'università, alla scuola, per formare le persone, gli uomini e le donne del nostro Paese, e per dotare il sistema delle imprese, anche delle piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro settore produttivo,

rispetto a quali sono i settori strutturali della nostra economia, in cui vale la pena di investire per il futuro del Paese. E mi sarei anche aspettata una legge di bilancio che, accompagnata a una inesistente politica industriale nel nostro Paese, ponesse le basi termine a qualche crisi industriale, non per continuare a sommare, alle vecchie crisi, nuove crisi cui nessuno risponde. È vergognoso ciò che è successo ieri all'incontro sull'Ilva. Io capisco le divergenze interne alla politica. Ci sono sempre state e ci saranno sempre ma non sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici, né tantomeno sul futuro industriale di questo Paese. Immaginiamo, continuamente, senza far nulla, di accompagnare la chiusura della più grande impresa siderurgica del Paese, con quello che produce, anche per le imprese italiane che hanno bisogno di acciaio.

quelli che si stanno avvicinando alla pensione e quelli che, invece, sono molto lontani da quello che ormai è diventato, in in questa instabilità occupazionale continua, non più il momento conclusivo della vita lavorativa. È diventato l'obiettivo della salvezza. Sulle pensioni siete riusciti a fare davvero di tutto e di più. Io sono stata eletta in Sicilia e ho fatto la campagna elettorale in quell'isola, che sarà spolpata, insieme alla Calabria, delle risorse del Fondo per per lo sviluppo e la coesione per il fantomatico Ponte sullo Stretto. *(Applausi)* In Sicilia i soldi che sottrarrete ai siciliani, ai calabresi, alle siciliane e alle calabresi faranno in modo che continuino ad avere e a viaggiare su strade fatiscenti fatiscenti e che la loro linea ferroviaria continui a essere monorotaia. Ebbene, in quella campagna elettorale ho ascoltato le parole di molti partiti della maggioranza, quando rassicuravano le elettrici e gli elettori che il reddito di cittadinanza sarebbe rimasto - perché questo dicevate in campagna elettorale - ma ancor di più, che avreste cancellato la cosiddetta legge Fornero. Quante persone hanno dato il voto ai partiti di questa maggioranza certe, dalle dichiarazioni e dai comizi, che questo si sarebbe avverato? Ebbene, siete riusciti in un capolavoro che onestamente, da persona che si è occupata di questi temi, non avrei mai immaginato che qualcuno potesse riuscire a fare. Avete di molto peggiorato la riforma Fornero. Dovete delle scuse alla professoressa Fornero per tutto quello che avete detto e quello che oggi avete deciso di fare. *(Applausi)*. Avete peggiorato la pensione per tutti.

Siete riusciti a peggiorare l'APE sociale per quei lavoratori e quelle lavoratrici che hanno grandi problemi di salute

Avete deciso che oltre il rinnovo del contratto di lavoro per i lavoratori sanitari - e ci mancherebbe anche che non lo si danno un po' di soldi in più ai privati, non alle strutture pubbliche, per le liste d'attesa. Quante persone devono ancora morire nel Paese perché non hanno il diritto alla cura? *(Applausi)*. È possibile che nemmeno la pandemia abbia spiegato come un Paese privo di sanità territoriale vede i poveri morire più facilmente e prima degli altri? altri? Chi è abbiente può utilizzare la sanità privata, ma chi è povero può solo o pregare e credere in un miracolo o morire prima. Poi sul sociale faccio solo una battuta per economia dei tempi: vi ricordate tutto il dibattito sul disegno di legge sugli anziani, su come volevamo valorizzare la figura degli anziani? L'unica cosa che avete fatto

Sarebbe stato più giusto, avrebbe dato più dignità a questa manovra che, signor Presidente, è una manovra recessiva, che non guarda il futuro e rende le diseguaglianze più insopportabili nel nostro Paese.

siamo qui oggi per discutere uno dei provvedimenti più importanti dello Stato, cioè il disegno di legge di bilancio, su cui c'erano molte aspettative, soprattutto per quanto riguarda la sanità e tutto il personale medico e sanitario. Posso dire in tutta tranquillità che non ne avete veramente azzeccata una. *(Applausi)*. Quando è apparso il vostro testo e abbiamo letto quella che dovrebbe essere la vostra ricetta per salvare il nostro Servizio sanitario nazionale,

insufficienti risorse sul fondo del Servizio sanitario nazionale, insufficienti risorse per il rinnovo dei contratti; misure non efficaci per abbattere le liste d'attesa. Mentre le risorse per le armi o per il Ponte sullo Stretto di Messina le avete trovate, vi siete dimostrati totalmente inadeguati per quanto riguarda la sanità. Era chiaro che bisognava intervenire in Commissione per aggiustare le cose e, visto che la maggioranza aveva ricevuto l'ordine di non fare emendamenti, tutte le aspettative si sono riversate sulle minoranze. Abbiamo cercato di farvi capire cosa non andasse bene, raccogliendo le osservazioni di associazioni e sindacati, che nel frattempo hanno cominciato ad indire scioperi e continuano tuttora a farli, perché i lavoratori si sentono presi in giro, perché le risorse per il rinnovo del contratto non sono sufficienti. Ve lo stanno dicendo tutti ed è sufficiente prendere una calcolatrice e fare due conti per capirlo, però voglio aiutarvi anche in questo.

Torniamo però al 5 dicembre 2023: mentre accadeva tutto questo, il ministro Schillaci a una domanda su cosa pensasse dello sciopero, quindi della sofferenza di medici e infermieri, sempre più costretti a scappare via dall'Italia, ha dichiarato: «Mi indichi una sola volta in cui i medici siano rimasti soddisfatti. In base a ciò che rivendicano oggi, comprendo che siamo sulla strada giusta».

poi devo ricordare un'altra intervista, c'è quella al direttore generale dell'INPS Caridi sul taglio delle pensioni di medici e infermieri, in cui ha dichiarato: «In generale, credo che incoraggiare i lavoratori ad andare in pensione più tardi sia sempre un bene per la sostenibilità dei conti pubblici».

Siamo tutti d'accordo che fare l'impiegato o il senatore non è la stessa cosa che andare su un'impalcatura o lavorare in un reparto ospedaliero, vero? Penso che qui dentro spesso si perda il contatto con la realtà, quindi su questo siamo tutti d'accordo.

Qui si capisce dove volete andare, perché portare a lavorare questo personale fino a sessantasette anni all'interno dei reparti ospedalieri e delle RSA vuol dire aver perso il contatto con la realtà.

le più colpite sono le donne. Prendendo come esempio l'Emilia-Romagna, il 32 per cento degli infortuni sul lavoro denunciati riguarda gli infermieri. Capite perché non va bene giocare con le pensioni di queste persone? Capite perché questo personale medico e infermieristico anche in questi giorni è in piazza? Io credo di speriamo che abbiate capito questo caso. Comunque, andiamo avanti: vogliamo parlare di liste d'attesa? La vostra ricetta è la detassazione degli straordinari e l'aumento delle prestazioni aggiuntive. Lo sapete, vero, che una giornata è fatta di

Vi comunico che sulle loro spalle in esclusiva c'è già il carico dell'inefficienza delle Regioni nella gestione della sanità, dove i vostri piani sociosanitari raschiano il fondo del barile con l'antipatico sistema del minutaggio per calcolare il fabbisogno del personale nelle strutture. Vi ricordo anche che è sempre più frequente il ricorso alle esternalizzazioni, che troppo spesso corrisponde a personale sottopagato, che lavora in condizioni peggiori: è uno dei motivi per cui le persone in questo ambiente non vogliono più andare a lavorare e si stanno licenziando. Nell'intento di avviarmi alla conclusione, signor signor Presidente, ho solo una domanda, che, per suo tramite, vorrei far arrivare alla maggioranza e al Governo, che mi sto ponendo in questi giorni: se qui nel nostro Paese dovesse ripresentarsi un'emergenza sanitaria, quello che mi chiedo io è: con che faccia andrete a chiedere a medici e infermieri di sacrificare la loro vita

insieme all'inizio di agosto in quest'Aula, con l'approvazione della delega fiscale. Sarebbe meglio dire l'avete posto, perché in quell'occasione il Partito Democratico votò convintamente contro la delega. Allora Governo e maggioranza festeggiarono, dicendo che avevano fatto la rivoluzione fiscale. Mese dopo mese, decreto attuativo dopo decreto attuativo, quell'afflato rivoluzionario è precocemente appassito; e verrebbe da dire per fortuna, visti i principi ai quali si ispirava. Quello che permane è invece il segno e la direzione di marcia, il modello di patto fiscale che che condivide un'idea di patto sociale che quelle misure prefigurano. Ed è un modello sbagliato, perché profondamente iniquo e particolaristico nella sua definizione. La bandiera della *flat tax* non ha trovato abbastanza vento e si è rattrappita convertendosi, nella legge di bilancio, nella rimodulazione delle aliquote degli scaglioni, che passano - come sapete - da e nell'incremento delle detrazioni per lavoro dipendente, nell'abbattimento, per i redditi superiori a 50.000 euro, di 260 euro su una serie di detrazioni. Per fortuna avete fatto marcia indietro sulla cancellazione delle detrazioni per le erogazioni liberali al terzo settore *(Applausi)*, misura veramente indegna per un Paese che fa del terzo settore un pilastro sussidiario del *welfare* e della solidarietà dell'Italia. Questa rivoluzione, poi, è anche a tempo determinato. Come è noto, la riduzione degli scaglioni è finanziata solo per il 2024. 2024. Non solo quale rivoluzione, ma quale riforma può essere quella che si dà un orizzonte temporale così breve? La scelta di introdurre in legge di bilancio misure valide solo per un anno, come anche nel caso dell'abbattimento del cuneo fiscale, che affrontano quindi singoli aspetti della tassazione, interessando platee sempre più limitate di contribuenti, piuttosto che concentrare le risorse su interventi organici e strutturali, aumenta la complessità del sistema e peggiora le criticità esistenti, i costi amministrativi e di adempimento, anche per gli enti territoriali, che saranno costretti a ricalcolare le proprie aliquote per un solo anno, con costi di personale e procedurali che tutti gli amministratori locali che siedono in questo Senato potranno riconoscere. Sarà forse per questa ragione, per la complessità conseguente alle scelte che avete fatto, che il decreto sull'Irpef martedì scorso è entrato in Consiglio dei ministri, ma non ne è uscito? *(Applausi)*. Avete rimandato al prossimo Consiglio dei ministri l'approvazione del decreto che stiamo finanziando con la legge di bilancio che probabilmente approveremo nella giornata di domani. Anche il vantaggio fiscale derivante da questa operazione può risultare estremamente variabile, se si tiene conto della presenza di detrazioni per oneri e addizionali regionali e comunali. Dunque il vantaggio fiscale medio sarà di 175 euro per famiglia, con un massimo di 260 euro per i più fortunati. Presidente, chiedo ai colleghi, tramite lei, quale utilità può avere un risparmio di questo tipo per una famiglia di ceto medio, quando un esame diagnostico ormai comune (mettiamo una colonscopia), che è impossibile ottenere se non con un'attesa di mesi, se non anni, dal Servizio sanitario nazionale, costa ben più di 175 euro. Non era meglio utilizzare quei quasi cinque miliardi di euro che finanziano l'operazione Irpef per la sanità, o facendo un'operazione di maggiore equità destinata a tutti i cittadini e a tutte le famiglie? Quello sull'Irpef, Presidente e colleghi, è un intervento finalizzato esclusivamente a tenere alta una bandiera, quella della *flat tax*, che voi avete promesso in campagna elettorale, che se resa effettiva, non potrebbe che tradursi in tagli brutali al *welfare* e alla sanità, come dimostrano tutti i Paesi e tutte le economie dove questa misura veramente implementata. Non si tratta di modelli di equità sociale o fiscale, a cui guardare; spesso si tratta di Paesi che hanno dei problemi anche con la democrazia. D'altronde, Presidente, domandiamoci perché, ma soprattutto per chi dovrebbe essere desiderabile un fisco che fa parti uguali tra disuguali? Già decenni fa il maestro di Barbiana, don Milani, ci ha spiegato che fare parti uguali tra disuguali è la più crudele delle ingiustizie. *(Applausi)*. Perché dovremmo desiderare di inserire questo principio nel nostro sistema e nel nostro modello fiscale, per avvantaggiare soltanto una parte della società? È un'ottica sempre più particolaristica ed è il principio a cui si sta ispirando tutta la delega per la riforma fiscale. La rivoluzione da fare sarebbe quella contro l'erosione fiscale, che deriva da una fuga continua e di lungo periodo dall'Irpef e dalla progressività fiscale, che invece è sancita dalla Costituzione. La moltiplicazione dei regimi separati e cedolari avvantaggia la rendita finanziaria o immobiliare a discapito del lavoro e del profitto, anche degli introiti da attività produttive. Anche gli economisti liberali, senza dover arrivare a Keynes, sapevano che questa è la strada che porta un'economia al declino. In effetti, sugli stimoli alla crescita, il disegno di legge di bilancio ha voltato la testa dall'altra parte. economica), le imprese danno al bilancio molto più di quanto non ricevano e non basta la nuova Sabatini a invertire questa tendenza. I saldi lo dicono chiaro

L'ACE costituisce un incentivo permanente alla patrimonializzazione delle imprese e la sua abolizione, senza correttivi, aumenterà il costo degli investimenti, autofinanziati in un momento in cui gli alti tassi di interesse, come ben sapete, rendono proibitivo il ricorso al credito bancario. Il tutto accade in mancanza di una strategia di politica industriale e di un disegno complessivo sulla crescita, come dimostra anche la cattiva *performance* che il Governo ha fatto nella giornata di ieri con i sindacati rispetto alla vicenda Ilva. Inoltre, la previsione di 20 miliardi di liberalizzazioni, se non fosse irrealistica, sarebbe da temere, sarebbe preoccupante e tragica, in una fase geopolitica in cui tutte le grandi economie nazionali tengono e si conservano i propri *asset* produttivi, i propri campioni nazionali. È un momento in cui è necessario investire con forza su crescita, investimenti e attività produttive del Paese. Questa sarebbe la vostra patriottica attenzione verso i produttori nazionali? Non riusciamo a scorgere il disegno e una strategia in questa legge di bilancio: questo è preoccupante, non per l'opposizione ovviamente, ma per il Paese. La legge di bilancio si può dire che abbia drammaticamente smarrito la via dell'equità prima e della crescita dopo, per le ragioni che ho detto. In tutta sincerità, Presidente, noi abbiamo invece smarrito la presenza del ministro Giorgetti *(Applausi)* che in passaggi delicati, come la discussione in Assemblea o le ore notturne trascorse dai colleghi in Commissione, non si è mai visto.

contrariamente a quanto invece volete far passare. Vorrei intanto ringraziare il Presidente della Commissione bilancio, i relatori e tutti i colleghi per il lavoro svolto nelle numerose sedute per l'approvazione del bilancio. Ci accingiamo a concludere un anno complesso, che ha visto la necessità di interventi da parte del Governo per fronteggiare diverse criticità emerse nel corso dell'anno. Pensiamo, alla siccità e all'alluvione. Tra poco voteremo la legge di bilancio per il 2024 e le poche risorse di cui disponiamo sono state concentrate in generale su interventi che ricadono direttamente sulle famiglie, in modo particolare su quelle maggiormente in difficoltà. Si è lavorato per difendere il potere d'acquisto a fronte dell'aumento del costo della vita, unitamente al sostegno alla crescita. Una manovra concreta che non disperde risorse perché non ce lo possiamo permettere e, contrariamente a quanto qualcuno vuol far passare, non contiene mance o mancette, ma indirizza gli sforzi su grandi temi, dandosi delle priorità. Mi consenta, Presidente, di tranquillizzare il collega Io non ho ristrutturato la casa con il superbonus 110 per cento e direi che se hanno del tempo da perdere per andare a spulciare quanto i colleghi denunciano, vuol dire che proprio non sanno come spendere meglio il loro tempo. Mi piace anche smentirlo sul fatto di attribuire la scelta dei banchi a rotelle ai dirigenti scolastici. Vorrei ricordare che il bando per l'acquisto dei questi banchi a rotelle arriva dal commissario Arcuri ed è proprio l'ex ministra Azzolina a rivendicarne la scelta, definendoli una grande innovazione per il Paese e ritenendolo un investimento dello Stato sugli arredi, cosa che non avveniva da anni. Ebbene più che definire un investimento l'acquisto dei banchi a rotelle per 400 milioni di euro, lo definirei uno spreco di denaro pubblico, visto che si sono rivelati inutili, inadatti e dannosi, finendo nei magazzini. Direi per fortuna per gli studenti,

nelle priorità troviamo l'aumento degli stipendi per il comparto difesa e sicurezza, a cui aggiungere la copertura per la stipula di polizze assicurative riguardo la copertura sanitaria ed infortunistica complementare; dettaglio non secondario in quanto il comparto è escluso dalla copertura INAIL. Viene definita anche una quota destinata al salario accessorio, che riguarda in modo particolare il pagamento dello straordinario per le Forze armate e la Guardia di finanza. Sono state destinate risorse anche per le pensioni dei lavoratori del comparto difesa e sicurezza, aumentando il coefficiente di trasformazione del montante contributivo che vedrà pensioni più alte. Quello fatto oggi è un primo passo, consci di dover mettere mano a quello che nel giro di poco tempo potrebbe diventare un problema serio e che le risorse messe a bilancio bastano per qualche anno. Il nostro ordinamento infatti riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativi richiesti. L'obbligo - ripeto, l'obbligo - per il comparto di ritiro dal lavoro a sessanta-sessantadue anni ha come conseguenza minori contributi versati e quindi pensioni più basse, visto che per il loro calcolo si va verso il sistema contributivo puro. Tale personale risulta svantaggiato proprio sul versante previdenziale in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo previsto dalla legge n. dalla legge n. 335 del 1995. Ciò determina una penalizzazione per chi si è arruolato dopo quella data e comporta una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato per il quale sono state trovate idonee risorse e ha permesso di attivare i fondi necessari a una compensazione. Per questo motivo sono state depositate in Parlamento più proposte di legge da diversi partiti. La Lega ne ha presentata una, a mia prima firma, a dimostrazione della consapevolezza del problema. Credo che garantire un trattamento pensionistico adeguato a questi settori... non possono essere penalizzati proprio a causa della specificità, della peculiarità del loro ruolo, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, sia un modo per dire loro grazie per quanto fanno ogni giorno. Nonostante abbiamo assistito a una politica che spesso si è vergognata a parlare di difesa e di militari, quando però si è di fronte a un'emergenza, quando la normale macchina organizzativa statale va in tilt o non riesce a fronteggiare situazioni al di fuori della normalità, allora la difesa e i suoi uomini vengono chiamati in soccorso, e li troviamo sempre pronti a rispondere a tutte le chiamate. Lo possiamo vedere anche con il personale dell'operazione Strade sicure, presente nelle stazioni, nei luoghi sensibili, a supporto delle prefetture. Qualcuno - il Governo Conte II - aveva stabilito un processo graduale di riduzione. Questo Governo, invece, tale processo di riduzione lo ha invertito, portando a un incremento del personale di 1.000 unità. Per noi, a differenza di voi, la sicurezza è al primo posto. Mi lasci concludere facendo gli auguri di buon Natale e di un buon 2024 a tutte le famiglie italiane, in modo particolare a tutti gli uomini e alle donne in divisa. Un ultimo passaggio. Il presidente Meloni non ha bisogno della mia difesa, visto che prima è stata tirata in causa sul fatto di aver risposto a una *influencer*. Ebbene, anch'io ho criticato l'*influencer* per aver utilizzato una una carità pelosa per trarne vantaggio. C'è chi critica certi personaggi, c'è chi invece li sceglie come propri portavoce.

Ma vi siete incartati da soli e ancora una volta siamo qui oggi a discutere senza che ci sia stata la possibilità di un confronto di merito sulle scelte strategiche che il Paese deve affrontare: questo dovrebbe essere la manovra di bilancio. Siamo di fronte a un Paese che con la destra frena, perché questo ci dicono i dati, a prenderli sul serio. Oggi ci troviamo una manovra che sovrastima la crescita e in cui sono assenti misure espansive; una manovra senza visione: questa è la verità. Altro Altro che *made in Italy*: non c'è nulla per le imprese e c'è un piano di privatizzazioni per oltre 20 miliardi. Quello che rimane concretamente anche del tanto citato aiuto alle famiglie sono misure *spot* che non intervengono a sostenere davvero le scelte di genitorialità, tanto meno la condizione delle donne; anzi, rischiano di acuire le diseguaglianze territoriali. Una manovra senza visione e iniqua. Si configura una destra delle diseguaglianze territoriali di genere e generazionali, un accanimento contro i diritti alla salute, all'istruzione, al lavoro. E così rimane l'Italia dei privilegi, perché l'opposto di diritto è privilegio. Invece di rafforzare l'assegno unico, di investire sui servizi educativi, di finanziare la non autosufficienza (questo significa aiutare le famiglie), di raccogliere la sfida che anche qui vi abbiamo lanciato con un emendamento sui congedi paritari per sostenere la condivisione del lavoro di cura nelle famiglie, le misure rivolte alle donne aggiungono qualcosa, ma mai in modo strutturale e solo a quelle che già hanno figli, almeno due, con buona pace delle altre che non possono farli perché le condizioni economiche non lo consentono o che non li desiderano. Nulla, appunto, si investe sul sistema dei servizi educativi da zero a sei anni, quindi sui diritti delle bambine e dei bambini. Anche la decontribuzione ed un piccolo e non strutturale intervento per le mamme, non tutte, che lavorano e hanno due o tre figli: una minoranza di donne che vivono al Centro Nord, dove già nascono più bambini e bambine dove già è più alta la frequenza del nido. Vorremmo, infatti, sommessamente ricordare che uno dei problemi delle famiglie è la scarsa presenza di servizi, soprattutto nel Mezzogiorno. Vorremmo anche dire che il vero nodo di questo Paese, che blocca anche la natalità, è il lavoro per le donne. Ma mai si interviene sulla precarietà. Avevamo anche proposto, con un emendamento che ha ricordato anche la collega Camusso, un fondo per andare a vedere che cosa significano quelle dimissioni volontarie, quelle 40.000 donne che lasciano il lavoro perché non riescono a conciliarlo con i bisogni della loro vita, e per proporre misure di flessibilità. *(Applausi)*. Ma nulla si è potuto discutere e queste misure le lasciamo alle aziende più illuminate, invece di sostenere un *welfare* universale, che faccia anche promuovere i *welfare* aziendali. Invece, altre diseguaglianze nel mondo del lavoro. Per non parlare degli interventi sulle pensioni, che restringono ulteriormente, rispetto a Opzione Donna, la platea di chi potrà beneficiare della misura, con buona pace del riconoscimento del contributo dato dalle donne a questo Paese. In fondo, infatti, a voi basta il successo di alcune, un soffitto di cristallo che si rompe, ma di dove finiscono i cocci e del destino di tutte le altre non vi interessa nulla, perché quello che non perseguite è l'eguaglianza.

e di istruzione. È un circolo vizioso: tagli, diritti negati, disoccupazione femminile, donne che sono il *welfare* del Paese, ma a cui non date la possibilità di scegliere davvero. Il Governo ha scelto *spot* di corto respiro. riforme a scadenza, persino la riforma fiscale. È un Paese che non sa cosa succederà domani. Del resto, così si va avanti sulla scuola, con riforme improvvisate, come la filiera tecnico professionale che abbiamo licenziato stamattina in 7ª Commissione o il liceo *made in Italy,* che abbiamo votato ieri, che dovrebbero essere già pronti a gennaio, per l'anno scolastico 2024-2025. Una modalità improvvisata di intervenire su un settore strategico e delicato come quello dell'istruzione, dove nulla avete messo per sostenere i meritevoli, anche privi di mezzi, perché il vostro merito è la selezione di chi è più forte. Ma il Governo ha bisogno di *spot* di corto respiro, che non invertiranno alcuna tendenza economica e demografica, che nulla miglioreranno nella vita di tante ragazze e donne disoccupate e lavoratrici, precarie e non. Cultura, scuola, università. Questa destra ha scelto di non ascoltare i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, di tradire la riforma dell'indennità di discontinuità. Ha scelto di non ascoltare gli studenti e le studentesse, i ragazzi delle tende, che hanno sollevato per tutti il tema del caro affitto. Questa è una manovra sorda al futuro anche su questo Studiare è sempre di più un lusso, come ci hanno spiegato anche Federconsumatori e l'Unione degli studenti universitari nel *report* «Universitari al verde», specialmente se si fa lontano dalla propria città di residenza. Mediamente, si spende, per materiale, tasse, alloggio, passi, trasporti: più di 9.000 euro annui se in sede, più di 10.000 se pendolari, più di 17.000 per i fuori sede. Ancora una volta, altro che capaci e meritevoli. Nulla su queste domande, nulla sul diritto allo studio. Nulla sul *welfare* studentesco, poco per il Parlamento. Qui vi abbiamo sfidato. Rinunciate ai piccoli interventi localistici, alle mance; proviamo, insieme, a fare un'operazione che affronti una priorità del Paese. Insieme, uno scatto di orgoglio di un Parlamento silenziato nella possibilità di intervento. Le opposizioni lo hanno fatto, affrontando la violenza maschile contro le donne. Non solo norme servono contro la violenza, e non solo norme penali, ma misure politiche. Formazione, per non sottovalutare mai più il rischio che una donna corre, come ancora è successo per la morte di Vanessa Ballan. Non ne possiamo più di denunciare la sottovalutazione del rischio. Per questo abbiamo chiesto fondi per la formazione delle operatrici e degli operatori. milioni in spesa corrente che consolideranno i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, rafforzando il reddito di libertà e l'inserimento lavorativo delle donne che hanno subito violenza, violenza, oltre alla rete dei servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, perché c'è sempre troppo poco per questo, e alla formazione, per cui non siamo riusciti a ottenere i soldi nell'ultima legge che abbiamo approvato, ma che come opposizioni vi abbiamo imposto nella legge di bilancio, e alla costruzione costruzione di case di rifugio. Non siete stati capaci di fare con noi queste scelte; vi siete chiusi nel cortile di casa vostra, perché questo è il segno di questa manovra senza visione e senza futuro, per un'Italia dei privilegi.

Presidente, la legge di bilancio non è soltanto un documento contabile fatto di numeri e di tabelle. La legge di bilancio è un po' il riflesso della sensibilità del Governo, delle reali priorità politiche e sociali di un Governo. Non è importante soltanto ciò che si fa, ma è importante anche capire quello che si trascura. Quello che salta all'occhio è che la prima cosa che avete trascurato sono proprio le promesse elettorali. Risulta evidente che avete costruito una campagna elettorale sull'illusione; il vostro programma era costruito sul nulla. Avete dichiarato di essere pronti a governare e state dimostrando di essere capaci di comandare, incapaci di governare e soprattutto incapaci di portare a termine e di rispettare le promesse che avete fatto. Con grande disinvoltura avete parlato di una *flat tax* al 20 per cento, avete parlato di 1.000 euro per tutti i pensionati, 1.000 euro con un *clic*. Ora tutte queste illusioni vi stanno crollando sotto i piedi come un castello di sabbia e adesso ci volete dire che la coperta è corta? Presidente, non ve lo potete permettere di dire che la coperta è corta, perché lo sapevate già ed è un'offesa all'intelligenza degli italiani.

rappresentate: state smantellando lo Stato di diritto attraverso riforme istituzionali che ci stanno indirizzando verso una deriva autoritaria che sta cancellando la democrazia rappresentativa. State smantellando lo Stato sociale. Allora andiamo a vedere qual è la verità, perché alle parole qui si sostituiscono i fatti. La legge di bilancio ci sta mettendo di fronte a una verità che non è quella che voi raccontate in giro. Andiamo a vederne alcuni, di questi fatti. La verità ci sta dicendo che aumentate la cedolare secca sugli affitti, se sulle seconde case. Va benissimo, ma state penalizzando i *bed and breakfast* e quelle persone che magari vivono solo di questo. Non pensiate che gli affitti siano soltanto quelli che si pagano nella Capitale: nei piccoli centri urbani, con un paio di affitti non ci si sbarca il lunario. State cancellando il superbonus per beceri motivi politici, sapendo benissimo di mettere in difficoltà migliaia di imprese.

Che cosa ci volete dire? Che non vi volete occupare nemmeno di questo? Volete privatizzare la sanità e non vi occupate delle catastrofi naturali. Allora mi dite per quale motivo i cittadini vi dovrebbero pagare le tasse?

adottate misure di sviluppo nelle aree del Paese economicamente depresse. Li avete respinti, ma le aree economicamente depresse non sono soltanto le Regioni del Sud, ci sono anche - se ve ne siete accorti - le aree di crisi industriale complessa. Queste ultime, signor Presidente, non sono soltanto al Sud, ma sono geograficamente distribuite su tutto il territorio nazionale, come lo sono anche le aree economicamente colpite dalle catastrofi naturali, che d'ora in avanti si dovranno arrangiare da sole. Si dovranno pagare loro la polizza e anche nella sanità vedrete che ci farete pagare una polizza sanitaria, perché non siete capaci di coprire quelle spese. State dimostrando di saper comandare e di non saper governare. Allora fate un piccolo sforzo, provate a copiare dagli altri Paesi: guardate guardate cosa succede in Europa, guardate cosa fanno l'Irlanda e la Spagna, guardate quello che ha fatto la Germania, non oggi, ma già dopo la caduta del muro di Berlino. Tutti si stanno muovendo per risolvere le crisi economiche a partire dalle aree economicamente depresse, tranne voi. voi. Questo però non ci sorprende. State usando una politica in cui, invece di risolvere i divari territoriali, cercate di spaccare il Paese con questa folle idea dell'autonomia differenziata, che oltretutto creerà un'Italia arlecchino in cui cinque Regioni si occuperanno dell'istruzione, altre cinque dei trasporti e ognuno farà un suo piccolo feudo in cui le regole saranno diverse da una Regione all'altra. voi è questa la soluzione; non vedete ciò che chiede l'Europa, quello che vogliono fare gli altri Paesi. Io però non mi sorprendo perché la vostra indifferenza verso i deboli, la vostra indifferenza verso i territori in difficoltà, ha una linea di coerenza con le vostre politiche, perché volete sempre fare i forti con i deboli e i deboli con i forti. Non ci avete dimostrato di saper governare,

provo a riavvolgere le lancette del mio orologio di quarant'anni e tornare sui banchi dell'università, quando studiavo economia politica. Ricordo che il professore di economia politica con i suoi disegnetti ci spiegava bene il meccanismo della domanda e dell'offerta

Se quei libri non li volete studiare, imparate dall'esperienza, vedete quello che è successo in Grecia, in Spagna e quello che è successo in Italia quando abbiamo applicato politiche di *austerity*. Ricordo anche che quel professore ci diceva che a questa regola non sfuggono neppure le aziende: se un'azienda è in crisi e i suoi prodotti non si vendono, comincia a tagliare le spese e a ridurre la produzione, si avvia verso la chiusura; se vuole rimettersi sul mercato, deve investire nell'innovazione, deve rinnovare i prodotti, investire in comunicazione, spendere oggi per poter guadagnare domani. Nella vostra banale semplicità, pensate che sia molto più semplice spiegare che quando ci sono troppe spese bisogna tagliare. Io non Io non sto dicendo che non dovete tagliare; il problema è che voi state sbagliando su cosa decidere di tagliare: voi tagliate sulle pensioni e sulla sanità, dovete tagliare sugli sprechi e la corruzione *(Applausi),* perché quando il MoVimento 5 Stelle ha portato in Aula lo spazza corrotti vi siete messi di traverso. Non la volevate quella legge; eppure, grazie a quella legge, oggi in Europa ci dicono che abbiamo fatto passi avanti.

alla conclusione, signor Presidente, la legge di bilancio deve essere un modo in cui il Governo ascolta le esigenze di tutti i cittadini. È una legge che non deve soltanto bilanciare i conti, deve creare equilibri economici e sociali, deve rimuovere le divergenze territoriali, deve risolvere i problemi del Paese. Anche sulle infrastrutture, se si investono 11 miliardi soltanto per una infrastruttura e si lasciano a secco tutte le altre Regioni, come quelle del Centro che hanno problemi enormi e che non riescono ad attirare investimenti proprio per carenze infrastrutturali, si sta utilizzando quella coperta corta per coprire un solo problema dell'Italia e questo non è il comportamento di quello che dovrebbe essere il buon padre di famiglia. perde di vista il bene comune, rischia di far precipitare il Paese in un abisso di ingiustizia e di disuguaglianza senza confini. Ora voglio ritornare al discorso di apertura: dietro quelle tabelle, quei numeri e quelle proiezioni, signor Presidente, c'è la vita reale delle persone e ci sono gli uomini e le donne che hanno difficoltà; c'è la realtà. Ecco,

che anche ascoltando gli interventi dei miei colleghi in questi giorni non ho potuto non notare un sostanziale cambio di tono e di contenuto. Un anno fa le forze di minoranza e di opposizione si cimentavano in argomentazioni nel merito dei provvedimenti; in questi giorni, invece, la sottolineatura si focalizza molto anche sul metodo. Dopo un anno abbondante di lavori di Assemblea e di Commissione, è oramai evidente a tutti che in questa istituzione le parole dell'opposizione rimbalzano contro un muro di gomma, che ormai è pura utopia pensare di intervenire nell'ottica di un costruttivo dialogo parlamentare, perché questa maggioranza si è rivelata totalmente sorda e cieca, supponente e prepotente. Nella trattazione in Aula si è arrivati al punto che in sede di manifestazione del parere sui vari emendamenti, il Presidente chiede espressamente al relatore di evidenziare eventuali pareri favorevoli, piuttosto che esprimere un puntuale parere contrario su ciascuno. Parere del relatore? Contrario. Governo? Conforme. Votazione: respinto. *(Applausi)*. È questa la litania che inesorabilmente si ripete oramai da più di un anno, fine di una discussione che in realtà non è mai iniziata. Neanche nella precedente fase di trattazione in Commissione, infatti, vi è traccia di una seria e approfondita discussione. Gli atti compaiono dal nulla, improvvisamente: entrano nelle aule delle Commissioni con scadenze talmente ravvicinate da uscirne con la stessa velocità con cui vi sono entrati, spesso trovando impreparati gli stessi relatori a cui sono stati assegnati. E se si osa provare a entrare nel merito, ci si scontra con la vacuità delle risposte di chi a volte pare non sapere bene di cosa si stia parlando.

se si stesse trattando di una questione mia personale invece che della gestione della cosa pubblica: imbarazzante e sintomatico del grado di approssimazione e di prepotenza con cui vengono licenziati atti che poi regolamenteranno e condizioneranno la vita degli italiani. Ho già evidenziato in altre occasioni che in questo modo si viaggia col paraocchi e che l'ascolto di un altro punto di vista non può che portare vantaggio alla qualità degli atti. Parole al vento, come dicevo prima: gli scranni sono vuoti e i giochi sono fatti, perché perdere tempo ad ascoltare? Peraltro, cosa ci si deve aspettare da un Governo che azzittisce i propri stessi parlamentari, impedendo loro di proporre modifiche al testo della legge di bilancio, e che fa un uso spropositato della fiducia? Devo dire che la delusione circa l'operato della Presidenza del Consiglio, incarnata dalla signora Giorgia Meloni, ha superato le mie aspettative. Sbagliando, confidavo nel fatto che una donna avrebbe saputo essere inclusiva, pur rimanendo fedele al programma elettorale con cui si è presentata agli italiani; e invece, né l'uno né l'altro. Voglio solo rammentare qui, per correttezza e con soddisfazione, che è stata accolta la proposta comune delle opposizioni di destinare alla lotta contro la violenza di genere la propria quota del fondo per le modifiche parlamentari, il cosiddetto tesoretto, che ammonta a 40 milioni di euro, un'allocazione di risorse su un capitolo trascurato dalla legge di bilancio e invece meritevole di attenzione, anche in considerazione della gravità e della diffusione di un fenomeno che vede le donne vittime non sufficientemente tutelate e gli uomini maltrattanti bisognosi di rieducazione. Potrei anche chiudere qui il mio intervento, se non fosse che questa è una seduta pubblica, quindi proseguirò rivolgendomi - per suo tramite, signor Presidente - al pubblico presente e agli italiani che hanno ancora voglia di seguire questi lavori parlamentari, a cui resta l'utilità della denuncia dell'esautoramento della propria funzione e del fatto che, giorno dopo giorno, decreto dopo decreto, fiducia dopo fiducia, questo Governo sta portando l'Italia verso il baratro della stagnazione e in vista di una recessione. I dati infatti non premiano la marcia solitaria di questo Governo. A inizio dicembre Istat ha rilevato il crollo dei principali indicatori economici: il PIL precipita, gli investimenti crollano, la produzione industriale continua a diminuire, prosegue il *trend* in calo dei redditi e la spesa delle famiglie si contrae. Mi viene da sorridere all'idea che, mentre chi osa parlare del concetto di decrescita felice viene irriso, questo Governo ci stia portando veramente verso una decrescita, per di più priva del connotato della felicità. Eh sì, perché la decrescita, per essere felice, deve essere volontaria e portare a una riduzione selettiva e controllata della produzione economica e dei consumi, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Oggi invece assistiamo a una infelice decrescita, frutto di scelte sbagliate. In questa manovra infatti non c'è nulla a favore della crescita, ma ci sono tagli di spesa e rincari. Per far quadrare i conti, si riduce la spesa per servizi e non si fanno investimenti produttivi. Ma dove vogliamo andare così? Spiegateci qual è la strategia. In un momento di crisi, leggendo la crisi come la combinazione del pericolo da scongiurare con l'opportunità da cogliere, si dovrebbe analizzare il contesto, valutare le opzioni e investire in modo da creare valore aggiunto. È ciò che ha fatto il Governo Conte con il superbonus, che ora questa maggioranza demonizza come il male assoluto, senza invece considerare che la spinta che ha dato è riuscita a rimettere in moto un'economia immobilizzata e annientata dalla pandemia. Una misura virtuosa, che investe per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico, inducendo un risparmio nella spesa per energia e contestualmente promuovendo l'autoproduzione di energia nella direzione dell'indipendenza energetica, il tutto passando attraverso la creazione di posti di lavoro e alimentando l'indotto del settore edilizio. creando crescita, andando ad innalzare il PIL e, in ultima analisi, consentendo l'aumento della spesa. Ma perché sto a ripetere qualcosa che è di dominio pubblico, qualcosa che anche questa stessa maggioranza, che ora lo combatte, invece ha sostenuto e promosso in campagna elettorale? Pare che persino i membri di questo Governo se ne siano avvalsi: Salvini, Zangrillo, Sangiuliano, Calderoli, Valditara e la stessa Meloni. Ora dite che è una truffa ai danni dello Stato? Che i cittadini si sono rifatti la casa a spese dello Stato? Bene, allora, se questa è una truffa, siate coerenti e restituite il maltolto. Lo stop repentino e non modulato al superbonus e le modifiche apportate al suo sistema di finanziamento hanno messo in crisi famiglie e imprese; si salveranno le prime solo se salveremo le seconde. Ma cosa sta facendo questa legge di bilancio per le imprese? Nulla. Mi chiedo se questo Governo sappia cosa significa fare impresa: significa avviare un'iniziativa, è la combinazione della capacità di analisi di un mercato accompagnata dall'intuizione di un possibile sviluppo di un'idea produttiva di benefici. Come può uno Stato aiutare le imprese? Allo stesso modo: analisi, intuizione e sviluppo, precostituendo le condizioni per agevolare l'operato delle imprese. Ma occorre avere una visione, analizzare profondamente il contesto e le prospettive, trovare le risorse e poi avere il coraggio di investirle. Tutto ciò è assente. Le risorse non si sono volute trovare laddove si sarebbero potute trovare: mi riferisco alla tassazione degli extra profitti bancari, assicurativi e farmaceutici e mi riferisco al taglio dei sussidi ambientalmente dannosi. Tutto ciò perché manca fondamentalmente la visione, manca l'individuazione della direzione dove andare. Le imprese sanno bene dove sta andando il mondo, ma non trovano il sostegno di un Governo ancorato ad antichi meccanismi, che non sa riconoscere come obsoleti. L'Italia rischia di isolarsi e di restare indietro, perché la logica del mercato è implacabile: o arrivi tra i primi o ti restano le briciole, e poi devi rincorrere la concorrenza a caro prezzo. La sintesi perfetta di questo concetto me l'ha offerta un collega di maggioranza in una pausa dei lavori. Diceva, citando un detto popolare: dove c'è sparagno non c'è guadagno (dove «sparagno» sta per risparmio). La spavalderia di questo Governo si sgonfia davanti all'evidenza. In Europa viaggiamo con il freno a mano tirato e la nostra politica interna ne risente. Per esempio, sulla proposta di regolamento degli imballaggi l'Italia di recente è stato l'unico Stato membro a votare contro, sulla base della considerazione che quel regolamento quel regolamento punta al riuso, mentre la nostra industria è forte nel riciclo e noi vogliamo difenderla, senza capire che impresa significa dinamismo, che impresa significa saper leggere il mercato e non perdere il treno. Manca la fiducia nella capacità delle imprese italiane di sapersi riconvertire al momento giusto, affiancando magari una produzione all'altra. Come si può pensare di far quadrare i conti senza porre solide basi per garantire alle nostre imprese di essere presenti sui nuovi mercati e di essere competitive? Anche sul tema della transizione ecologica e delle risorse energetiche, questo Governo dimostra di avere poche idee e confuse e di non saper cogliere l'opportunità del PNRR per cui ha combattuto il MoVimento 5 Stelle con il presidente Conte. Come raggiungeremo gli obiettivi della riduzione al 2030 delle emissioni di gas serra al 55 per cento? Come raggiungeremo il *target* della percentuale di aumento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica? Quando elimineremo i SAD? Dove sono gli sforzi verso la decarbonizzazione? Dove sono gli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici? Vogliamo parlare poi della scatola vuota del piano Mattei, ieri prontamente ribattezzata dal collega Lorefice "piano piano Mattei"? *(Applausi)*. Non è dato sapere quale sia la strategia, se il sostegno all'Africa sarà dato in tema di progetti per energie rinnovabili, oppure di sfruttamento di quelle fossili: non mi pare una questione marginale. Poi, non vogliamo mettere la ciliegina su questa torta malriuscita? Parliamo Parliamo del Ponte sullo Stretto: visto che siamo in ristrettezze economiche, prendiamo 12 miliardi, che potrebbero tornare utili per garantire servizi essenziali, e buttiamoli in un'opera che nessuno vuole e che sicuramente non è né urgente, né indispensabile. Un'opera che vorrebbe collegare tra loro gli inadeguati sistemi viabilistici di Calabria e Sicilia; un'opera tanto inutile quanto ambientalmente dannosa, finanziata anche definanziando lo sviluppo delle due Regioni *(Applausi)*. Due Regioni che avrebbero invece bisogno di investire per potenziare la viabilità interna, i servizi di trasporto pubblici, creando una rete adeguata, sicura ed efficiente. Sembra uno scherzo e allora scherzo per scherzo, propongo di fare un bel ponte a rotelle,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo in Aula per discutere del provvedimento più importante dell'anno parlamentare, quello che forse incide di più sulla vita degli italiani e delle italiane. Potrei soffermarmi sull'aumento dell'IVA sui prodotti per l'infanzia, sulla diminuzione del *bonus* psicologico dai 25 milioni dell'anno scorso ai soli 8 per il 2024; potrei parlare del pasticcio sui fondi per il Ponte sullo Stretto, sottratti dai fondi di coesione per il Sud, ma in questo mio intervento, Presidente, vorrei concentrarmi esclusivamente sulle mancate politiche per gli italiani all'estero in questo disegno di legge di bilancio e in generale da parte di questo Governo. Vi ricordate lo *slogan* «prima gli italiani»? questo *slogan* ha dominato la propaganda della maggioranza negli ultimi anni, ma evidentemente il ragionamento non vale per gli italiani residenti fuori dai confini nazionali, che secondo gli ultimissimi dati hanno raggiunto i sette milioni di iscritti AIRE, senza contare i moltissimi cittadini che ancora non sono iscritti al registro e chiaramente i milioni di oriundi italiani nel mondo. Lo dico a lei, Presidente, e per suo tramite alla maggioranza: io sono stata eletta nella ripartizione Nord e Centro America e ho l'onore di rappresentare circa 500.000 concittadini, senza contare centinaia di migliaia di italiani che sono in attesa di riacquistare la cittadinanza. Come saprà, infatti, i termini per il riacquisto sono chiusi da ormai Ogni anno il numero degli iscritti AIRE aumenta - come sottolineato poc'anzi - e così aumenta anche il numero di concittadini che necessitano di servizi efficienti. Immaginate se ogni anno una città come Agrigento, Benevento o Carrara sparisse del tutto dal territorio italiano per riapparire in varie parti del mondo. Per ben oltre un decennio, il blocco del *turnover* del Ministero degli affari esteri ha comportato una drastica riduzione del personale di ruolo nelle nostre sedi consolari, ma questo Governo continua ad ignorare l'importanza dei servizi consolari, non riconosce che fornire servizi adeguati degni di una Nazione occidentale e ricca, qual è l'Italia, ha un diretto impatto sulla reputazione del nostro Paese nel mondo e rappresenta, o almeno dovrebbe rappresentare, il nostro biglietto da visita all'estero. E con l'aumento ogni anno dei connazionali che decidono di trasferire la residenza all'estero, si dovrebbe avere un piano mirato e lungimirante proiettato verso il futuro. futuro. Questo Governo sceglie invece di guardare dall'altra parte ed ignorare le criticità della nostra rete diplomatico-consolare che prima o poi toccano tutti gli italiani nel mondo. Ebbene, proprio per questo, per cercare di colmare questa lacuna, ho presentato un emendamento che chiedeva di bandire uno o più concorsi pubblici o di far scorrere le graduatorie vigenti, con il fine di aumentare ulteriori 100 unità di personale per il 2023 e 420 per il 2024. Un emendamento che però è stato bocciato. Sempre a sostegno della nostra rete consolare ho presentato un emendamento per aumentare la dotazione del rimborso spese ai nostri consoli onorari nel mondo, i quali forniscono un servizio prezioso al MAECI, praticamente praticamente a costo zero. Tale emendamento chiedeva un aumento di appena 400.000 euro per tutti i 344 consoli onorari nel mondo; una cifra sostanzialmente irrisoria. Ma anche questo mi è stato negato. Passiamo al turismo di ritorno o turismo delle radici, un tema che chi conosce il mio impegno parlamentare sa che mi sta molto a cuore e per il quale mi sono spesa. Come sicuramente saprete, il MAECI ha intitolato il 2024 anno delle radici italiane; un grande evento di richiamo per gli immigrati italiani nel mondo e per i loro discendenti. Alla luce di questo importante appuntamento per i connazionali italiani all'estero, ma soprattutto per il settore turistico di questo Paese, ho presentato due emendamenti importanti. Presidente, nella legge di bilancio di tre anni fa, cioè del 2021, all'apice di un periodo così difficile dal punto di vista economico e sanitario per il nostro Paese, sono riuscita a fare approvare un emendamento che per gli ultimi tre anni ha consentito l'ingresso gratuito agli iscritti ai musei pubblici e ai parchi archeologici statali. In questi tre anni, nonostante il Covid, sono milioni i concittadini nel mondo ad aver usufruito di questo mio emendamento, come ha dichiarato tempo fa anche l'ex ministro del turismo Garavaglia, esponente importante di questa maggioranza. In un momento così difficile per il nostro Paese questi nostri concittadini hanno contribuito alla ripresa economica dell'Italia, con introiti che hanno superato di gran lunga il costo associato alla scontistica prevista, poiché hanno pernottato, mangiato e comprato italiano durante il loro soggiorno. *(Applausi)*. Peccato però che questo Governo non abbia voluto riconoscere il valore di questo emendamento e che non abbia voluto rinnovarlo. Peccato che questo Governo si riempia la bocca di orgoglio italiano nel mondo senza mai dimostrarlo nei fatti. *Idem* per quanto riguarda la modesta scontistica proposta dalla sottoscritta per incentivare il turismo ferroviario sul territorio nazionale, sempre per gli iscritti AIRE. Per i nostri Comites, organismi di rappresentanza di base presenti in tutto il mondo, dove vi è una comunità italiana importante a sostegno soprattutto dei nuovi arrivati, che forniscono un servizio fondamentale,

Cari colleghi della maggioranza, le mancate politiche a favore degli italiani nel mondo in questa legge di bilancio e da parte di questo Governo, in generale, non sono un torto che si fa agli emigrati, ma rappresentano invece un grande torto all'Italia. Gli italiani del mondo non hanno bisogno di mancette, ma di politiche lungimiranti che sappiano valorizzare questo grande bacino con enorme potenziale, soprattutto economico, e che sono tra l'altro i più grandi promotori del *made in Italy* e contribuiscono alla ricchezza di questo paese. Peccato, l'ennesima opportunità sprecata.

se questa manovra di bilancio fosse un libro e dovessi dare un titolo a questo libro... *(Brusio).* Scusi, Presidente, non riesco a parlare. Come dicevo, se questa manovra di bilancio fosse un libro e dovessi dare un titolo a questo libro, non avrei assolutamente dubbi. Il titolo perfetto sarebbe: «Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde» perché quello che è scritto, nero su bianco, in questa manovra di bilancio è esattamente tutto il contrario di quello che Giorgia Meloni e gli esponenti delle varie forze di maggioranza propagandavano di essere pronti a fare. Giorgia Meloni-dottor Jekyll in campagna elettorale tuonava contro l'Europa, contro i soffocanti lacci del Patto di stabilità. Ebbene, Giorgia Meloni-mister Hyde in questa manovra applica esattamente questi lacci senza batter ciglio, tagliando la spesa pubblica, riesumando politiche di austerità vecchie di vent'anni e riproponendo feticci tanto cari ai falchi d'Europa. Mi sto riferendo all'avanzo primario. Un esempio evidente e lampante sono i tagli alla sanità pubblica, con oltre tre decimali di punti in meno di spesa sanitaria sul PIL, cioè 6 miliardi in meno per combattere le liste d'attesa; 6 miliardi in meno per incrementare il personale; 6 miliardi in meno per adeguare gli stipendi di medici ed infermieri, semmai drenando fondi verso il settore privato. Insomma, il diritto di tutti alla sanità in Italia diventa il privilegio di pochi. Che dire poi di Salvini-dottor Jekyll, che in campagna elettorale giurava e spergiurava che avrebbe cancellato la riforma Fornero? Salvini-mister Hyde, per mano del suo ministro Giorgetti, non solo riesce a mettere nero su bianco l'elogio della cosiddetta legge Fornero nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, ma addirittura riesce a rendere più difficile andare in pensione: di fatto, viene cancellata opzione donna e l'APE sociale *(Applausi)*, e vengono tagliate le pensioni di 700.000 dipendenti pubblici, tra medici e insegnanti. Ne abbiamo anche per Forza Italia-dottor Jekyll, che in campagna elettorale difendeva a spada tratta il bene supremo delle famiglie italiane. Sì, sto parlando della casa, la stessa casa che Forza Italia-mister Hyde in questa manovra riesce a tartassare aumentando sensibilmente le tasse. Come? Attraverso l'aumento delle ritenute sui bonifici parlanti; attraverso l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi; attraverso la cancellazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa degli *under* 36. Il vero capolavoro, Presidente, è quello che tutte le forze di maggioranza riescono a fare - attenzione - non in campagna elettorale, ma proprio mentre sono al Governo. Sapete a cosa mi riferisco? Mi riferisco a quando il dottor Jekyll si presenta agli italiani e annuncia una norma sulla tassazione degli extraprofitti bancari. Leggo testualmente le parole di Giorgia Meloni-dottor Jekyll, che dichiara: «In seguito alla discutibile decisione della BCE di alzare i tassi d'interesse che porta all'aumento del costo del denaro si è creata una distorsione: le banche hanno aumentato gli interessi sui mutui ma non hanno alzato quelli sui depositi, a favore dei risparmiatori». Che dire, sarebbe stato perfetto ed effettivamente sarebbero entrati circa due miliardi che potevano essere destinati agli italiani che fanno fatica a sostenere il peso delle rate dei mutui, che sono cresciute fino al 75 per cento in più. E invece no, perché si ripresenta in Aula mister Hyde, che riscrive abilmente la norma, e ciao ciao due miliardi da extraprofitti bancari. Come se non bastasse, al danno mister Hyde aggiunge anche la beffa. I due miliardi spariti dalla norma sulla tassazione degli extra profitti bancari riappaiono in questa manovra di bilancio. Sapete come? Come due miliardi di nuove tasse sui cittadini italiani; come ad esempio le tasse sulla casa, di cui ho parlato prima, o come le tasse sui beni dell'infanzia e sui beni per le donne. Sì, perché anche qui Giorgia Meloni, dottor Jekyll, a parole sostiene la maternità, la famiglia, le donne e poi, appena diventa mister Hyde, di fatto raddoppia l'IVA sul latte in polvere, sui pannolini, sui prodotti per l'igiene intima della donna. Cancella Opzione donna: esemplare, devo Signor Presidente, c'è di più. Questa è una manovra totalmente inadeguata a rispondere alle vere emergenze dei cittadini, perché, non solo non c'è nulla contro il caro mutui, ma non c'è niente di significativo neanche contro il caro vita. Infatti, la tanto propagandata rimodulazione, ripresentazione, riconferma del taglio del cuneo fiscale, con un beneficio, di fatto, già totalmente eroso dall'inflazione, non metterà altri soldi in tasca agli italiani, che purtroppo, a fine gennaio, si ritroveranno con la stessa identica busta paga di fine dicembre. È una manovra pavida, perché volutamente non va a tassare la montagna di extra profitti dei colossi dell'energia. Però, gli italiani, durante quest'anno, hanno versato nelle casse dello Stato oltre sei miliardi di tasse semplicemente andando a fare il pieno di benzina alla propria auto. Ed è una manovra senza visione, perché non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla che contrasti la tendenza, ormai purtroppo consolidata per tutto il 2023, che vede un crollo verticale della produzione industriale. E non lo dico io. Lo certifica Istat, che a dicembre ha fotografato il nono calo consecutivo. Se questa manovra di bilancio fosse solo un libro, frutto della fervida fantasia di uno scrittore, il lettore potrebbe giungere alla fine della lettura, chiudere il libro e dimenticarlo sullo scaffale più alto della libreria a prendere polvere. Purtroppo per gli italiani, però, questa è la legge di bilancio, che parte dagli appunti di Giorgia e finisce col condannare l'Italia alla stagnazione, col rendere l'Italia fanalino di coda, tra le ultime, tra i Paesi membri dell'Europa, per crescita nel 2024. Saremo dietro Paesi come la Spagna, Paesi come la Grecia. Il tutto non muovendo un dito, non solo per i più deboli, ma dimenticando totalmente anche il ceto medio, perché non c'è un solo straccio di provvedimento a sostegno di quel 63 per cento di famiglie italiane che - come ha certificato Eurostat - non arriva alla fine del mese. A meno che, per suo tramite, signor Presidente, il Governo e voi della maggioranza non siate realmente convinti che bastino provvedimenti come il carrello tricolore. il carrello tricolore. In questo caso, non c'è dubbio che sareste bravissimi a scrivere libri di barzellette. La realtà, purtroppo, è che avete deciso di scrivere una manovra lacrime e sangue

Presidente, questo provvedimento traccia una linea di demarcazione molto chiara, netta, tra fantasia e realtà: la fantasia della vostra perenne campagna elettorale e la realtà, quasi come un contrappasso, per voi che urlavate «la pacchia è finita», senza sospettare che poi potevate essere voi stessi i primi destinatari di quella profetica affermazione. Per uno strano gioco del destino, magari architettato dai tantissimi poteri forti a voi avversi e dei quali continuate a lamentarvi in continuazione, questa legge si chiama legge di bilancio - lasciatemelo dire - il bilancio di questi mesi del Governo Meloni è chiaramente e totalmente a saldo negativo. Partiamo dalle misure adottate nel settore delle infrastrutture. Qualcuno al Governo ha deciso di sfilare la felpina e di indossare un bel costumino da supereroe che sblocca i cantieri. Scopriamo, però, che il fondo che sblocca i cantieri - dovete sapere che esiste un fondo *ad hoc*, definito, appunto, fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, quindi un fondo che sblocca i cantieri, sul quale mi aspettavo venissero

Poco prima avevo letto che l'ultima ripartizione di questo fondo a 3.000 enti locali che ne avevano fatto richiesta è risultata nel mese di luglio del 2023 pari a circa 460 milioni di euro: quindi esce 460 e voi ci rimettete 300. Fatemi capire: andiamo a coprire solo un mesetto a partire da gennaio? Ho proposto, allora, di incrementare questa dotazione, portandola a un miliardo di euro, una proposta decisamente trasversale: non è un fondo gestito da una parte politica oppure da un'altra, ma è un fondo utilizzato dai Comuni e dagli enti locali che, a causa dell'aumento dei prezzi, prezzi, fanno richiesta d'accesso. Troveranno poco per la distribuzione. Qualcuno dovrebbe dire al ministro Salvini che si può togliere il costumino e si può rimettere la felpetta, perché a quanto pare la parte del supereroe dello sblocca cantieri non gli riesce Allo stesso modo, avete bocciato un'altra mia proposta che, sempre per andare incontro alle esigenze degli enti locali, prevedeva l'istituzione di un fondo *ad hoc* presso il Ministero delle infrastrutture per la realizzazione, progettazione e manutenzione di strade, ponti e viadotti

un ponte che pochi conoscono, ma che collega la bassa Regione Abruzzo con la parte alta del Molise; un ponte chiuso che ha necessità di essere ripristinato per il collegamento dei cittadini di quelle aree. So che la Provincia di competenza ha chiesto al Governo la quota di 16 milioni di euro per il ripristino di questo fondo. Leggo il subemendamento molto interessante che stanzia 15,5 euro. chiesto un correttivo, ma il correttivo non passa, perché riformulate l'emendamento e invece che i 16 milioni chiesti dalla Provincia di competenza, ovvero dalla Provincia di Isernia, ne stanziate 9. 9. Comunque meglio di prima. Immaginatevi il presidente della Provincia di Isernia se si fosse visto arrivare un bonifico di 15,5 euro. *(Applausi)*. Con nove milioni ne fate la metà, di questo ponte, ma meglio di 15 euro. Va bene, andiamo avanti. Ho chiesto poi la stabilizzazione del *bonus* trasporti, in modo da renderlo strutturale e non una semplice misura *spot.* Ma niente da fare, alla faccia di studenti e pendolari che - loro no - non possono chiedere di scendere dove vogliono quando il treno è in ritardo. *Bonus* trasporti *spot.* Stendo poi un velo pietoso sul potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, progetto da voi definanziato ed escluso dal PNRR. escluso dal PNRR. Il Presidente di Regione e i suoi sodali continuano a dire che l'opera resta prioritaria e verrà fatta, ma continuate a non dire con quali soldi. Allora mi sono permessa di avanzare una proposta, visto che si tratta della mia Regione: diamo un impulso, facciamo vedere che comunque comunque quest'opera è veramente importante e stanziamo qualcosa. Ho proposto di buttare in legge di bilancio 100 milioni, in maniera da riprendere quei lotti, che pare ormai vi siate dimenticati. Niente, anche questa proposta bocciata. Niente di niente. Sul superbonus si è detto

il *bonus* campagna elettorale nelle mani di Salvini, togliete risorse fondamentali a Sicilia e Calabria, ma levatemi una curiosità: avete detto ad Elon Musk che, mentre lui sviluppa un treno *hyperloop* a levitazione magnetica, in gran parte della Sicilia e della Calabria i treni vanno a gasolio e che, se vanno su un binario unico? *(Applausi)*. Immagino che non glielo abbiate detto. Così come non avrete detto al patron di Tesla anche della vostra avversione per l'elettrico o che per voi lui è il colpevole di un reato universale, visto che ha fatto ricorso alla maternità surrogata.

Signori, c'è ben poco di cui gioire e di cui vantarsi. Come *slogan* della vostra recente *convention* avete scelto il seguente titolo «Bentornato orgoglio italiano». fantastico. Avete quasi distrutto il Paese nel 2011. Siete sempre gli stessi e adesso siete tornati per completare l'opera. Peraltro orgoglio di che cosa? Di come avete abbandonato le famiglie in difficoltà; dello stipendio dignitoso che avete negato a quattro milioni di italiani, affossando il salario minimo; delle tasse sui prodotti per l'infanzia; dei soldi torti a Calabria e Sicilia per i capricci di un fannullone?

cedo due Mattarella per mezzo Putin; proteggeremo e tuteleremo il superbonus - sì, certo - faremo il presidenzialismo - questo c'era scritto nel programma di Fratelli d'Italia, mentre ora parliamo di premierato - 1.000 euro con un *click* per tutti, via le accise sulla benzina; via le commissioni bancomat; via la legge Fornero; tasseremo gli extraprofitti delle banche perché è una misura sacrosanta. Ecco, colleghi della maggioranza, le carte restano e sono tantissime e in continua battitura, come ad esempio il vostro fantastico ordine del giorno che avete approvato in Commissione che distribuisce soldi a pioggia su interventi localistici. Questo me lo aspetto da un bilancio regionale, non da un bilancio dello Stato.

i lavoratori sfruttati e sottopagati hanno il sacrosanto diritto di trascorrere un fine settimana su un prato bello verde, facendo buche.

all'ombra di un pianto greco mal recitato e fatto di continui e ripetitivi lamenti che poco hanno di sovranista e certamente non celano la vostra inadeguatezza. Allora, Allora, signori del Governo, fate luce voi stessi su queste tenebre. Fate luce sulle vostre bugie, sulle nomine ai parenti, sugli appartamenti, sui quadri, sull'uso distorto e a scopo politico di informazioni riservate.

presidente Meloni, che recentemente ha attaccato il MoVimento 5 Stelle dicendo che c'è chi ha creduto al partito fondato da un comico. Bene: non fate le vittime, gli *underdog*. Anche questa volta, vi assicuro che anche voi fate tanto ridere.

un film, un romanzetto di fantasia, ma io passerò a un documentario. Poco più di un anno fa, quando dovevamo ancora votare per le elezioni politiche - hanno portato evidentemente alla vittoria del centrodestra e alla formazione di questo Governo - ricordo molto, molto bene e non senza un sorriso come alcune forze e alcuni esponenti della sinistra dipingevano il centrodestra: arrivano i fascisti; manderanno a gambe all'aria il Paese; non hanno credibilità internazionale; lo *spread* li manderà a casa. Ecco, cari colleghi dell'opposizione, a essere mandati a casa siete stati voi e non dallo *spread*, ma dagli italiani, che sono molto più forti e molto più decisivi dei vostri spauracchi, ma non solo. Tutto quello che avevate previsto con assoluta certezza, come se solo voi aveste il dono del verbo, non si è affatto realizzato. Lo *spread* è più basso rispetto a quello di quando c'eravate voi, i mercati ci danno fiducia e le agenzie di *rating*, che qualcuno invocava e sperava ci declassassero, ci hanno addirittura promosso. Anche a livello internazionale, si è cercato di buttarci addosso del fango: qualcuno è andato a Bruxelles a parlare di pericolo di autoritarismo in Italia; altri parlavano con cancellerie internazionali per dipingerci come inaffidabili e novelli dittatori. Ora, non bisogna essere luminari di scienze politiche laureati ad Harvard per comprendere che a dipingere in questo modo le forze democratiche che stavano per vincere le elezioni si faceva il nostro male, che poi ci potrebbe anche stare - ci siamo abituati - ma si faceva il male del Paese, il male dell'Italia. Dipingere un'Italia isolata a livello internazionale, quando proprio questo Governo ha rilanciato il ruolo del nostro Paese a livello globale, mettendo al centro della nostra politica estera l'interesse nazionale e un nuovo *focus* sul Mediterraneo per difendere gli interessi strategici italiani in un'area per noi fondamentale, è stato un buco nell'acqua. Predire poi l'arrivo degli Unni in campo economico, e poi trovarsi invece la concretezza di un ministro dell'economia come Giancarlo Giorgetti, che con pragmatismo, serietà e competenza ha ridato credibilità al Paese, è stato un altro buco nell'acqua. grazie a questa grande concretezza, caratteristica inudibile della Lega, e a quella di tutto il Governo, abbiamo presentato la manovra in esame, che è seria, credibile e responsabile,

due guerre, una alle porte dell'Europa e un'altra in Medio Oriente, tra l'altro, con effetti geopolitici e geoeconomici impattanti. Voglio ricordare ad esempio cosa sta succedendo nel Mar Rosso: anche lì, c'è non solo il problema della sicurezza, ma anche quello economico delle rotte commerciali e navali. Le decisioni di questa manovra sono state adottate con la consapevolezza delle dinamiche globali, assicurando che l'Italia sia posizionata in modo competitivo sulla scena internazionale. Questa legge di bilancio riflette una visione strategica che mira a promuovere la crescita economica, a sostenere l'occupazione e a migliorare la vita dei cittadini. Le scelte del bilancio sono state guidate da una solida comprensione delle sfide economiche e sociali, evidenziando la determinazione nell'indirizzare le risorse verso quelli che riteniamo settori chiave.

è diventato una sciagura, una catastrofe per le casse pubbliche, a cui, proprio grazie a questo Governo, si è detto basta. Potrei elencarvi diversi provvedimenti contenuti nella manovra, ma vorrei soffermarmi su alcuni in particolare, esempio su quelli che vogliono contrastare la denatalità, come la decontribuzione delle madri lavoratrici, il bonus per gli asili nido, il potenziamento del congedo parentale, gli incentivi per le nuove assunzioni di mamme disoccupate, l'incremento dei *fringe benefit*, altri che pensano alle nuove generazioni, come il bonus mutuo giovani, le risorse per la formazione e la scuola. Grazie anche alla Lega - e questo vi dimenticate di dirlo, cari amici dell'opposizione - c'è la proroga della riduzione dell'IVA sui pellet; e poi ancora, grazie all'impegno del nostro ministro Matteo Salvini, investimenti massicci per nuove infrastrutture strategiche in tutta Italia, da Nord a Sud, includendo e non escludendo nessuno. Permettetemi poi, essendo componente della Commissione esteri e difesa, di evidenziare un provvedimento per il quale ringrazio la collega Pucciarelli, già componente del Governo, a cui ci tengo particolarmente: l'incremento dei fondi per la sicurezza, per dare agli uomini e alle donne della difesa stipendi più alti, *welfare* rafforzato e assicurazioni *ad hoc*. *ad hoc*. In tema di rischio idrogeologico - questo non è stato detto - sono state stanziate risorse grazie tra l'altro a un mio emendamento, che poi è stato trasformato in un ordine del giorno recepito dal Governo, per potenziare le risorse destinate alle autorità di bacino, che evidentemente hanno un ruolo strategico e fondamentale nel preservare le aree a rischio alluvionale. insomma, serio e responsabile, che tutela le fasce più deboli e che, allo stesso tempo, dà sicurezza ai *partner* internazionali. Presidente e colleghi dell'opposizione, di aver svolto bene in questa fase le nostre prerogative parlamentari. Lo abbiamo fatto attraverso continue interlocuzioni con i Ministeri, al fine di migliorare ulteriormente una legge di bilancio che vuole solamente dare risposte importanti e di prospettiva per il bene degli italiani e del Paese. Permettetemi in conclusione di ringraziare tutto il Gruppo Lega in Commissione bilancio, iniziando dalla relatrice Elena Testor e dal capogruppo Claudio Borghi, e tutti i colleghi della maggioranza, *in primis* i correlatori Guido Liris e Claudio Damiani, i sottosegretari Federico Freni, Sandra Savino e Lucia Albano, con i quali abbiamo condiviso un lungo e importante percorso, per terminare positivamente un lavoro fatto con la testa e con la responsabilità di chi vuole effettivamente il bene del nostro Paese.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, a proposito di Governo, vorrei solo far rilevare che il ministro Giorgetti non è mai venuto in quest'Aula e neanche in Commissione bilancio. Forse si è reso conto del disastro che ha fatto e non ci vuol mettere la faccia. Questo risulta, però, semplicemente in una mancanza di rispetto delle istituzioni. Quindi invito lei, Presidente, a chiedere al ministro Giorgetti di venire qua domani - è ancora in tempo - perché mi sembra opportuno che questa Aula abbia riconosciuta la sua dignità. In questa legge di bilancio si è fatto un gran parlare delle risorse destinate alla sanità, purtroppo facendo una gran confusione e alimentando aspettative che non corrispondono alla realtà. È infatti ormai assodato che nessuna risorsa è stata stanziata per incrementare il Fondo sanitario nazionale, cioè la quota riservata alle Regioni con cui si finanziano le prestazioni sanitarie, gli ospedali, la medicina territoriale. Corrisponde invece al vero che siano stati stanziati 3 miliardi, che però andranno a incrementare il fabbisogno sanitario, che è un'altra cosa rispetto al Fondo. Lo dico in quest'Aula, perché pochi giorni fa, proprio qui, persino la *premier* Meloni ci ha detto che i tre miliardi destinati sarebbero andati a incrementare il Fondo sanitario nazionale. Le cose sono due: o la *Premier* non sa la differenza tra fabbisogno e fondo sanitario, oppure mente sapendo di mentire. A tal proposito, non saprei quale tra le due sia la peggiore. A proposito delle risorse stanziate nell'ambito del fabbisogno, bisogna specificare che il disegno di legge di bilancio prevede esattamente come siano spese: dei 3 miliardi circa, 2,4 saranno utilizzati per il rinnovo dei contratti per medici e operatori sanitari per il triennio 2021-2024. È una scelta questa sacrosanta - ci mancherebbe altro - ma, mentre si aumentano gli stipendi, il Governo ha scelto di tagliare le risorse per le loro pensioni, ottenendo il risultato che moltissimi medici e operatori sanitari stanno fuggendo in pensione, almeno chi può. Poi, con uno dei tanti emendamenti, il Governo ha provato a correggere, ma la toppa è pure peggio del buco. Infatti, l'articolo 33 è rimasto lì e l'emendamento prevede solo alcune limitazioni della sua efficacia. Quindi, la misura resta e prevede una deroga per i sanitari e basta; una disparità rispetto a tutti gli altri soggetti interessati proprio da quell'articolo 33, che è lì ed è rimasto intonso. Insomma, la toppa è peggio del buco. Ma veniamo ai residui, circa 500 milioni, previsti: l'articolo 42 prevede un aumento della tariffa oraria degli operatori sanitari per l'abbattimento delle liste d'attesa, il cui costo è 280 milioni. Mi chiedo e vi chiedo: lo avete mai visto o incontrato un operatore sanitario? Pensate davvero che le liste di attesa si possano abbattere facendo lavorare ancor di più i sanitari? I medici e gli infermieri sono allo stremo delle forze. *(Applausi)*. È anche per questo che fuggono dal Servizio sanitario nazionale. Ad ogni modo, anche questa misura - come vedete - non va ad incrementare il Fondo sanitario. Poi c'è l'articolo 44, che prevede un aumento dell'aggio per le farmacie aperte al pubblico per la distribuzione dei farmaci. Io son pure farmacista. Figuriamoci! È certamente una misura condivisibile: costo 53 milioni. Ma anche questa misura non non va ad aumentare la spesa per le prestazioni sanitarie. Poi c'è l'articolo 46, che prevede l'aggiornamento del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni dal privato, costa 124 milioni. Questa misura rivela qual è il progetto della destra: finanziare e far correre il Servizio sanitario privato, così chi ha i soldi si cura e salta la fila e chi i soldi non li ha deve attendere mesi e mesi per ricevere una prestazione, oppure deve rinunciare a curarsi. Poi ci sono i 50 milioni per l'aggiornamento dei Peccato che il precedente Governo ne aveva stanziati 200 per il 2024. Quindi, anche qui, si è previsto un taglio. Ecco qua, il conto è presto fatto: neanche un euro andrà alle Regioni per incrementare le prestazioni. Spiegatelo alla presidente Meloni: neanche un euro andrà al Fondo sanitario nazionale. Se poi si considera che l'articolo 43 innalza il tetto della spesa farmaceutica, possiamo dire che le risorse per le Regioni sono tagliate per effetto di una riduzione del *payback* farmaceutico. Quindi, il punto non è che le risorse sono insufficienti per effetto dell'aumento del costo delle materie prime, dei costi energetici e dell'inflazione. Il punto è che si tagliano le risorse alle Regioni, che saranno costrette a tagliare le prestazioni, o a finanziarle con risorse proprie, magari aumentando le tasse. Come avete potuto ascoltare, non ho parlato del fatto che con queste risorse la spesa sanitaria scenderà nel 2024 al 6,4 per cento rispetto al PIL. Non vi piace parlare di percentuali rispetto al PIL, mentre è proprio attraverso questo parametro che si misura in tutti i Paesi OCSE lo stato di salute dei servizi sanitari pubblici. Si è stabilito che sotto il 6,6 per cento del PIL nessun servizio pubblico può resistere e può farcela. Voglio qui ricordare che il precedente Governo era arrivato al 7,4 per cento rispetto al PIL. Noi avevamo un'idea diversa per questa manovra. Abbiamo detto che sarebbero serviti quattro miliardi in più da destinare principalmente all'abbattimento del tetto di spesa per l'assunzione degli operatori sanitari, perché solo così si abbattono le liste d'attesa; e Mancano 25.000 medici e 70.000 infermieri; cifre assurde che non possono essere ignorate. E poi avremmo posto la necessaria attenzione alla riorganizzazione della medicina del territorio. A tal proposito voglio ricordare che già l'hanno passato il ministro Schillaci aveva promesso una fantomatica riorganizzazione, ma fino ad oggi niente si è visto e niente si è fatto. Avremmo poi fatto un'altra cosa; avremmo destinato risorse per la salute mentale, portandole

Le preoccupazioni che ho espresso e che denotano la gravità della situazione sono le stesse che hanno espresso medici e infermieri che aderiscono ad Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Nursing up, che qualche giorno fa hanno scioperato. Si è trattato di uno sciopero straordinario che ha raggiunto l'85 per cento di adesioni. Se leggiamo attentamente la manovra, non si possono non comprendere profondamente le ragioni dello sciopero. Noi rischiamo di assistere al crollo del Servizio sanitario nazionale, così come lo abbiamo conosciuto: gratuito e universale. Con questo intervento ho cercato di ripristinare la verità sui conti che il Governo vuole nascondere, che si trasformerà in un *boomerang*, anche se saremo tutti noi italiani

abbiamo pensato una manovra per imbavagliare il popolo italiano, per tartassare i cittadini, per dare di più a chi è più ricco. Siamo cioè delle persone che abbiamo preso i voti

In realtà quello che non viene detto è che noi ci troviamo a discutere e approvare una legge di bilancio in un quadro internazionale ed economico particolarmente complesso, ben due conflitti in questo momento che sconvolgono il mondo alle nostre porte. A ciò si sta aggiungendo l'emergenza della sicurezza dei trasporti marittimi nel Mar Rosso, dove stiamo inviando anche delle nostre forze militari e non perché amiamo il conflitto, semplicemente perché amiamo tutelare i nostri interessi nazionali *(Applausi)*. E, per questo, servono forze di difesa adeguate, che dobbiamo sostenere, pur mantenendoci ben al di sotto del 2 per

scelte, che - a nostro avviso - sono quelle della giustizia sociale e della crescita. Solo che noi le abbiamo orientate in maniera differente rispetto al passato. Ci siamo preoccupati dei redditi medio-bassi e quindi abbiamo finanziato con ben 10 miliardi il taglio del cuneo contributivo. Sarà una manovra in proroga - come vi è stato detto prima

avendo chiaro il costo del debito che in questo momento siamo costretti a sostenere, fatta sapendo che scellerata del superbonus, per come è stato pensato e congegnato, ci appesantisce di ben 20 miliardi di euro l'anno per i prossimi anni.

una manovra che punta alla giustizia sociale e alla crescita, e lo fa nel quadro anche di altre misure. Penso alla delega fiscale che stiamo attuando con i decreti che il Governo sta ponendo in essere in queste settimane. Penso alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

rimesso in ordine gli obiettivi che si voleva dare e che sta facendo delle opere pubbliche sostenibili e che hanno una loro logica; non era semplicemente un elenco della spesa messo purchessia.

Io ci abito e faccio politica in Sicilia, ma non ricordo queste forze politiche che hanno promesso di mantenere il reddito di cittadinanza. Vi ricordo che Fratelli d'Italia, a costo di perdere punti di consenso, ha promesso di abolire il reddito di cittadinanza e l'ha fatto. L'ha fatto non per andare contro i poveri, ma semplicemente perché crede che la dignità dell'uomo, del cittadino, non è vivere di assistenzialismo, ma vivere della dignità del lavoro. Ricordo le nostre misure di programma, tra cui favorire

per garantire una sanità che ci tuteli in qualsiasi passaggio. Tuttavia, per scelte non nostre ma del passato, non le abbiamo. Nonostante con coraggio, le risorse disponibili, oltre che per il taglio del cuneo contributivo, le abbiamo messe per incrementare il Fondo per il fabbisogno sanitario nazionale. Quindi abbiamo scelto di continuare a puntare sulla sanità, tanto è vero che in valore assoluto - qualcosa conterà - questo è il maggiore stanziamento degli ultimi anni. I tagli sono stati fatti negli anni dai "Governi dei migliori", dei tecnici, del centrosinistra, non da noi. Noi comunque abbiamo aumentato le risorse del fabbisogno sanitario. Questi Certo, abbiamo utilizzato anche risorse per lo scorrimento delle liste d'attesa, anche ricorrendo al privato convenzionato; vivaddio, le liste d'attesa esistono adesso, non quando riusciremo ad assumere le persone che dobbiamo assumere. Quindi abbiamo un'emergenza immediata di smaltire quello che si è accumulato anche durante l'emergenza Covid. Naturalmente, abbiamo la visione prospettica di una sanità pubblica e universalistica che deve funzionare, che ha anche un ramo di sanità convenzionata. Tale ramo non va demonizzato, va semplicemente messo nei limiti che la Costituzione e la politica gli devono dare.

di proposte di buon senso sono state accolte, con le risorse disponibili. Che io ricordi, nel passato questo non accadeva. C'era semplicemente un muro contro l'unica opposizione esistente, per un certo periodo, nella vita repubblicana, che era quella di Fratelli d'Italia. Una opposizione che, per la sua coerenza, ha ottenuto consensi e che quindi può procedere per realizzare il suo programma, anche con questa manovra di bilancio.

si capiscono le linee di azione di questo Governo, quali sono stati i suoi obiettivi, quali sono state le sue priorità. Sono sicura che il giudizio che se ne ricaverà non sarà un giudizio tanto positivo, anzi, sarà un giudizio in cui si metterà in evidenza come questo Governo, nel fare i conti, nel considerare le risorse disponibili, quali le possibili entrate e quale il tasso di indebitamento col quale fare i conti, alla fine ha abbozzato una manovra miope, discriminatoria, che penalizza sempre le stesse fasce, che sono le famiglie, i lavoratori, le donne e che, per l'ennesima volta, dopo più di un anno di Governo, non prevede nulla per il Sud lo lascia nuovamente a bocca asciutta; dopo le sue trionfalistiche dichiarazioni di sostegno verso il meridione, alla prova dei fatti concreta e pratica (e la legge di bilancio è la prova dei fatti per qualsiasi Governo) queste risorse non ci sono. Io condivido tutti gli interventi che mi hanno preceduto da parte delle forze di opposizione, perché in ognuno di essi è stato trattato ed approfondito un argomento: dalle varie misure che sono mancate, al sostegno che non si è verificato, a quelle che sono state le fasce discriminate. Quindi, focalizzo il mio intervento su due punti. Uno è relativo alle misure a sostegno della donna e l'altro è relativo alla sanità e al Sud. Sono due interventi, due *focus*, che devo fare. Signor Presidente, io ero convinta che il primo Governo della storia della Repubblica italiana con un Presidente del Consiglio donna sarebbe stato un Governo che si sarebbe caratterizzato per delle misure a sostegno della donna, della donna intesa come persona, della donna intesa come lavoratrice, come imprenditrice e anche come madre. Invece, questo Governo, non soltanto non si caratterizza per nessuna di queste misure, ma addirittura continua ad adottare misure improntate a una retorica sulla natalità che è davvero odiosa e insopportabile. Come se le donne meritassero tutela solo nel momento in cui sono madri. *(Applausi)*. Ma non basta neanche essere madri. Attenzione: bisogna essere madri con almeno più di un figlio, perché se ne hai solo uno

vale per il *bonus* asili: la donna ne usufruisce soltanto se ha più di un figlio. Allo stesso modo, le aziende che assumeranno una donna nel 2024 potranno beneficiare della decontribuzione, a condizione che questa lavoratrice abbia più di un figlio.

Altrettanto discriminatorio, spalmando questa discriminazione sulle fasce di reddito più basse, è l'aver eliminato l'esenzione dell'aliquota IVA sui prodotti per l'igiene personale per le donne e per gli alimenti per l'infanzia. Ancor più brutta e ancor meno sostenibile è la motivazione adottata, quando il Governo dice di averle eliminate perché tanto l'aumento del costo di questi prodotti avrebbe comunque neutralizzato l'esenzione. Ma come?

Così come, signora Presidente, la misura sicuramente più coraggiosa che ha varato questo Governo nella legge di bilancio non è appannaggio del Governo, ma la si deve alle forze delle opposizioni, alle quali va il mio ringraziamento come donna e come avvocato. *(Applausi)*. Mi riferisco al finanziamento di 40 milioni di euro che tutte le forze di opposizione, decidendo di lavorare in modo corale collaborativo, hanno deciso di destinare alle donne vittime di violenza. È stato sicuramente un grande esempio di buona politica, che però è venuto dall'opposizione, non dalla maggioranza, mi dispiace. *(Applausi)*. Il fondo parlamentare - diciamolo, i fatti vanno ricapitolati - era di 100 milioni a disposizione delle opposizioni, ma il Governo lo ha arraffato,

nessuno ha nulla da ridire, ma l'avrebbe potuto e dovuto fare con le sue risorse, non prendendo quelle destinate alle opposizioni. Con questi 40 milioni, responsabilmente le forze dell'opposizione

della Commissione bilancio, la mia collega, senatrice Paita, per essersi battuta fino all'alba per difendere questa misura *(Applausi)* e tengo a chiarire che non c'è una investitura, non c'è stata una federazione delle forze dell'opposizione in capo alla senatrice Gelmini, perché anche su questo la verità storica va ricostruita.

che è miope e anche temporalmente limitata. Pensiamo, ad esempio, al cuneo fiscale, che viene tagliato, ma soltanto per il 2024. Le fasce Irpef vengono ridotte, ma soltanto per il 2024. Non vorrei fare mai il lavoro del commercialista, ma neanche quello del funzionario dell'Agenzia delle entrate che si troverà fra un anno a dover fare le verifiche sulle dichiarazioni dei redditi del 2024, perché si troverà a dover articolare dei controlli che hanno avuto una durata temporale di un anno, su una manovra fiscale di un anno, sulla dichiarazione dei redditi di un anno. È l'orizzonte più limitato possibile, meno dell'esercizio annuale non c'è nulla, e questo è davvero sintomatico e riflette una politica asfittica, che ha un orizzonte veramente brevissimo. E pensare che il Governo aveva detto che il bilancio dell'anno scorso era sostanzialmente imposto, c'era piccolissimo margine di manovra, perché se l'era ritrovato sostanzialmente già impostato, mentre quello dell'anno successivo sarebbe stato finalmente il bilancio espressione del Governo, salvo poi dire che anche questo non è il bilancio espressione del Governo e sarà quello dell'anno prossimo. Ve bene, noi buttiamo sempre il cuore oltre l'ostacolo e speriamo in tempi migliori, ma la speranza non è sufficiente per sostenere l'economia degli italiani e soprattutto per migliorare la loro qualità della vita, che non si attesta fra le migliori, soprattutto non si attesta fra i migliori il tasso di occupazione femminile. Per questo, signora Presidente, non basta dire che si varano misure come il superbonus o come la decontribuzione quando non si tiene conto del fatto che il divario dell'occupazione femminile rende l'Italia fanalino di coda in tutta l'Unione europea: l'Italia è il Paese dove l'occupazione femminile è ai livelli più bassi in assoluto.

è certamente ancor più aggravato. Abbiamo chiesto due misure al Governo, la prima delle quali era volta all'istituzione di un fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti dell'insularità per il personale sanitario. Si tratta di un fondo modesto, chiedevamo un investimento di cinque milioni di euro da destinare ai medici che accettano di prendere servizio nelle isole minori, al fine di incoraggiare e incentivare la loro presenza. Signora Presidente, fra ricordare la situazione dell'ospedale di Lipari, un ospedale ridottissimo, con pochissimo personale sanitario che però deve far fronte a un'utenza importante, quella di tutte le isole Eolie.

di un trasporto in elisoccorso, quando non si potenzia o non si danno i mezzi alle isole minori per avere la loro sanità. Questo emendamento non è stato accolto, però il Governo ha accolto l'ordine del giorno nel quale è stato trasformato e si è impegnato a destinare le risorse per creare questo fondo di sostegno all'insularità. Di questo lo ringrazio, però al contempo dico che noi vigileremo, perché l'impegno non deve restare lettera morta, non deve restare sulla carta, ma si deve trasformare in realtà. realtà. Signora Presidente, un altro ordine del giorno che avevo presentato riguarda il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Questa è una tematica che mi sta ancor più a cuore di quella delle isole minori; si tratta di un centro di eccellenza per il quale avevamo chiesto di dare una dotazione annua di due milioni di euro (non abbiamo chiesto somme impossibili). un segnale di attenzione e soprattutto di rispetto verso un centro che opera a beneficio di tutta la Sicilia, della Calabria, nonché delle popolazioni dell'Africa e del Nord Africa, facendo anche attività di formazione professionale. anche in questo caso il Governo ci ha detto che la misura non poteva trovare ingresso nella legge di bilancio, però ha accolto l'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento e si è impegnato ad assicurare le risorse necessarie per garantire la piena tutela del diritto fondamentale alla salute, secondo i criteri di efficacia, efficienza e prossimità.

cercherà nuovamente di chiudere questo reparto vitale ed efficientissimo in nome di una politica sanitaria di riduzione degli sprechi, io potrò dire (e tutti i parlamentari lo potranno dire con me) che il Governo Meloni lo ha riconosciuto formalmente come un centro sanitario indispensabile e di eccellenza, la cui esistenza e operatività costituisce attuazione del diritto fondamentale alla salute, declinato in conformità ai principi di efficacia, efficienza e prossimità.

sul mondo della casa. Intanto ricordo alcuni inserimenti nel bilancio: per esempio, abbiamo rifinanziato il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, dotandolo di 282 milioni, e abbiamo prorogato la possibilità di usufruire della garanzia massima all'80 per cento. Sul regime fiscale delle locazioni brevi, per chi opta per la cedolare secca, grazie a Forza Italia il primo alloggio messo in locazione avrà una tassazione del 21 per cento invece che al 26 per cento. Di fatto, quindi, abbiamo aiutato tutti i piccoli proprietari immobiliari che mettono in affitto l'alloggio per periodi brevi. però non abbiamo lavorato e non stiamo lavorando solo al bilancio, perché sono *in itinere* importanti provvedimenti: ricordo il nuovo piano casa per l'Italia di cui si sta occupando il Governo, tramite il ministro Salvini; qui in Senato in 8a Commissione ci stiamo occupando della normativa sulla rigenerazione urbana, di cui sono relatore, che sarà il vero futuro per le nostre città, in una nuova *partnership* tra pubblico e privato, per rigenerare gli immobili insieme alle periferie e ai centri urbani, al fine di rendere le città più a misura d'uomo e più ecosostenibili. Come vedete, quindi, il centrodestra e Forza Italia stanno stanno facendo molto per il settore della casa: manca solo un nodo, legato a un aspetto del superbonus al 110 per cento. Intanto, voglio sgomberare il campo dal fatto che pensiamo cento sia stato una misura folle, voluta principalmente dai 5 Stelle, che ha fatto tanti danni al bilancio dello Stato - abbiamo sentito il ministro Giorgetti più volte fornirci i numeri

quindi era un disastro annunciato. In più, si sono cambiate le regole decine di volte (mi sembra 26 in totale), creando confusione nella cittadinanza, ma anche nei tecnici. Ha permesso inoltre molte truffe, soprattutto all'inizio.

dei cittadini onesti, delle imprese oneste, dei fornitori onesti e dei professionisti onesti, cioè di tutte quelle persone che si sono fidate delle leggi dello Stato e che quindi giustamente hanno iniziato i lavori usufruendo

io spero che, prima della fine dell'anno, riusciamo in qualche modo, magari con un provvedimento apposta o nel milleproroghe, a prevenire il problema, che è sempre meglio, anziché doverlo curare poi l'anno prossimo.

la *Premier* aveva annunciato una novità assoluta nella storia italiana: la manovra di bilancio sarà approvata entro il 15 dicembre. siamo al 21 dicembre, qui in Aula, ancora in fase di discussione generale. Domani, 22 dicembre, voteremo *in extremis* in prima lettura la manovra finanziaria. Ma gli annunci della Presidente non si fermano: è una manovra senza emendamenti della maggioranza. Beh, l'abbiamo sentito che poi gli emendamenti della maggioranza ci sono stati, li abbiamo visti e sentiti in quest'Aula dagli interventi dei colleghi, ma li abbiamo visti ancora di più chiamo in causa i colleghi della Commissione bilancio - con gli emendamenti del relatore, con gli emendamenti del Governo e con tutte le contrattazioni che abbiamo visto, perché le contraddizioni interne alla maggioranza si sono viste anche nella valutazione degli emendamenti del relatore e del Governo. Altro annuncio, sempre a fine novembre: la manovra è espansiva. Questa è stata proprio l'affermazione più assurda, dopo aver letto la manovra. Però mi sono messa nei panni dei colleghi della maggioranza, perché in effetti siamo di fronte alla seconda manovra di questo Governo di destra, un Governo politico, come più volte ci ricordate. Anzi, quando ne avete occasione, ce lo ricordate sempre: finalmente un Governo politico, finalmente un Governo con un'investitura popolare, finalmente un Governo di legislatura. Dunque con quale coraggio vi potevate presentare davanti agli italiani, con l'atto politico per eccellenza di un Governo, un atto che determina le scelte finanziarie di spesa pubblica, che incide sulle politiche economiche, sociali e fiscali, che influenza direttamente la vita dei cittadini e l'andamento dell'economia nazionale? Come potevate dire che invece la manovra è austera, fatta di tagli e di nuove tasse? Una manovra con poche risorse, recuperate tra l'altro in *deficit*, non espansiva (l'abbiamo già detto), senza risorse per investimenti, quindi senza crescita, che addirittura presenta dei tagli, come ho detto poco fa, e che immette nuove tasse. Per quanto riguarda i tagli, mi riferisco al non rifinanziamento di fondi importanti, come quelli per la ricerca, per la cura e per la sanità. L'abbiamo visto, abbiamo fatto alcune discussioni in Commissione bilancio e per fortuna che ci sono stati alcuni emendamenti portati portati avanti dall'opposizione. Parlo anche di nuove tasse, in particolar modo dell'aumento dell'IVA sui prodotti per l'igiene femminile e per l'infanzia (i pannolini, il latte, i seggiolini). Si bloccano le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli *under* 36, si blocca la detrazione IVA al 50 per cento per l'acquisto di case con classi energetiche superiori. Una manovra che mette la pietra tombale sulla crescita e sulla qualità della vita nel nostro Paese. Zero misure per il lavoro e no al salario minimo. Almeno avete gettato la maschera della sedicente destra sociale, che ha preferito introdurre nuove tasse e fare cassa sui poveri e sulle pensioni con il falso pretesto della coperta corta. Perché dico falso? Perché la coperta l'avete resa voi corta. È corta perché il Governo Meloni non ha avuto il coraggio neanche di sfiorare i miliardi di extra profitti dei grandi settori economici, che hanno conseguito utili record grazie a circostanze eccezionali quali la pandemia, la crisi energetica e la guerra. La coperta è corta perché questo Governo ha scelto di stare con le banche e non con i poveri cittadini che percepiscono salari da fame. Ha scelto di stare con le case farmaceutiche e non con le piccole e medie imprese. Ha scelto di stare con l'industria bellica, anziché con chi non riesce a entrare, o rientrare nel mercato del lavoro, ma questa è la tipica politica di un Governo di destra. di destra. Qualche giorno fa, proprio a quell'evento che la Meloni dipinge come politico, ma che si traduce in una semplice ovazione al pensiero del *leader* allargato ai suoi familiari, dopo tutti gli annunci fatti a fine novembre, la *Premier* afferma candidamente che siamo di fronte a una manovra di bilancio molto seria e realistica; attenzione, non austera, come dicono le opposizioni. Beh, sarà che io sono dell'opposizione e l'ho letta austera questa manovra, però - ne dobbiamo dare atto *Premier* afferma che non è espansiva: almeno questo lo afferma. Continua la *Premier* affermando che è molto fiera del risultato raggiunto, anche grazie ai sacrifici e ai tagli alla spesa che tutti noi abbiamo fatto a Palazzo

In linea con le misure scioccanti che la destra sempre si inventa, avete messo in finanziaria 9,3 miliardi per l'ormai leggendario Ponte; meno male che la coperta era corta, meno male che non c'erano soldi *(Applausi)*, però i soldi per il Ponte li abbiamo trovati, svuotando e ipotecando un intero Ministero delle infrastrutture (basta leggere le tabelle allegate). Tra l'altro, lo si fa con un progetto, il cui *iter* per arrivare al progetto definitivo non è stato concluso, come affermato dal sottosegretario Freni in Commissione bilancio. Ora, è arrivato il momento di fare un po' di chiarezza, soprattutto ai siciliani e ai calabresi che avranno - su questo non ho alcun dubbio - un'inutile mostruosità al modico prezzo della rinuncia di 1,6 miliardi di investimenti in infrastrutture. Mi riferisco allo scippo del Fondo sviluppo e coesione, avvenuto con la benedizione in Consiglio dei ministri dell'ex presidente della Regione Musumeci. Sembrava meno d'accordo l'attuale Presidente della Regione siciliana, ma pare che abbia cambiato idea. Comunque dovrà spiegare ai siciliani che devono continuare a viaggiare su reti ferroviarie con percorrenze imbarazzanti, strade buone nemmeno per i muli, strade

un'opera che non è detto che costerà 11,6 miliardi (9,3 miliardi più 2 miliardi e qualcosa del Fondo di sviluppo e coesione), proprio perché il progetto definitivo non c'è ancora e secondo me, visto che sono siciliana, potrebbe avere lo stesso destino di tante autostrade siciliane che sono ancora incompiute, come la Siracusa-Gela che aspettiamo *(Applausi)* e la prima pietra fu messa nel 1970. Poi, parliamo dei vari siparietti sul calo demografico. Il Presidente del Consiglio attua bene tutti gli schemi classici della distrazione di massa, impiega il suo tempo a parlare di Ferragni o in inutili battibecchi a distanza, senza contraddittorio. Tutto, purché non si parli di questa manovra: una manovra senza emendamenti, ma con gli emendamenti, senza marchette, ma con le marchette; espansiva, ma profondamente recessiva; senza nessuna traccia di investimenti su scuola, sanità, infrastrutture vere, gestione del territorio, giustizia, imprese; questa nuova Madonna dei miracoli che con la sola presenza fa aumentare l'occupazione, fa calare il prezzo della benzina, dei generi alimentari, fugge dal contraddittorio che darebbe il corretto significato delle statistiche sull'occupazione

come tutto passa nella vita. Molti atti saranno insignificanti, ma alcuni continueranno a dispiegare i loro effetti molto tempo dopo la loro approvazione. La valutazione dei fatti e degli atti di questo Governo lascia emergere tutto l'atteggiamento predatorio che la maggioranza ha verso il Sud, me lo lasci dire. Ogni investimento viene pagato con i fondi per il Sud, la riserva di caccia del ministro Fitto e di questo fondo delle meraviglie del Governo Meloni. Il Ponte e i progetti non finanziati con il PNRR fanno ricorso al fondo delle meraviglie, alla riserva di caccia di Fitto. Domani il Sud pagherà di tasca propria l'attuazione dell'autonomia differenziata, oltre alle sue devastanti conseguenze. la realtà storica emergente è chiara e se a questo si lega anche il progetto di reintroduzione delle gabbie salariali, allora la realtà storica emerge senza possibilità di occultamento. Il Mezzogiorno d'Italia deve continuare la sua decadenza demografica, economica, sociale e culturale. Il suo destino è quello di essere fornitore di manodopera a basso prezzo e questo questo non potrà cambiare, così come si devasta il territorio con opere faraoniche che servono solo a fare arricchire chi le costruisce. Arretratezza e mancanza di infrastrutture non è per voi un *gap* da combattere e colmare, ma una precisa necessità del capitalismo decadente italiano che state rappresentando per continuare a sommare profitti sulla vita dei siciliani, dei sardi, dei calabresi, dei campani.

in Commissione bilancio, nonostante le molte ore che abbiamo passato insieme ed il favore

Damiani ha parlato di adeguamento ai problemi che ci sono. C'è questa doppia linea che io non riesco a capire. La cosa mi turba, da cittadino prima ancora che da legislatore, perché se non si comprende che questa legge di bilancio è un fallimento nel metodo e nel merito (spiegherò perché tra un minuto), allora gli errori che sono stati compiuti sono destinati a riprodursi. Questa è la cosa che a me oggi preoccupa di più proprio nel passaggio tra l'entusiasmo e la consapevolezza. Per sintetizzare questa cosa che non capisco da parte della maggioranza, mi è venuta in mente una frase di Churchill che forse voi avete interpretato come una ammissione, ma era una battuta. Churchill diceva che il successo è il passaggio da un fallimento ad un altro con entusiasmo. Ecco, mi pare che questo possa definire la coesistenza dell'entusiasmo nel definire da parte della maggioranza successo quello che invece a me appare un fallimento, nel metodo e nel merito. Nel metodo noi abbiamo dimenticato che questa legge di bilancio conclude un anno straordinario di *record* nella fiducia, nella decretazione d'urgenza, dell'*omnibus*. Sembra che questo Governo debba scrivere a Palazzo Chigi qualcosa che somiglia a ciò che sta nell'oracolo di Apollo a Delfi. Lì c'è scritto «conosci te stesso», a Palazzo Chigi bisogna scrivere emenda te stesso. La capacità di questo Governo di produrre emendamenti a se stesso è una cosa storica; abbiamo il gusto della sorpresa.

agli emendamenti del Governo, che emendavano la legge proposta dal Governo medesimo, sono stati bocciati anche dalla maggioranza per poi sentir esprimere da parte dei relatori un parere conforme alla bocciatura del Governo dei propri subemendamenti agli emendamenti del Governo. Si potrebbe dire con una battuta una storia infinita, senonché è una storia un po' triste perché, anziché, come nel romanzo di Ende, contrastare il nulla, sembra generarlo. La questione che mi ha preoccupato è che a un certo punto abbiamo superato il *record*, quando abbiamo visto il ministro Ciriani domenica sera, arrivare alla riunione e dire: a proposito dell'ultimo decreto che abbiamo presentato un'ora fa, siamo detti "perché questa fretta?" E lo chiedete a noi? Chiedete a noi perché non presentarlo con calma? Perché non capire di cosa si sta parlando? Lì credo che abbia prevalso l'umano sentimento di stabilire un altro *record*, cioè proviamo a superare noi stessi, in questa rincorsa ad autoemendarsi, che non la materia specifica. Fuori dalle battute, parliamo di merito. Questa è una legge di bilancio che nel migliore dei casi ha questo numero: 0,2 - l'ha detto molto bene la collega Furlan prima - come moltiplicatore, nel primo anno di un Governo politico, come voi ripetete, post-pandemico. Questa è una sconfitta enorme: stiamo già vedendo gli effetti del rallentamento del progetto del PNRR. Non solo, ma quel PNRR si andrà a congestionare nella parte finale, con un enorme razionamento dal lato dell'offerta, per cui non riusciremo a fare quel tipo a fare quel tipo di investimenti in tempo. Abbiamo visto anche gli interventi sulla sanità. L'ha detto molto bene la collega Zambito e non mi ripeto. È evidente che qui non si tratta di giocare con i numeri, ma si tratta di giocare col fatto che dall'uscita dalla pandemia tutti i Paesi avanzati si stanno ristrutturando, e lì bisognava concentrare l'unico intervento. Invece il Governo ha voluto pensare a livello di propaganda, perché siamo in campagna elettorale, a seminare delle briciole per avere dei titoli; briciole che negli effetti non solo producono una crescita sostanzialmente inesistente: oggi la Banca d'Italia dice che sarà la metà di quello che c'è scritto. Quindi già sappiamo che nella prossima legge di bilancio, oltre a dover coprire eventualmente la misura del cuneo fiscale, che è soltanto provvisoria (un anno), quindi abbiamo già una copertura da fare,

un'azione economica di visione, di prospettiva su moltissime questioni. Ne cito alcune semplicemente per ricordarcele: oltre al PNRR, la questione del taglio di misure sulla crescita; la questione che riguarda l'ACE, cioè la parte di incentivo alle imprese che per ammissione

ma sappiamo che una serie di questioni sono rimaste fuori. Gli enti territoriali: tagli per 600 milioni. Sui fragili veramente grida vendetta il fatto che un tentativo di superare il momento della scadenza per andare al milleproroghe, che aveva una quota molto riservata, e l'emendamento presentato su questa materia dalle mie colleghe senatrici siano stati bloccati dal Governo, nel momento in cui purtroppo c'è di nuovo un rilancio della pandemia e del contagio. Questo grida vendetta perché nello stesso momento, nella stessa notte, nella stessa Commissione, abbiamo avuto un comma - mi pare il quinto quinto - di un emendamento che finanziava la Croce Rossa, e che in questo impulso di soccorso soccorreva anche il ministro Lollobrigida, autorizzando 2 milioni di assunzioni per la collaborazione diretta del Ministro. Abbiamo avuto un finanziamento a una che deve fare educazione finanziaria. Non sono riuscito a trovare il nome del comitato scientifico, perché non è scritto nel sito *web*, al quale è stato dato 1,2 miliardi. C'è una strada che sicuramente va fatta, a Vibo Valentia, ma non credo che quel tipo di costo, per quella strada, potesse essere una priorità rispetto a creare dei fondi, a sommare delle risorse, per rispondere a queste esigenze che riguardano la vita e il lavoro delle persone.

ma sono state anche cancellate le norme e gli emendamenti da noi proposti che la ripristinavano. Altre misure, che sono state già citate e che sono esemplificative, riguardano il Ponte è un caso straordinario: intanto, perché il Ponte non c'è, ma noi già ne parliamo. Peraltro, vi è un nuovo emendamento. Anche qui, per non farci mancare niente, il Governo ha presentato un secondo emendamento,

si è realizzato un balletto straordinario, che mi ricorda il film "Totò, Peppino e la malafemmina", quando Totò ruba a Peppino dei soldi, che deve a Peppino, glieli restituisce e poi li riprende indietro dicendo: a questo punto siamo a posto, abbiamo compensato tutti i crediti. In questo caso, la figura di Totò la fa il Presidente della Regione siciliana, che, nel giro di qualche giorno, ha sottratto 300 milioni di euro a ospedali, strade, infrastrutture, per un accordo politico che fa di questa opera, che dovrebbe essere europea, un'opera che invece sottrae risorse importanti. Questo nel momento in cui, attenzione, molte risorse del PNRR sono state cancellate dal PNRR per essere inserite nei fondi di sviluppo e coesione, sostenendo che così avremo più tempo per realizzarlo, quando quegli stessi fondi, poi, vengono dirottati nuovamente verso il ponte.

per un'alternativa. Dobbiamo organizzare dei *tour*, per fare vedere agli italiani il Ponte, per fare vedere le liste d'attesa che non ci sono più, per far vedere gli ospedali che funzionano, per far vedere come le famiglie staranno ancora meglio e spezzare questo racconto illusorio prima

ad un anno dalla costituzione del Governo Meloni, è forse il caso di dare qualche numero sullo sforzo profuso e inquadrare nella giusta cornice l'azione di politica economica del Governo. Chiaramente, gli interventi contro il caro energia e quelli per frenare gli effetti della corsa dell'inflazione sulle tasche di famiglie e imprese hanno assorbito buona parte delle risorse disponibili. Lo scenario economico globale ha certamente condizionato le scelte dell'Esecutivo, con il conflitto in corso da un anno e mezzo in Ucraina, arrivato dopo due anni e mezzo di pandemia di Covid-19, che ha innescato la crescita dei prezzi in tutto l'Occidente ed ha aperto le porte ad una politica monetaria aggressiva da parte delle banche centrali. Va ricordato che abbiamo registrato dieci rialzi dei tassi in quattordici mesi per la BCE. Una politica da falchi del rigore monetario al quale il nostro Governo, pur rispettando le scelte, non ha risparmiato appunti nella convinzione che la sola leva monetaria non sia sufficiente se non accompagnata da una spinta alla crescita. Nonostante la congiuntura difficilissima, fra tassi di interesse in netta salita e due conflitti, gli indicatori macro dell'ultimo anno hanno comunque mostrato una sostanziale tenuta dell'economia italiana, pur nel contesto di salari più bassi rispetto alla media europea. Le agenzie di *rating* non hanno declassato l'Italia, anzi l'agenzia Moody's ha migliorato l'*outlook* da negativo a stabile. I dati sull'occupazione sono particolarmente incoraggianti, abbiamo il più elevato tasso di occupazione che non si registrava da anni. Nonostante il contesto terribile, il Governo ha optato per una linea improntata giustamente alla prudenza al dialogo. Va ricordato che il Governo Meloni si è insediato due mesi dopo il picco del prezzo del gas al megawattora, 339 euro, e ha lavorato subito per tentare di sostenere i redditi medio-bassi e le imprese nel fronteggiare le bollette energetiche, divenute in alcuni casi astronomiche, dedicando due terzi delle risorse della prima manovra a questo obiettivo. Avevamo poi stanziato 1,2 miliardi per escludere dal versamento dell'IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché attività commerciali. Abbiamo iniziato a ridurre la quota dei contributi previdenziali, iniziativa potenziata con il decreto 1° maggio e prorogata con questa legge. Avevamo previsto una serie di sgravi contributivi, in particolare l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, la proroga per il 2022 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato apprendistato di primo livello e tantissime altre misure. Non c'è tempo di ricordare quella prima manovra di bilancio. Il senso, però, di rievocarla è perché vi è una linea chiara che stiamo andando a perseguire e che viene mantenuta per tutta la legislatura: ridurre la pressione fiscale e contributiva sui cittadini e le imprese *(Applausi)*, sostenere i redditi medi e bassi, ridurre la spesa corrente a favore degli investimenti. Per reperire le risorse necessarie senza eccedere nel debito pubblico, a differenza dei due Governi Conte, abbiamo dovuto optare anche per il contenimento della spesa. Mi riferisco, per esempio, alla revisione integrale del reddito di cittadinanza, sostituito da due distinte misure: quella destinata ai veri bisognosi e quella destinata agli occupabili in cerca di lavoro, da accompagnare con un sussidio ponte. Ci siamo quindi concentrati invece sul fisco per liberare risorse con l'approvazione di una legge delega pensata per semplificare il rapporto fra cittadini e imposte a cui sono seguiti a tempo di *record* i decreti attuativi, grazie all'incessante azione del vice ministro Leo. La riforma fiscale punta a ridurre gradualmente le aliquote Irpef, che diventeranno tre nella prospettiva di arrivare in futuro ad una sola e a omogeneizzare l'IVA per rendere l'imposta più aderente ai criteri dell'Unione europea. La scarsità di risorse a disposizione è un altro fattore che determina le scelte politiche economiche del Governo. Auspichiamo una riforma del Patto di stabilità che si sta componendo in queste ore, sul quale abbiamo alacremente lavorato anche come Commissione bilancio del Senato, che sia favorevole alla crescita e agli investimenti. Il rapporto debito-PIL è in discesa, gli interessi sul debito purtroppo, come dicevamo, sono in salita, il *deficit* è quasi dimezzato rispetto al Governo Draghi, ora al 4,3 per cento, e si va nella direzione di una razionalizzazione della spesa a livello centrale, con una riduzione di 7,8 miliardi del livello ministeriale. Stiamo sostenendo il denominatore del rapporto debito-PIL, incrementando quindi il prodotto. Due terzi delle risorse sono impiegate per sostenere i redditi medio-bassi, famiglie e servizio sanitario: dieci miliardi per ridurre il cuneo fiscale, quattro miliardi per ridurre le tasse di quegli scaglioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, un miliardo per la natalità. Possiamo fare di più? Su questo abbiamo fatto molto, ma dobbiamo fare ancora di più, vista l'emergenza in questo ambito così delicato. Abbiamo sulla salute, 280 milioni per gli straordinari di quei medici che tanto alacremente hanno operato e continuano e ad operare in questi tempi. Il principio che ricorderete del nostro programma per cui più assumi e meno paghi lo troviamo nella maxi deduzione per le imprese che assumono a tempo indeterminato. Vi è il fondo per le politiche agricole, gli investimenti per le grandi opere (475 milioni per le ferrovie, 350 per i porti, 125 per il Giubileo di Roma), 100 per 100 per contrastare il disagio abitativo, 1,8 miliardi per il Mezzogiorno, 350 milioni per la sicurezza, in particolare per rinnovare i mezzi in tale ambito e 113 per il trattamento economico. Come potete ben constatare, siamo stati e continueremo ad essere al lavoro per mantenere comunque, nonostante la difficoltà congiunturale economica dell'epoca che stiamo attraversando, un'intonazione espansiva, per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie,

ci aspettavamo una legge di bilancio autentica, perché lo scorso anno la prima manovra del Governo Meloni fu giustificata dicendo: non è la nostra legge di bilancio, in fondo siamo arrivati da

non è sorpreso che anche questa manovra sia così radicalmente diversa rispetto alle promesse elettorali, perché è proprio della natura dei sovranisti promettere determinate cose e, una volta andati al Governo, fare radicalmente qualcosa di diverso. Non ci spaventa, pertanto, che per fortuna i conti non sono stati sconquassati dalle promesse elettorali che avevate preannunciato ai ai cittadini, che avrebbero consentito di andare in pensione praticamente appena raggiunta la maggiore età, che avrebbero permesso di avere una quantità di soldi pubblici per ogni esigenza. Quello che non ci si aspettava è che fosse una manovra che aumentava le tasse, perché se c'era una caratteristica dei Governi del centrodestra di berlusconiana memoria era quella di promettere la riduzione delle

Ho pensato che fosse la sinistra più radicale, quella contraria alla cancellazione dell'IMU che fece inciampare al *premier* Renzi, ma nonostante questo l'IMU sulla prima casa fu cancellata.

contro di loro. Li accusate più o meno del fatto che le coppie non riescono ad avere un affitto in centro storico, dell'aumento dei prezzi, più o meno delle cavallette africane. Mi sembra un eccesso di attenzione nei confronti di realtà che consentono anche quel turismo che poi a parole ci piace sottolineare nei numeri. Non mi aspettavo che fosse cancellata l'Irpef agricola: ma come, il ministro Lollobrigida che dice che finalmente si fa una politica seria sull'agricoltura, toglie l'Irpef agricola alle aziende agricole? Perché? Ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B? Il famoso taglio del cuneo fiscale - che non è così storico, ve lo comunico: sarà quasi impercettibile sulle buste paga - non è per tutti: tutti: per esempio, non è per gli agricoltori. Mai l'agricoltura ha avuto così poche risorse: ha avuto molti tagli di nastri, quelli sì, e ha avuto molte leggi bandiera, ma poche risorse. Quello che manca assolutamente è la voce cultura: avete cancellato la 18app, perché avete detto che c'erano un sacco di truffe. Perfetto, allora mettetela sul resto. Non ci doveva essere la Carta giovani nazionale a sostituire la 18app? Non è pervenuta in un anno e ovviamente avete deciso di cancellare completamente questa voce, perché pensate che il disagio giovanile si combatta aumentando le pene, non aumentando la cultura. È la vostra cifra, ne siete convinti; noi invece continuiamo a dire che un euro di sicurezza dev'essere controbilanciato da un euro in cultura, ma è cosa di tanti Governi fa.

e abbiano una deduzione fiscale come avviene per il restauro: perché per il restauro sì e per la creazione di cultura no? Cos'è, non vi piace proprio la parola "cultura", vi sta sul

la conseguenza della guerra tra Ucraina e Russia se l'è dovuta sopportare ancora il Governo Draghi, tant'è vero che avevamo fatto alcune misure, che all'epoca erano state considerate insufficienti da chi

allora giunto il momento, visto che governate e, a vostro dire, lo farete per l'eternità, di chiedere scusa

dando e mettendo soldi nelle tasche degli italiani. Oggi infatti non solo non mettete soldi nelle tasche degli italiani, ma aumentate le tasse. che questo Paese stia vivendo un momento di grande difficoltà. C'è una congiuntura internazionale che non aiuta: la Germania e la Cina che non crescono economicamente non sono una buona notizia per l'Italia, che è un Paese esportatore. Non avete neanche cercato di raddrizzare la rotta, cercando di introdurre delle misure per aumentare la produzione economica interna e per aumentare i consumi interni. Delle due l'una: quando la bilancia internazionale non funziona, di solito si mettono in campo delle misure che servono ad aumentare la domanda interna. Invece questo non è accaduto. Non è accaduto su tutti i fronti, dal lavoro alla sanità, alle pensioni; non è accaduto in nessuna delle voci che sono nel sangue delle persone comuni. Avete aiutato qualcuno, qualche piccola nicchia vostra referente; ma questi non sono italiani, sono delle piccole nicchie. E allora chiudo veramente, Presidente, dicendo che, se ci sono tutte queste risorse sulla sanità, ditelo ai medici che continuano a protestare, perché forse non se ne sono accorti, come gli italiani non si sono accorti che arriveranno valangate di soldi nelle loro tasche. E lo si è visto da questo Natale, così arido e avido nei consumi.

così come è stato negli ultimi anni, dedicherò questo mio intervento per fare il punto sul fondo indennizzo risparmiatori, che ha interessato i risparmiatori truffati dalle banche, in particolare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e che è stato attivato - come molti colleghi ricorderanno - con la legge di bilancio del 2020. Inizierò con le note liete, Presidente. Sta procedendo a tambur battente l'erogazione della seconda rata dell'indennizzo da parte di Consap. I pagamenti sono davvero a buon punto e credo che per fine anno tutti gli aventi titolo riceveranno il dovuto, così come aveva ipotizzato qualche settimana fa Sestino Giacomoni, presidente Consap, cui va il mio sentito ringraziamento per il lavoro che sta facendo. Credo che sia giusto anche riconoscere il giusto merito del ministro Giorgetti, che, sempre su nostra istanza, su nostro pungolo e su nostro impulso, ha dato il via libera a questo importante aumento dell'indennizzo, che, come credo vada ricordato, per gli azionisti delle banche fallite passa dal 30 al 40 per cento del prezzo di acquisto, con un incremento davvero significativo del 33 La necessità di questo intervento l'avevo portata all'attenzione del Ministro esattamente un anno fa, nel corso del dibattito sulla legge di bilancio 2023; durante l'ultimo esercizio siamo riusciti ad ottenere questo aumento. È un'autentica boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà, in tempi complicati per l'economia. Peraltro questa seconda *tranche* di indennizzo era tutt'altro che scontata alla vigilia; richiedeva uno specifico intervento normativo ed è stata erogata in un periodo certamente tutt'altro che facile per il Paese e per la sua finanza pubblica, tra caro bollette, crisi energetica ed effetti negativi del superbonus 110. Molto bene, quindi: l'impegno che ci eravamo assunti nella scorsa campagna elettorale è stato adempiuto e di questo siamo particolarmente orgogliosi. È doveroso oggi darne atto con grande soddisfazione. Passiamo alle note meno liete e un po' critiche. Non è stato possibile in questa legge di bilancio ottenere dal Governo, come invece avremmo auspicato, il via libera al riesame, da parte di un organo terzo e imparziale, delle domande di indennizzo respinte in tutto o in parte. La questione l'avevo già portata all'attenzione del Governo mediante due ordini del giorno, che erano stati anche approvati: il primo in sede di decreto sulla competitività dei capitali e il secondo con il milleproroghe. In effetti, tutte le domande che sono state respinte non avevano una chiara ed analitica motivazione; peraltro la commissione tecnica non era tenuta a fornirla. Il termine per il ricorso al TAR contro i dinieghi nel frattempo è scaduto, a causa anche di qualche aspettativa generata nei risparmiatori e nelle loro associazioni per effetto di diversi tentativi di modifica in sede parlamentare della normativa primaria o di sanatoria di irregolarità delle domande. Ci sono ad esempio delle domande che contengono errori ai quali la rigidità del sistema non ha consentito di porre rimedio. C'è chi ha dichiarato in via telematica di avere 100 azioni; invece ne aveva mille, ma non è stato in grado di modificare in alcun modo questo dato, per cui l'indennizzo si è limitato alle 100 inizialmente indicate. Ci sono domande respinte solo per motivi formali. Avevo suggerito, con i citati ordini del giorno che sono stati accolti dal Governo, che queste domande potessero essere riesaminate da un soggetto o da un giudice terzo ed imparziale. Avevo individuato nell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) l'organo più adatto; questo perché l'ACF non necessita di formalità particolari, si pronuncia in tempi rapidi, è poco costoso e non richiede neanche l'assistenza obbligatoria di un legale. Questa rimane la proposta che sottopongo al Governo e ai tecnici del MEF, che però - ahimè - non l'hanno ancora accolta.

e approfitterò di questo mio intervento per iniziare un contraddittorio tecnico sul punto. Secondo tutti i dati acquisiti fino ad oggi, le domande respinte sono circa 4.800; le somme residue, secondo una mia stima, ammontano sicuramente a più di 100 milioni, stima che ho maturato alla luce dei seguenti dati che sottopongo all'attenzione del Governo. Al 31 dicembre 2022 sono stati erogati complessivamente indennizzi per 1,3 miliardi. La Consap, La Consap, a sua volta, ha detto che nel corso del corrente mese sono stati disposti i bonifici per ulteriori 275 milioni. Non sono invece disponibili, Presidente, i dati delle somme erogate dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest'anno, quando ha concluso i suoi lavori la Commissione tecnica. Diciamo che, verosimilmente, dello stanziamento iniziale di 1,55 miliardi residuano tra i 100 e i 200 milioni. Allora, quanto costa prevedere un riesame delle domande respinte? Faccio un conto approssimativo, sicuramente arrotondato per eccesso, perché ovviamente è impensabile che tutte le domande respinte siano ora accolte. L'indennizzo medio fino ad oggi erogato si può calcolare in 9.200 euro *pro capite*, dato che che si ottiene dividendo la somma di 1,3 miliardi fino ad oggi complessivamente erogata per le 140.000 posizioni accolte. Se poi moltiplichiamo i 9.200 euro per le 4.800 domande respinte, otteniamo complessivamente 44 milioni di euro, che, a mio giudizio, è una stima corretta del costo per il bilancio della misura che propongo. Siamo quindi molto al di sotto del residuo accantonato. Ripeto: 44 milioni è certamente un dato in eccesso, perché non è pensabile che tutte le domande respinte siano accolte in sede di riesame. Avrei piacere di confrontarmi con i tecnici del MEF su questi dati. Proseguirò pertanto, Presidente, nei prossimi mesi e in occasione dei provvedimenti economici del Governo che saranno portati all'attenzione di quest'Aula, nella mia opera di *moral suasion* e di iniziativa legislativa, perché credo che la chiusura ordinata della questione FIR necessiti di una verifica finale da parte di un soggetto terzo ed imparziale sulle decisioni della commissione tecnica. Come ho detto, io ho individuato nell'ACF questo organo, è stata una mia iniziativa, ma certamente sono disposto a confrontarmi con il Governo, coi tecnici del MEF e con chi si vorrà per individuare quello che può essere il giudice idoneo, il TAR o il giudice ordinario con una rimessione in termini, piuttosto che l'arbitrato che io ho

del Governo e della manovra che stiamo esaminando. Il Governo sta guidando con mano sicura in questi anni così complessi il nostro Paese e credo che il giudizio che possiamo dare sia assolutamente positivo. PRESIDENTE.

Presidente, questa credo sia la sesta manovra di bilancio a cui assisto da quando sono in Senato ed è senza dubbio la più anomala. Solo pochi giorni fa in quest'Aula avevo detto come questa maggioranza e questo Governo avesse ideato una novità assoluta, quella dell'austerità preventiva. aspettativa di che cosa? Ebbene, oggi questo mistero è stato definitivamente sciolto. Oggi è andato in onda lo *showdown* dell'Europa solidale, la fine di quell'Europa che con enormi sforzi diplomatici, di persuasione, di credibilità, era stata portata avanti dal presidente Conte nel 2020 e che aveva generato il Next generation EU. Cosa è successo? Io mi sento di fare un complimento, anche se non so bene a chi o a cosa, quindi dico genericamente all'ufficio comunicativo di Giorgia Meloni e della maggioranza. Sono riusciti infatti a coprire questo assoluto fallimento che l'Italia ha incassato in Europa dietro uno spettacolo pirotecnico che hanno mandato invece in onda alla Camera. Il no al MES Camera. Il no al MES ed esultano e cantano vittoria. Qui c'è un dovere morale di dare una spiegazione ai cittadini. Mi rendo conto che è una questione complessa e anche noiosa. Io l'ho sempre trovata francamente ed enormemente noiosa. Va però spiegata. Il no alla Camera al MES è un no alla sua modifica. Si tratta della modifica migliorativa per cui si era lavorato. Il MES rimane esattamente lì dove è. O forse non è corretto neanche dire questo. Che fine ha fatto in realtà il MES? Il MES è un arnese vecchio, come noi abbiamo sempre detto. È un arnese inutile ed antiquato, che era stato concepito agli inizi degli anni Duemila ed era stato approvato dal Governo Berlusconi, di cui Giorgia Meloni era Ministra. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Era stato approvato nel 2011 in un contesto socio-economico, internazionale e nazionale completamente diverso.

del pacco di Natale che questa maggioranza e il Governo Meloni stavano preparando per i cittadini italiani. Il pacco di stabilità e decrescita che è stato deciso dall'asse, ripristinato, franco-tedesco, da Berlino e da Parigi, dove Roma, Giorgetti e Meloni non hanno assolutamente toccato palla. Condizionalità che sono soltanto per il primo triennio leggermente più lievi per tutti i Paesi - guarda un po' - fino al 2027. Cosa succede nel 2027? Finisce il mandato di Macron e finisce il mandato di Scholz. Finisce però anche il mandato di Giorgia Meloni. Dopo quella data quindi l'Italia sarà lasciata come una barca in mezzo ai marosi di un'Europa tornata ad essere quella di prima della pandemia, tornata ad essere quella dei tecnocrati e quella assolutamente un minimo di flessibilità, strozza le economie delle Nazioni. Questo è il capolavoro che sono riusciti a fare e che per il momento stanno riuscendo a coprire con un armamentario comunicativo a cui io mi sento di fare i complimenti perché stanno continuando a mentire. Non solo Giorgia Meloni è venuta in quest'Aula

Non avete alcuna vergogna, alcuna remora. In questa legge di bilancio ho ascoltato tante parole. Non ho mai vissuto una legge di bilancio così anomala; prima per l'imposizione e il bavaglio messo alla maggioranza, poi, resisi conto che era una cosa insostenibile e che c'erano anche degli errori da emendare nel testo della legge di bilancio, si sono affrettati a mandare emendamenti dei relatori nottetempo per correggere ed inserire nuove cose, che non c'erano. Di certo, quello che c'è in questa legge di bilancio è un taglio di 21 miliardi alle pensioni dei dipendenti pubblici un taglio di 37 miliardi in dieci anni all'indicizzazione delle pensioni. Quindi si fa cassa sul sacrificio

Appena le banche hanno fatto un colpetto di tosse, immediatamente è sparito tutto e i grandi patrioti hanno alzato bandiera bianca, alla faccia invece del patriottismo e anche della dignità di questo Paese. Cos'altro c'è in questa legge di bilancio? C'è l'aumento delle tasse su pannolini, assorbenti, latte in polvere. Ho sentito dire in precedenza ai colleghi della maggioranza che si investono risorse sulla natalità. Ebbene, i fatti ancora una volta vi smentiscono, perché purtroppo vi riempite la bocca con il tema del contrasto alla denatalità, ma poi andate ad aumentare le tasse proprio sui prodotti che servono alle mamme, ai bambini e alle famiglie.

che contraddistingue questa maggioranza e in particolare Giorgia Meloni, che sta varando una legge - adesso arriverà anche qui in Senato, dopo essere stata approvata alla Camera - per cui viene dichiarato reato universale la gestazione per altri (Gpa), minacciando di mettere in galera cittadini e cittadine comuni italiane, ma invita con tutti gli onori sul palco di Atreju Elon Musk, che ha avuto ben due figli con la Gpa *(Applausi)*. Non è un criminale universale Elon Musk? Allora perché non l'avete ammanettato sul palco invece di applaudirlo? È veramente un'ipocrisia sconvolgente, perché come sempre siete forti con i deboli e deboli con i forti. Parlavo del Patto di stabilità, il "pacco di stabilità", che prevede che torni in auge l'austerità. Perché cantano vittoria? Perché sono riusciti ad inserire lo scorporo di alcune spese. Attenzione, questo è importante, perché inserire lo scorporo delle spese è un vantaggio per il Paese: significa che in quell'ambito possiamo permetterci di spendere senza pagare le penali sul debito che si accumula. Quali sono queste spese? Quelle per le armi, le spese per la difesa. E Giorgia Meloni ha detto: peccato, non siamo riusciti a inserire anche lo scorporo per il *green*. Ci crediamo molto che sia dispiaciuta, visto quanto sta puntando sulle energie rinnovabili e quanto sta puntando sul contrasto alla crisi climatica, che invece si ostinano a negare. Tutto questo per non parlare della sanità, che sarebbe

per cento in sanità. Ho bisogno solo di un altro minuto di tempo, perché noi delle opposizioni abbiamo concordemente deciso di devolvere quella piccola parte che spettava a noi, 40 milioni, a un tema unico che ritenevamo prioritario con le piccole risorse che avevamo, ossia il contrasto alla violenza contro le donne, e ne siamo orgogliosi. Ci siamo chiesti: ma cosa ha fatto invece la maggioranza dei suoi 60 milioni? Avranno trovato altri obiettivi nobili per cui spendere quelle risorse, piccole

Inizialmente era denominato "Littorio", in seguito "degli Sports" ed è stato usato dall'Unione sportiva fascista Barletta fino agli anni Settanta. È meraviglioso. Basta andare su Wikipedia per trovare queste informazioni. Prevede, ancora, 400.000 euro in favore del comune di Mura per la realizzazione di un immobile di destinazione turistico ricreativa: facciamo cioè gli hotel a spese dei contribuenti. Ma c'è di più: un contributo di 100.000 euro a favore dell'Associazione nazionale G*rano Salus*, con sede legale a Foggia. Andiamo a vedere che cos'è: c'è la mail personale di Saverio De Bonis, l'ex senatore Saverio De Bonis, passato a Forza Italia. Adesso mi spiego perché lo vedevo aggirarsi nei corridoi del Senato in procinto della legge di bilancio! È tutto vostro Saverio De Bonis! È tutto vostro, assolutamente! Chiudiamo questa onorevolissima carrellata con il campo da golf:

propinato in ogni ambito, in ogni settore: l'appropriazione del potere, l'arroganza. Tutto questo, tra l'altro, avviene senza bandi, senza trasparenza, senza gara. Alla faccia del merito, di cui Meloni ha tessuto l'elogio ad Atreju: il merito, non più gli amici degli amici! E questi chi sono, se non amici degli amici?

Signor Presidente, userò questi minuti per concentrare l'attenzione sul tema dell'agricoltura e degli enti locali, vista anche la presenza di un collega sindaco in Aula. Noi, in questa manovra, come anche in Commissione, nei quattordici mesi dall'insediamento del Governo, abbiamo notato che di provvedimenti in materia agricola non ne sono passati molti. Sono passate tutte misure - come correttamente ha detto qualche collega prima di me - istitutive di fondi: fondi emergenziali contro le malattie fitosanitarie, fondi emergenziale per l'emergenza idrica, fondo a sostegno del credito d'imposta sui carburanti. Tutte forme emergenziali, ma quello che noi notiamo è la carenza di una programmazione stabile in un settore in un settore che ha necessario bisogno di programmare, perché i suoi tempi di produzione, di trasformazione e di vendita sono molto lunghi e non ammettono estemporaneità. In questa legge di bilancio troviamo i fondi, ma senza contenuti. Mancano contenuti significativi per il rimboschimento delle aree interne, per il sostegno ai comparti agricoli in crisi, alle filiere, alla successione generazionale in agricoltura, in favore dell'imprenditoria femminile, al credito d'imposta per l'acquisto sul gasolio agricolo. Sono istituiti alcuni fondi, ma privi di un valore economico significativo per un settore che, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, attraversa il nostro intero Paese con criticità, con differenze, con bisogni completamente diversi. Dall'inizio della legislatura sosteniamo l'esigenza di un grande lavoro infrastrutturale in favore delle aziende agricole, per consentire la digitalizzazione. Spesso viene detto che sono state messe risorse in questa materia, ma purtroppo alle aziende agricole ancora la fibra non arriva. Il segnale per il collegamento e per la vendita *online* non arriva. Questo soprattutto accade in quelle aree interne che sono ancora più lontane dai mercati, dove la differenza la fa poter avere clienti in giro per il mondo e in giro per

hanno densità abitativa bassa, ma con gli stessi bisogni che hanno le popolazioni delle aree metropolitane e spesso chi in esse vive è un custode o un presidio per il territorio.

Purtroppo, quello che diceva anche la collega Maiorino mi fa pensare che in questo Paese non siamo tutti uguali, perché c'è chi si può permettere di veder scritto il nome del proprio Comune su una legge di bilancio per un campo sportivo o per un asilo. Ma i campi sportivi, le biblioteche e le associazioni sono in tutto il Paese e, se c'è una formula che dice "la legge è uguale per tutti", questo luogo dove siamo chiamati a legiferare dovrebbe essere il primo in cui si dà l'esempio che effettivamente la legge è uguale per tutti e non ci sono persone raccomandate in questo territorio. Tutti i sindaci, tutti gli amministratori, tutti i cittadini hanno diritto di poter avere le stesse opportunità, perché sono non per loro stessi, ma per i popoli che amministrano. Questo è un grave segno, e lo dico anche da sindaco di un Comune di questo Paese. molto preoccupato per il Patto di stabilità, perché so benissimo - come tanti altri colleghi - che cosa ha significato il Patto di stabilità quando era in vigore: contrazione degli investimenti in settori estremamente importanti come l'edilizia scolastica

ci sono centinaia di migliaia di ponti in questo Paese che hanno bisogno di avere la giusta manutenzione. *(Applausi)*. Credo che, prima di fare una grande opera, bisogna manutenere quelle esistenti, per cui non ci sono risorse sufficienti per garantire quella rete di viabilità sui nostri territori. Parlo anche da parlamentare del territorio. Abbiamo un ponte che è da dieci anni

Per quel ponte e per quella strada, però, non c'è dignità. Come non c'è dignità per quelle centinaia di migliaia di chilometri che percorrono la rete stradale nazionale. È necessario che, quando si varano le misure, lo si faccia tenendo conto anche dell'esistente e non dei sogni che vogliamo inseguire, perché molto spesso i sogni aiutano a vivere meglio, ma non risolvono i problemi. *(Applausi)*. In conclusione, auspico che ci sia attenzione anche rispetto ai trasferimenti agli enti locali, perché il fondo affitti è stato depotenziato; ci sono stati tagli ai trasporti, al fondo sociale per i deboli e, se avvenissero ulteriori tagli ai trasferimenti, i nostri enti locali non sarebbero più in grado di garantire i bisogni dei cittadini. E parlo di enti locali di destra, di sinistra, di centro e civici. Le fasce

ha delle difficoltà maggiori e delle sofferenze. E nessuno si vuol tirare indietro rispetto a delle condizioni anche straordinarie. Ma non possiamo lasciare soli gli amministratori, non possiamo lasciare soli i territori, non possiamo lasciare soli i cittadini e gli amministratori locali. Per questo credo che purtroppo oggi, per l'ennesima volta, dobbiamo constatare che siamo di fronte a un provvedimento che non ha una programmazione e non mette il giusto accento sul futuro strategico del nostro Paese, la nostra Italia. Signor Presidente, colleghe e colleghi, normalmente quando si arriva a discutere la legge di bilancio, ci si perde in mille rivoli e in mille dettagli, invece dobbiamo cercare di andare alla sostanza. La legge di bilancio contiene anche dei micro-interventi, ma poi quello che conta è la sostanza. Partiamo dal principio di fondo: può piacere o meno, ma questa è politica. Per la Lega, per questa maggioranza, prima di redistribuire un reddito, il reddito

e che è ulteriormente complicato da due fattori particolari e peculiari per l'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Il primo è il PNRR: è stato deciso così, sono decine e decine di miliardi

è dato dall'anomalia dei *bonus* edilizi, su cui oggettivamente abbiamo esagerato, con pesantissimi dubbi sugli effetti anche dal punto di vista dell'obiettivo dell'efficienza energetica. I recenti dati

diamogli il nome giusto - e, sempre tornando all'esempio di prima, è particolarmente antipatico se è andato a beneficio di una famiglia abbiente: che senso ha regalare la ristrutturazione a una famiglia abbiente?

Sul lavoro si è cercato di fare la cosa più giusta possibile: c'è l'inflazione, una tassa che colpisce soprattutto i redditi più bassi. Che cosa fa questo Governo di centrodestra?

Giusto, e andava fatto così. E va fatto così esattamente perché, nel momento in cui la Banca centrale europea, data l'inflazione, alza i tassi, cosa fa un Governo dotato di buon senso? Non può fare misure che aiutano tutti,

altrimenti si vanifica l'azione della BCE, che alza i tassi per abbassare l'inflazione. Ciò detto, ci auguriamo che adesso sia anche abbastanza veloce ad adeguare i tassi all'inflazione che cambia. Ma questo è un altro discorso.

di andare nella direzione di fare quello che abbiamo detto, secondo la filosofia di fondo, ossia creare posti di lavoro, lavoro e ricchezza tramite il lavoro. Non esiste la ricchezza per decreto. Questa è una fesseria e diciamocelo una volta per tutte.

La spesa centrale, fatta 100, è diventata 173. Visto quindi che si parlerà di autonomia, parliamone: siamo così certi che il centro sia così efficiente, nel momento in cui riesce a crescere da 100 a 173 e gli enti territoriali da 100 restano a 100? La risposta è no: il centro non è efficiente. Cosa fa allora - giustamente - il Governo? Dovendo tagliare la spesa, dove la taglia? Al centro:

collocate là dove servono e non per la pasta lavamani, tanto per capirci. Bene, chiudo. Questa è la filosofia di fondo di questa legge di bilancio. Può piacere o no, ma per la Lega funziona così: si premia chi lavora e chi produce ricchezza. E così si fa anche con la delega fiscale, dove si va a premiare chi lavora e chi produce ricchezza. Noi siamo convinti che l'unico modo che ha questo Paese di rispettare le nuove regole europee è di creare più PIL possibile. *(Applausi)*.

L'avevamo capito con la NADEF: nel Documento di economia per i prossimi anni si disegnava e si continua a disegnare qualche nota dolente per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche per le coperture dei

si dice a Roma. In effetti, purtroppo le cose non sono andate meglio da come erano state annunciate. Poi è arrivato il decreto-legge anticipi, dove sembrava che ci sarebbero state le grandi risposte ai nodi che non sarebbero stati risolti in una legge di bilancio che era stata annunciata come blindata e che doveva essere chiusa per il ponte di Sant'Ambrogio. Invece, purtroppo, il decreto-legge anticipi non ha anticipato la legge di bilancio e neanche le risposte ai nodi irrisolti.

Esatto, va creato. Una delle grandi mancanze di questa legge di bilancio e - permettetemi - delle non misure presentate da questo Governo in quasi un anno e quattro mesi dalle elezioni è che non ci sono misure per la crescita economica del Paese. Un altro membro della maggioranza ha detto che questa è una manovra espansiva, nel senso che ci sono delle risorse; ma certamente non la si può definire una manovra che produce una visione di crescita nel Paese per i prossimi anni. Anzi, di crescita qui non ci si occupa. Non c'è un passaggio che delinei una visione dell'Italia sulle politiche industriali, sulle politiche economiche, sulle politiche del commercio. Sono i settori i settori che tanto sono stati declamati - guardo il collega Franceschelli - negli scorsi giorni con il *made in Italy*, dalle grandi eccellenze italiane dell'*agrifood* a tutto il comparto agricolo, alla moda, al settore dell'industria e della chimica farmaceutica. Non c'è

più di dieci anni, possiamo dire da dodici o tredici anni in cui abbiamo ballato purtroppo non bei balli, ma siamo passati da una crisi di sistema all'altra. Lo dico anche perché spero che sia finita la storia della retorica - come dice il mio collega Manca - della maggioranza sul "noi" e sul "voi", perché adesso è toccato a voi. Nelle fasi difficili la congiuntura intorno alla quale ci si muove è negativa; abbiamo visto quando c'è stata

e ora le guerre e l'inflazione. Quindi non è che questo Governo si sia risparmiato - mi piace essere oggettiva - la sua dose di problemi. Ci sono i problemi. Ma, quando ci sono i problemi, si deve avere la capacità non solo di fronteggiare fronteggiare l'emergenza, ma anche di disegnare come uscirne. Noi ci ritroviamo che nei prossimi due anni, anzi da oggi al prossimo anno e mezzo, abbiamo una previsione di caduta degli investimenti nel nostro Paese. Gli investimenti calano

questo non è il rimbalzo del gatto morto sulla tangenziale di Roma: era un dato di una politica che ha pompato non solo risorse, ma anche investimenti strutturali strutturali nel Paese per riuscire a riprendere il tratto espansivo rispetto alla contrazione drammatica della pandemia. In questa legge di bilancio, se è vero che - da un lato - si è cercato di fare qualcosina per i bassi redditi - ricordiamoci che gli investimenti sul cuneo fiscale sono soltanto per un anno dall'altro lato, per il settore dell'impresa. Anzi, cosa assai strana, si è tolta l'unica cosa che c'era e funzionava, ossia l'ACE: un miliardo in meno. Non solo vi è un miliardo in meno sull'ACE, non abbiamo nuove politiche sul *patent* rispetto a quello che si sta facendo in Europa o negli Stati Uniti, come risposta alle politiche monetarie per attrarre investimenti, e essere competitivi e lavorare sulla crescita. Si è fatta una misura come quella del taglio sull'Ires, su cui gli stessi industriali ci hanno detto che non hanno questo problema, vogliono assumere, e mancano 800.000 persone da assumere. Quindi, vogliono la possibilità di investire sul capitale umano,

con la preoccupazione di come fare una manovra anticiclica, cioè come fronteggiare il prossimo anno e mezzo, i prossimi due anni, con quali promesse. Non servono le promesse: serve una visione di politica economica per il Paese, una visione di politica industriale. Così si costruiscono opportunità di lavoro e di reddito. Qui rispondo al senatore Garavaglia: in questa legge non c'è niente di ciò, ma ancora di più quello che è mancato in un anno e mezzo le riforme da finanziare. Solitamente nella legge di bilancio si appostano le risorse per le riforme. È evidente che noi ci siamo lamentati che c'erano poche risorse per gli investimenti, ma è anche vero che non ci sono state riforme. Dove sono le riforme di questo Governo? Dove sono le riforme per organizzarci e andare avanti rispetto alle alluvioni e alle crisi climatiche, alla grande questione ambientale? Non ci sono neanche le risorse per Prato. Ma non c'è neanche una visione di medio e lungo termine da finanziare. Le crisi non si fronteggiano in un minuto, dall'oggi al domani, quando sai già che succederanno. Non ci dobbiamo immaginare niente, non ci vuole una cartomante per dirci qual è il futuro. Sappiamo quello che succederà. La stessa cosa mi permetta di dirla sulla sanità. Sulla sanità è inutile che Garavaglia mi dica che noi non dobbiamo ragionare in termini di PIL. Signori, è così che si ragiona nel mondo. L'OCSE ci calcola così e i termini di sostenibilità di un Paese sono in base al PIL, in percentuale alla spesa. Quindi, se noi andiamo al 6,2 cento, andiamo sotto la soglia di sostentamento del 6 e sotto il 7, che è la media europea: qualcosa vorrà pur dire. Si è mai vista una cosa del genere? Abbiamo un'agitazione permanente di medici, infermieri e personale sanitario ormai da mesi *(Applausi)*. Non ricordo una crisi come questa. Dobbiamo andare agli anni Settanta per vedere il personale sanitario in piazza in questo modo, quando ancora non c'era la riforma, quando ancora non c'era il Servizio sanitario nazionale, quando c'era una situazione di grandissima difficoltà.

È cambiato il mondo e non possiamo affrontare questi temi con le stesse tabelle della Ragioneria dello Stato degli ultimi quindici anni *(Applausi)*; con lo stesso modo di ragionare della Conferenza Stato-Regioni; con il MEF che ti viene a dire che un farmaco non lo devi autorizzare perché costa troppo. Vallo a dire alla gente che che poi muore perché non ha quel farmaco, mentre chi ha i soldi va in America e se lo va a prendere. Questo è quello che sta succedendo sulla carne viva della gente. Quanti soldi ci vogliono? Quante risorse in più?

più nel Fondo sanitario nazionale. Stiamo parlando di una riforma del personale sanitario che renda competitivo essere medici e infermieri in Italia. Stiamo parlando di rimettere in piedi Aifa che è più di un anno che è bloccata *(Applausi)*, perché non riuscite a trovare un nome che vi piaccia, non riuscite a fare le nomine. E avete bloccato l'Agenzia del farmaco italiano per questo. Vergognatevi! *(Applausi)*. Nessuno ha avuto questo livello di ignavia nel nostro Paese.

gli operatori sanitari, le parti sociali e il mondo sanitario scientifico le grandissime sfide che ci sono avanti e che non si possono affrontare con questi sistemi e modelli, non ce la si fa. se non si apre una nuova stagione di riforme con tutti quanti al tavolo. Solo così, come è successo già nel passato, non si avranno scioperi e si riuscirà a concertare una strada, una *road map*, per salvare il nostro Servizio sanitario nazionale... *(Il microfono

ringrazio innanzitutto il Presidente della Commissione bilancio, i relatori e i componenti della Commissione stessa, oltre ai funzionari. La discussione della legge di bilancio per riconoscere l'impegno che tutti i commissari della Commissione bilancio mettono nel fare al loro meglio il ruolo di senatore. È anche l'occasione per ribadire le prerogative dei parlamentari rispetto alla legge di bilancio. Rivolgo quindi un ringraziamento ai colleghi della Commissione per il lavoro che hanno svolto e ai rappresentanti del Governo. Noi oggi svolgeremo due considerazioni, alcune di tipo tecnico e altre di tipo più politico. Partiamo dicendo che da anni uno dei cavalli di battaglia del centrodestra è stato il superamento della legge Fornero. Credo, dopo quello che abbiamo visto con questa legge di bilancio, che gli italiani dovranno organizzare dei comitati civici per chiedere non l'abrogazione della legge Fornero, ma la sua integrale applicazione Da quello che è contenuto sul tema pensionistico in questa legge arriva un messaggio chiaro: andare in pensione più tardi e prendere meno soldi. soldi. *(Applausi)*. È l'esatto contrario di quello che prevede l'attuale legge Fornero. Per il rotto della cuffia, sul personale medico si è sventata su questo tema una controriforma che avrebbe spinto migliaia di medici ad andare subito in pensione, aggravando così lo stato in cui versa il Sistema sanitario. Tuttavia, nonostante il passo indietro sul ricalcolo della base retributiva *ante* 1992, c'è un pesante giro di vite per quei medici che decidono di andare in pensione anticipata, anche se hanno alle spalle quarantadue anni e dieci mesi di lavoro. Sulle donne, dopo le promesse di ripristino della vecchia Opzione donna, il Governo ha ulteriormente ristretto le norme in vigore nel 2023, quelle cioè

che, con un taglio del 17 per cento dell'assegno, rischia di rivelarsi una non misura, tanto che secondo le stime vi accederanno meno di 5.000 persone. Anche gli iscritti alla ex cassa pensioni degli enti locali, la ben nota CPDEL, pagheranno un prezzo molto alto. In sostanza, sono misure che riducono la capacità di spesa dei futuri pensionati e peggiorano il loro potere d'acquisto non solo di beni, ma anche di servizi; in sostanza, li rendono più poveri. Ma non c'è solo il capitolo pensioni. Nella conferenza stampa di presentazione della manovra, la Presidente del Consiglio aveva parlato di decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli e di asilo nido gratuito per il secondo figlio. Scopriamo invece che la decontribuzione per le madri con due figli è di appena dodici mesi e che, per asilo nido gratuito, si intende un aumento del contributo alle famiglie, che però riguarderà solo quei secondi figli che nasceranno nel 2024. In fondo non ci voleva molto a capirlo, visto che, su 24 miliardi della manovra, appena 1 miliardo viene dedicato alle famiglie e alla natalità. Si introduce invece un inaspettato regalo per le famiglie che soffrono meno, con lo scorporo dei BTP fino a 50.000 euro ai fini del calcolo ISEE, sulla cui base vengono stilate le graduatorie per le borse di studio, gli alloggi universitari, i posti nel nido, le rette nelle mense scolastiche. L'unico elemento positivo è la conferma del taglio del cuneo fiscale, ma gli importi in busta paga compensano solo in minima parte l'aumento del costo della vita; così come l'aumento del Fondo sanitario nazionale non compensa gli aumenti dei costi per il sistema nazionale ospedaliero. Poi ci sono tutte le mancanze, come ad esempio la proroga del mercato tutelato, su cui bisognava avviare un confronto in Europa, spiegando che, per come è messo il mercato italiano, si sta andando non verso la libera concorrenza ma verso una tempesta che si abbatterà sulle famiglie. Di recente, ARERA ha stimato che, per via delle pratiche commerciali, scorrette, il 61 per cento delle persone che hanno accettato un'offerta telefonica ha visto aumentare le loro bollette di luce e gas. Sulla crescita, mancano misure in grado di fare da moltiplicatore economico. Manca un sostegno alle imprese per spingerle a investire con convinzione sull'innovazione e sul rafforzamento della propria competitività, come in passato è stata Industria 4.0. Signor Presidente, conosciamo già l'obiezione: non c'erano risorse. Eppure, in estate il Governo aveva trovato il modo per recuperarle, attraverso la tassa sugli extraprofitti al sistema bancario, per poi chiedere un utilizzo di tali risorse clamorosamente diverso da quello auspicato. Per non dire della mancata lotta all'evasione fiscale. I recenti dati sui versamenti IVA dicono che l'evasione è tornata a crescere, per via di una politica che, da un anno a questa parte, strizza strizza l'occhio agli evasori, con una serie di piccoli e grandi condoni fiscali. Insomma, c'erano margini di recupero delle risorse. Queste dovevano essere usate per finanziare una grande misura simbolo, per la crescita e per dare dimensione strutturale al taglio del cuneo fiscale e alle decontribuzioni per le assunzioni. Si è, invece, scelta la strada delle misure frammentate e temporanee, con un effetto nullo sulla ripresa e poca possibilità di programmazione per gli investitori economici. Non è, dunque, una manovra prudente; è una manovra timida, perché non prende di petto nessuno dei problemi strutturali del Paese quali la bassa crescita, le prestazioni sanitarie in bilico, la perdita di potere d'acquisto delle famiglie, per non dire delle promesse elettorali, quasi tutte disattese. A chi oggi pensa che la mano invisibile, a lungo andare, risolverà ogni problema senza ricorrere ad interventi da parte dei Governi, non possiamo che rispondere con le parole del grande economista del secolo scorso: nel lungo periodo, siamo tutti morti. Quindi, è tempo di darsi da fare.

del Governo, colleghi, questa, come hanno detto altri esponenti di Italia Viva, è la prima legge di bilancio totalmente vostra. Sì, perché, nella precedente occasione, vi era anche facile accampare una serie di alibi per attribuire ad altri la responsabilità di scelte a metà oppure di problemi che in qualche modo venivano ereditati. Anche se, in seguito, darò qualche dato, che dovrebbe aprire gli occhi agli italiani rispetto a problemi, che non solo non erano ereditati, ma sarebbero stati anche opportunità. Quindi, questa è la vostra visione di crescita. i vostri obiettivi, le vostre priorità. A guardarla, questa manovra, vi è una tale sproporzione, tra la capacità di comunicazione che avete dimostrato e la capacità reale di governare, che lascia quasi increduli.

Quando di mezzo c'è Giuseppe Conte, le genialate si sprecano. Quindi, non è che non sia vero che il superbonus sia stata una misura a dir poco grottesca. Stiamo, infatti, parlando di una misura con la quale, banalmente, si danno ai cittadini più soldi rispetto a quelli che davvero spendono per mettere a posto le loro abitazioni. Quindi, qualcosa che va oltre ogni immaginazione, che altera il mercato della concorrenza e che ha aumentato il tema dei prezzi. Sono tutte cose vere, ma davvero è possibile immaginare che solo ed esclusivamente questa misura abbia condizionato la vostra capacità di investimento, di crescita, di visione del Paese? Lasciatemi dubitare della solidità di questa argomentazione. Da cosa traggo la conclusione che in realtà il problema voi lo avete sul tema degli investimenti, sul tema della visione

È assente la visione sul tema della semplificazione, della velocizzazione, della riforma della pubblica amministrazione. Il tutto però è compensato da una obiettiva abilità nella comunicazione, tutta incentrata sul provincialismo, sul vittimismo e sulla chiusura a riccio. Sono tre chiavi di lettura di come voi descrivete il Paese e vi rapportate all'opinione pubblica. La Meloni ha circumnavigato il globo ormai, è stata ovunque. È davvero impegnata in un *tour* incessante,

portato il suo saluto, la sua visita istituzionale. A giudicare, però, dai risultati sul tema del Patto di stabilità e dalle figure barbine sul tema del MES che avete fatto oggi, mi convinco di un elemento, ovvero che questa è una maggioranza nella quale Forza Italia non conta più nulla, perché se ci fosse stato Berlusconi, Forza Italia non si sarebbe chinata a una figura internazionale come quella del voto contrario in Aula sulla ratifica del MES. È che ormai siamo arrivati al punto che questa maggioranza è completamente, trasversalmente, compreso il presunto centro, a rimorchio dell'ondata sovranista. Ma tornando al *tour* della Meloni, di fronte al continuo andare in giro e cercare di attribuirsi una qualche credibilità internazionale, faccio una domanda semplice, da cittadina: ma forse non sarebbe stato meglio stare un po' più nel nostro Paese per pensare a come governare l'Italia? Qualche giorno in ufficio, magari, giusto per capire cosa fare in questa manovra?

economica. La destra ha fatto della bandiera della diminuzione delle tasse uno degli elementi portanti portanti della campagna elettorale e oserei dire di tutto il suo percorso di maturazione politica nel Paese. Vi leggo un elenco che ho sintetizzato: assorbenti, tamponi, pannolini, seggiolini, alimenti per l'infanzia, casa, locazioni, ritenute IMU, imposta dei valori, immobili all'estero, accise. Mi fermo perché a Natale siamo tutti più buoni, ma potrei andare avanti. Questa è una manovra nella quale l'aumento delle tasse è trasversale e riguarda ogni categoria sociale.

Sul tema della famiglia, altro falso mito di progresso, avete costruito un racconto che ha avuto una certa presa sugli italiani: attenzione alla famiglia, fare più figli, investire sui servizi. Poi però siete arrivati al Governo. Il Governo che doveva essere più vicino alle famiglie fa saltare gli investimenti sul PNRR per gli asili e, come dicevo prima, aumenta ogni genere che riguarda l'infanzia. Io non ho capito cosa vi hanno fatti

di avere la possibilità di un briciolo di autonomia, di avere fiducia nel futuro, di fare un investimento in un'opera d'arte, in un cinema, in un teatro, in una qualsiasi forma di espressione musicale, cioè la 18app

potevano andare a vedere anche la mostra di Tolkien, non era vietato. Lo dice una persona che ama Tolkien, perché avete tentato in tutti i modi di attribuirvi anche quel gusto culturale.

quale motivo, a fronte di queste argomentazioni, rispondiate che voi date risorse solo alle famiglie poverissime. Vi do un'altra notizia: ci sono famiglie ricchissime che non amano investire sulla cultura dei propri ragazzi. È l'autonomia delle persone a fare di quei ragazzi uomini che nel futuro sappiano avere un approccio critico, che sappiano avere i propri punti di vista. Io penso che questo sia un tema su cui il Paese deve cominciare a riflettere, ma forse è bene guardare un altro falso mito del progresso, il tema delle pensioni. Infatti, ce l'avete coi bambini, con le donne, coi giovani,

veramente c'è da mettere i puntini sulle "i", perché è vero che il sistema sanitario nazionale non sta male solo ed esclusivamente per responsabilità di questo Governo in carica da un anno; è vero che i problemi strutturali del sistema sanitario nazionale sono complessi, quindi lungi da me voler far demagogia. Però in questo anno una vostra impronta in termini di riforma del sistema nazionale, di proposta di qualcosa che possa essere in grado di interrompere la spirale di crisi che c'è, un'idea, una strategia, un po' di investimenti per la riduzione delle liste d'attesa non l'ho vista. In compenso, però, ho visto uno spettacolo

a una categoria come quella dei medici, degli infermieri e delle professioni sanitarie, che durante l'epidemia del Covid hanno rischiato la vita per tutti noi *(Applausi)*, fa il balletto che avete messo in campo voi (prima tentando

significa che non ha rispetto per un segmento professionale che è il bene più prezioso che questo Paese ha e che andrebbe preservato anche dalle politiche miopi di questo Governo stesso, incapace di offrire al sistema sanitario una prospettiva.

bisognerebbe cominciare ad essere più seri e a evitare lo sfascio di tutto il sistema. che, a ragion veduta, l'unica politica che in questa legge di bilancio, dal punto di vista degli investimenti, possa essere sbandierata dal Governo sia il tentativo di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina,

Ho fatto battaglie anche quando le maggioranze di cui facevo parte non erano pienamente convinte dell'opera, quindi non sono contraria e lo voglio anche considerare un elemento capace di dare un segno sotto il profilo degli investimenti, anche in questa legge di bilancio.

decidendo che i costi del ponte fossero desumibili da un progetto definitivo. Da che mondo è mondo, un ponte di quel tipo, con una campata unica, ha determinate complessità tecniche che sono tutte affrontabili, perché siamo un grande Paese,

Come saprete portare avanti il tema della realizzazione dell'alta velocità? Quel ponte infatti è stradale, ma anche ferroviario. Quando si arriva alla fine del ponte, bisogna sapere dove andare, ma se invece di andare in una zona ad alta velocità, ci si va ad imbottigliare in una che ospita solo i treni Intercity, non è stata realizzata una cosa utile per il Paese. Non sono per mettere avanti una cosa rispetto all'altra, dico che ci vuole una visione organica, fatta di un minimo di correlazione anche intermodale,

perché i presupposti tecnici con i quali state lavorando sono molto spesso sbagliati e, in alcuni casi, costruiti sulla propaganda e sulla comunicazione. Ma guardate che poi le persone se lo ricordano se il ponte c'è o non c'è; non è che basta dire che quel ponte voi lo farete, bisogna anche farlo. E secondo me è difficile. Allora mi stupisce vedere che con una mano, la destra, si dice che si vuole realizzare il ponte e con la sinistra si cancellano dentro il piano di investimenti di RFI quasi totalmente i nuovi investimenti sull'alta velocità. *(Applausi)*. E non solo. Voi che eravate attenti alla sicurezza, voi che dicevate che i cittadini devono muoversi in sicurezza avete cancellato le risorse che

PNRR, con un colpo di bacchetta magica, 500 milioni che significano la garanzia per le persone a muoversi in sicurezza. Pensate davvero che, ogni volta che un treno è in ritardo, possa arrivare un Ministro a fermarlo? O pensate che per i cittadini ci debba essere qualcosa in più rispetto al "Lollo pensiero"? Io penso che questo sia il modo di governare un Paese.

qualcuno, cioè le forze dell'opposizione e la mia forza politica tra queste, con un protagonismo attivo, ha provato ad apportare una correzione di linea. In che modo? Lo dicevano bene prima la collega Musolino e la collega Fregolent. Noi abbiamo deciso di utilizzare le risorse del fondo parlamentare per dare un segno importante sul tema delle politiche per il contrasto alla violenza. Lo abbiamo fatto tutti assieme, come forze dell'opposizione; l'abbiamo fatto convinti che, dopo la discussione svolta in quest'Aula sulla vicenda di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne che dopo di lei hanno perso la vita a causa dei femminicidi, bisognasse dare una risposta seria e responsabile, una risposta capace di cominciare a mettere delle risorse su quelle politiche. C'erano 100 milioni a disposizione come fondo parlamentare; le forze dell'opposizione hanno deciso di non presentare emendamenti localistici (per non dire marchette) e di dedicare tutte queste risorse a una battaglia di civiltà. *(Applausi)*. Le forze della maggioranza - e vi invito a guardare cosa c'è dentro la legge di bilancio - hanno invece deciso di andare avanti con gli emendamenti localistici e di non farsi carico di un problema complessivo, rinunciando a una battaglia comune, che sarebbe stata una battaglia corretta nel merito, ma anche giusta nel metodo, perché una cultura diffusa di contrasto al tema della violenza di genere è una precondizione per far crescere nel Paese una motivazione e una reazione giusta. Non propaganda, ma fatti. Lo stesso abbiamo fatto sulla questione delle malattie rare, perché andare a scoprire preventivamente una malattia di questo tipo significa dare la possibilità a quelle persone di vivere e, in alcuni casi, di vivere meglio. Significa mettere un altro punto di innovazione, sempre in stretta coerenza con la scienza, per le persone che hanno bisogno d'aiuto. Lo stesso abbiamo fatto sull'Alzheimer, recuperando un vuoto che il Governo aveva avuto e la maggioranza con loro. Per tante ragioni, perché a noi interessa migliorare il Paese. Per tante ragioni, perché a noi non interessa fare propaganda. Per una ragione personale, perché io ho conosciuto, nella mia vita politica, due donne che per me hanno fatto la differenza nella mia idea di politica: Lisa Noja e Lucia Annibali. vi sembreremo velleitari, vi sembrerà che la nostra sia una battaglia in qualche modo da ridurre al chiacchiericcio di chi in questo momento, magari non ascolta,

perché migliorare qualcosa di sbagliato è per noi la visione più alta della politica. Voteremo contro questa legge di bilancio, ma siamo orgogliosi di averla anche per poco migliorata nell'interesse delle donne e dei cittadini...

Questo è il dato fondamentale. Voi prima di tutto avete fatto una manovra in *deficit* e avete rinunciato a prendere i soldi là dove ci sono. Ad esempio avete rinunciato al tesoretto degli extraprofitti che vi era stato dato dal Governo precedente. Non avete affrontato il problema degli extraprofitti delle case farmaceutiche e delle aziende energetiche. Basti pensare che l'Enel nei primi nove mesi del 2023 ha fatto 5,4 miliardi di plusvalenze oltre i profitti normali.

sulla questione climatica e transizione ecologica. Per fare questo bisogna avere i quattrini. Allora, anziché dare 22 miliardi di euro a chi continua a sfruttare le fonti fossili, forse è meglio spostare un po' di soldi su coloro che invece fanno qualcosa dal punto di vista del contenimento energetico, della

Come pensate di rispondere alla questione dell'Alitalia, della TIM, di Almaviva? Potrei fare decine di nomi di aziende in crisi che perdono posti di lavoro e che non avranno le possibilità che avevano prima.

sperano di avere la possibilità di avere un ascensore sociale e quindi di andare all'università. Ma per fare queste cose bisognerebbe abolire da una parte la precarietà,

che è l'unico modo per aumentare i salari e migliorare la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici senza che intervenga lo Stato, perché è un trasferimento dal capitale al lavoro. Capisco che vi dà fastidio questa terminologia: capitale e lavoro.

che vuol cercare di essere coeso, che vuol guardare a un futuro tranquillo, la prima cosa che deve fare è chiedersi come soddisfare i bisogni dei propri cittadini. Almeno, avendo io una certa età, ho sempre pensato così: come riesco ad andare in questa direzione? Voi nemmeno ci avete pensato. Non c'è quella parola, quindi non può esserci il soggetto. Avete eliminato l'unico strumento che era il reddito di cittadinanza non avete introdotto niente, scaricando sui Comuni la responsabilità di dare risposta sulla questione sociale,

contro la legge Fornero, ho perso la battaglia, quando facevo il sindacalista, contro la Fornero. Quindi, sono uno che ha fatto sempre una battaglia su questo terreno e non ho mai detto di sì. però, voi che cosa avete combinato? Abolire la legge Fornero, infatti, voleva dire continuare a dare la possibilità, alle persone che maturavano un'anzianità, di andare in pensione. Voi avete abolito l'anzianità, perché un lavoratore pubblico, se va in pensione per anzianità, paga pegno, fino a 200 euro al mese. Non so se è chiaro: perde fino a 200 euro al mese, dopo che ha lavorato magari quarantadue

che cercava di dare una risposta a una parte di medici rispetto ad altri, creando ulteriori problemi. È chiaro, infatti, che quando si dà un'impostazione alla finanziaria che fa cassa sulle pensioni dei medici, degli infermieri, delle *Authority* pubbliche,

l'unica proposta nei confronti delle donne è stata fatta da tutte le opposizioni, con un emendamento che affronta la questione della violenza nei confronti delle donne attraverso una proposta collettiva e non con le marchette a favore di ogni singolo parlamentare nel proprio territorio, facendo

che non ha nessuna prospettiva, povera, senza ambizione. Parliamoci chiaro, non ha nessun elemento strategico per il futuro. Quindi, avere almeno

e alle voci contabili, ci siamo preoccupati di entrare idealmente nelle case dei cittadini. Abbiamo sentito i loro affanni, i problemi, le difficoltà che vivono oggi, ogni giorno. Abbiamo mantenuto il rapporto di sempre, quotidiano, con il Paese reale e a lui abbiamo dedicato il nostro impegno. Con questa visione stiamo approvando misure concrete in favore di chi soffre, di coloro che vengono chiamati ultimi ma che, invece, sono i primi nei nostri pensieri e al centro della nostra azione di Governo. In questa direzione va il contributo straordinario per il caro energia, l'assegno di inclusione di 500 euro al mese per sostenere 737.000 famiglie in grave stato di difficoltà. Confermiamo la Carta Dedicata a te per l'acquisto di generi alimentari e incrementiamo i fondi per il *bonus* psicologo. Stiamo parlando di persone costrette quotidianamente a fare i conti con un sistema Paese che si porta sulle spalle anni e anni di cattiva amministrazione, un Paese che avrebbe dovuto erogare i servizi e che invece ha reso la vita impossibile ai cittadini. punto non posso che parlare di salute e di sanità. Ho sentito in quest'Aula parlare di tagli, di assalti della destra alla sanità pubblica, di smantellamento del Sistema sanitario nazionale. Non avete altri argomenti e allora usate la salute per fomentare il malessere e la paura. *(Applausi)*. Provate a dare la colpa a questo Governo se per fare una TAC ci vogliono sei-otto mesi, dimenticandovi di raccontare che in questi dieci anni in cui avete governato come azionisti di maggioranza non avete fatto programmazione sanitaria e ci avete lasciato un'organizzazione inefficiente e obsoleta ed è a causa della vostra cattiva gestione se oggi abbiamo un Servizio sanitario nazionale che costringe pazienti a interminabili liste d'attesa evitabili soltanto da chi ha la possibilità di ricorrere al privato. È il motivo per cui abbiamo alzato, sì, il fondo del Sistema sanitario nazionale a 136 miliardi di euro, cifra mai toccata prima - come fate a negare l'evidenza? con uno stanziamento aggiuntivo di tre miliardi per il prossimo anno, quattro miliardi per il 2025 e 4,2 nel 2026. Con queste risorse siamo intervenuti sul rinnovo dei contratti del personale sanitario, sull'aumento degli straordinari per medici e infermieri proprio per abbattere la lista d'attesa e sul potenziamento dell'assistenza territoriale. Dopo decenni di immobilismo, noi invertiamo la rotta. Ma la vera sfida sarà rendere competitivi i salari, questo sì, del personale sanitario, adeguandoli agli *standard* europei per evitare la fuga all'estero dei cervelli e delle nostre eccellenze. Mentre noi lavoriamo, dall'altra parte, invece, su questa manovra di bilancio abbiamo sentito troppa propaganda, fatta ingannando i cittadini con *spot* pubblicitari a favore di telecamere, con con quello che avreste fatto voi, senza tener conto del piano di realtà e la realtà la spiegava benissimo Margaret Thatcher quando diceva che non esistono soldi pubblici, esistono solo i soldi dei contribuenti ed è inutile illudersi che qualcun altro pagherà il conto, perché quel qualcun altro sono sono sempre i cittadini che lavorano e pagano le tasse. Vedete, non ci sono i soldi del Monopoli, non ci sono gli scambi elettorali con cui avete creato miliardi di buco ci sono i saldi, le coperture, il *deficit*. Certo, per voi è facile, non dovete rispondere al Paese, non dovete certo preoccuparvi che i conti tornino, perché anche quando governavate ve ne siete infischiati, prosciugando le casse dello Stato e allo stesso tempo affamando il Paese. Un'impresa difficile, ma ci siete riusciti benissimo. *(Applausi)*. La nostra ricetta, invece, è sostenere le imprese e i lavoratori alleggerendo il carico fiscale su chi produce ricchezza, tagliando i lacci della burocrazia e garantendo una giustizia rapida, perché vogliamo un Paese più dinamico, capace di produrre più ricchezza. Confermiamo pertanto anche per il 2024 il taglio del cuneo contributivo per le imprese che assumono, con l'obiettivo serio e concreto di renderlo strutturale e la revisione delle aliquote Irpef. Ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese è la nostra battaglia di sempre e lo sarà per tutta la durata della legislatura per favorire maggiori consumi, sviluppare occupazione e investimenti e per stimolare la crescita economica. Così si aumentano le risorse a disposizione dello Stato, non con le tasse, con la ridistribuzione dei profitti, ma che volgarmente si chiama patrimoniale, superando l'invidia sociale tanto cara a voi della sinistra, stando convintamente dalla parte degli italiani che si alzano presto la mattina per andare a lavorare e tornano tardi la sera, che vogliono realizzare i loro sogni con la forza del loro lavoro e non mendicando aiuti di Stato per poi perdere tempo sul divano di casa. *(Applausi)*. Un'attenzione particolare in mezzo a milioni di lavoratori che si sacrificano tutti i giorni l'abbiamo voluta dedicare al personale delle Forze dell'ordine di tutto il comparto sicurezza, impegnato con sacrificio a tutelare la nostra incolumità e la nostra vivibilità nei nostri quartieri sempre più a rischio. A loro va la nostra sentita gratitudine non soltanto a parole, ma con i fatti, destinando 100 per assicurare un migliore regime previdenziale e tutele sanitarie più forti. Una buona manovra di bilancio deve anche pensare a chi il futuro lo deve costruire. In una società dove quasi sempre entrambi i genitori lavorano, abbiamo l'obbligo, anche morale, di creare le condizioni per conciliare il potenziamento del *bonus* asilo, gli stanziamenti per i mutui sulla prima casa, l'estensione del congedo parentale sono la chiave di volta per mettere le famiglie in condizione di affrontare sfida straordinaria come è quella di mettere al mondo un bambino, un miracolo che dobbiamo consentire ai genitori di realizzare, sì, ma anche di vivere, perché fare figli significa anche avere il tempo di accudirli per crescerli. Anche sugli asili nido ho sentito veramente dire tante sciocchezze. Permettetemi di dirlo, perché è vero che in questa manovra non ci sono fisicamente, ma forse quando pochi giorni fa abbiamo illustrato il piano asili nido nel PNRR o eravate assenti o dormivate, perché c'è un investimento di 4,6 miliardi che renderanno disponibili più di 264.000 nuovi posti negli di quali tagli state parlando. Questo però non basta. Certo, di fronte all'ulteriore *record* negativo per la natalità registrata nel 2022, lo Stato ha il dovere di far sentire il proprio sostegno alle madri lavoratrici. Lo abbiamo fatto con la decontribuzione totale per donne con figli, per assicurare loro più soldi in busta paga, oltre ad incentivare ovviamente le assunzioni di donne che hanno figli. un altro modo per cominciare a colmare quel *gap* che vede le donne ottenere, a parità di mansioni, salari inferiori del 16 per cento rispetto a quelli degli uomini. Questa è la strada verso l'uguaglianza che si ottiene, non con la propaganda, non con la coreografia, il teatro parlamentare, e neanche con le lettere al Presidente del Senato per reclamare l'uso del termine «senatrice». *(Applausi)*. Ci vogliono i fatti, non le parole, i fatti sono anche che nel frattempo il Governo ha portato a termine con successo un negoziato complicatissimo in Europa sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Abbiamo scongiurato il possibile ripristino del precedente Patto e siamo riusciti a ottenere significativi margini di flessibilità che, per la prima volta, riconoscono uno spazio importante per la componente investimenti, per la spesa primaria sostenuta da quei Paesi che, come noi, sono impegnati nell'attuazione di PNRR particolarmente impegnativi. Certamente non è la migliore riforma possibile, ma sicuramente è una riforma sostenibile con queste condizioni caratterizzate, come sappiamo, dalla indisponibilità dei Governi dei Paesi cosiddetti frugali, a partire da quello socialista tedesco, che non hanno reso permanente lo scorporo degli investimenti dal computo del *deficit*. Per noi, però, l'europeismo è un valore fondante, decisivo; il nostro è e sarà sempre un europeismo maturo, adulto e soprattutto pragmatico. In definitiva, signor Presidente, questa è una manovra di bilancio protettiva e di prospettiva, che guarda all'oggi e si proietta verso il domani. Un domani che per l'Italia potrà essere finalmente luminoso, lasciandosi alle spalle le nubi e i problemi del passato grazie a questo Governo e a questa maggioranza, che hanno deciso di non lasciare indietro nessuno e di liberare le energie migliori della nostra Nazione, con buona pace dei pessimisti in servizio permanente, che anche oggi portano a casa un'altra sconfitta. Signora Presidente, chi mi ha preceduto ha detto che quando si scrive una legge di bilancio bisogna guardare al presente. Io invece penso che bisogna soprattutto saper guardare al futuro e saper leggere il passato e da quello voglio partire. Voglio partire da un anno fa, dal settembre 2022, quando il Paese era in forte crescita, il PIL era aumentato

industriale, ma soprattutto avevamo costruito per la prima volta una rete sociale che sostenesse i più deboli, perché quella che poi è diventata il bersaglio degli attacchi continui della destra non era altro che una misura di sostegno alla povertà, che esisteva in tutta Europa; mancava solo in Italia e in Grecia e noi l'abbiamo introdotta. Un anno fa c'era anche un altro elemento importante: avevamo a disposizione ben 209 miliardi di euro del PNRR, fondi ottenuti grazie al grande lavoro del presidente Conte, che, lui sì, è riuscito a frenare l'austerità europea

si utilizzasse uno strumento innovativo, gli eurobond, lo strumento del debito comune condiviso. Quei fondi servivano a continuare a far crescere il Paese su pilastri fondamentali, quali l'inclusione e la coesione sociale, la digitalizzazione e l'ammodernamento, nonché la transizione ecologica. Insomma, avete ereditato un Paese in crescita e in quella campagna elettorale avete promesso di fare ancora di più. Il vostro *slogan* era: siamo pronti a mettere fine all'austerità; siamo pronti ad abolire le accise; siamo pronti ad alzare a 1.000 euro le pensioni minime. E così, i cittadini vi hanno dato fiducia e siete andati al Governo, dove però piano piano, pezzo cominciato a demolire tutto quello che era stato costruito con fatica in quegli anni. Avete sperperato un'eredità e state sperperando addirittura il grande patrimonio del PNRR, rinunciando al raggiungimento di obiettivi che invece

Siete tornati a tagliare: alla spesa sociale, alla cultura, alla scuola (con il dimensionamento), alla sanità e, addirittura, alle pensioni, che avevate promesso di aumentare. Continuate invece a strizzare l'occhio alle *lobby* e agli evasori fiscali e poi portate avanti progetti scellerati di frammentazione del Paese, come l'autonomia differenziata, che purtroppo tra meno di un mese ci troveremo a discutere in quest'Aula: qui davvero aspetto di incontrare i patrioti di maggioranza, quando parleremo di frammentare il Paese. I dati di questo disastro non li elenchiamo semplicemente noi, ma li potete leggere in tutti i *report* economici che dicono che il PIL ormai è allo zero virgola e il debito pubblico è destinato a crescere, perché il Paese non sta crescendo, gli investimenti sono pari a zero, i consumi sono crollati all'1 per cento e la produzione industriale ormai è in crollo da nove mesi. mesi. Quella che all'inizio sembrava una furia ideologica contro le misure del MoVimento 5 Stelle, perché pensavamo - o forse speravamo - che il vostro fosse un accanimento solo verso di noi e le nostre misure, invece piano piano si sta dimostrando proprio una totale incapacità e un'inadeguatezza nella gestione del Paese. Abbiamo tutti sperato allora che finalmente in questa legge di bilancio potessimo capire quali fossero la vostra visione

su quei pilastri che avevate promesso di rafforzare. E tagli pesantissimi al *welfare*, tagli alle pensioni; la stima è che saranno tagliati, in vent'anni, ben 57 miliardi di euro, tra blocco delle rivalutazioni e tagli alle pensioni. Continuate a dirci che la coperta è corta, però poi 12 miliardi per costruire un inutile ponte li avete trovati, 2 miliardi da regalare alle banche, rinunciando ad incassare gli extraprofitti li avete trovati e non avete il coraggio di andare a reperire le risorse lì dove ci sono, dall'evasione fiscale, dagli extraprofitti bancari ed energetici, dai sussidi ambientalmente dannosi. Credo che in questa legge di bilancio questo Governo e questa maggioranza abbiano finalmente gettato la maschera. Ora almeno a noi la vostra visione di Paese è chiara. Parlo di sanità:

È chiara perché, anziché assumere nuovo personale sanitario e sbloccare il tetto delle assunzioni nella sanità, chiedete ai medici di fare turni aggiuntivi, quando in audizione in Commissione bilancio quei medici ci hanno detto che più di

E non è vero quello che sentivo dire poco fa, cioè che non c'è stata programmazione negli ultimi anni. Negli ultimi anni, rispetto ai 37 miliardi di euro sottratti al Fondo sanitario nazionale dal 2008 al 2018, da Governi di destra e di sinistra, quando il MoVimento 5 Stelle è stato al Governo sono stati investiti 27 miliardi di euro in sanità *(Applausi)*, 11 miliardi sul Fondo sanitario e 16 nella Missione 6 del PNRR. 6 del PNRR. Per la sanità dovevate lavorare a tre cose: aumento degli investimenti, per innalzare quella spesa media *pro capite* che è la più bassa d'Europa (3.200 euro, contro una media di 4.100),

diversi, quasi tutte le Regioni del Sud che non riescono a raggiungere la sufficienza nei livelli essenziali di prestazioni e ben 4 miliardi di euro che ogni anno spendiamo per la migrazione sanitaria, cioè per quei pellegrinaggi che dalle Regioni del Sud vanno verso il Nord, perché le persone al Sud non riescono più a curarsi. Per porre rimedio a questo disastro - Presidente, le chiedo un paio di minuti in più, per favore - abbiamo messo su una contromanovra scritta in ben 1.000 emendamenti, costruiti con grande fatica, con grande studio e con grande senso di responsabilità, ascoltando, come facciamo sempre, i territori, quel Sud che voi avete dimenticato, le aree interne, le famiglie, i giovani, i malati. I nostri emendamenti avevano al centro le pensioni, chiedendo di sopprimere l'articolo 33 e di ripristinare Opzione donna, il lavoro, chiedendo di detassare i rinnovi contrattuali e di potenziare lo *smart working* per i lavoratori fragili o delle aree interne, per la sanità, come vi ho detto, prevedendo più fondi chiedendo di raddoppiare le indennità di specificità per i medici del pronto soccorso, le imprese, soprattutto quelle che investono in innovazione, ricerca e sviluppo, l'ambiente, i giovani, chiedendovi di potenziare quel diritto allo studio che deve essere il baluardo su cui costruire il Paese Purtroppo, nonostante le lunghissime ed estenuanti sedute, in Commissione bilancio è stato bocciato tutto, senza un un briciolo di motivazione o di parere tecnico. Noi, con grande senso di responsabilità, anziché sperperare quei pochi fondi che erano a disposizione delle opposizioni, li abbiamo concentrati tutti in un pacchetto per il contrasto della violenza contro le donne. Voglio chiudere chiedendovi una cosa: questo è il momento, davvero, di dirci che cosa volete fare. Basta parlare di reddito: non c'è più, l'avete abolito. Basta parlare di superbonus: avete deciso di abbandonare 40.000 imprese. Basta parlare di banchi a rotelle; parlate di voi, cosa volete fare? Quali sono i vostri progetti? *(Applausi)*. Che cosa intendete mettere in campo per far crescere il Paese? Noi le nostre proposte le abbiamo, sono proposte serie, le leggete in questo disegno di legge di bilancio e in tutte le proposte che continuiamo, con grande senso di responsabilità, a depositare nelle Commissioni e in Aula. Noi vi chiediamo di diventare finalmente una forza di maggioranza, di cominciare a lavorare per costruire e non per distruggere, Presidente, perché riteniamo che nel momento di grande fragilità in cui si trova il Paese, davvero serva dalle istituzioni il segnale di attenzione e di ascolto che metta le persone al centro e faccia capire loro che in quest'Aula si lavora per il loro bene e non per il bene degli amici, a cui abbiamo regalato mancette anche in questa legge di bilancio.

mi rendo conto che, in certi casi, i concetti tendono a ripetersi. Quindi, cercherò di dire soltanto le cose che non sono state dette da altri. di alzare un minimo di sopracciglio su un paio di concetti che ho sentito essere ricorrenti negli interventi dei colleghi dell'opposizione. La collega Castellone ha terminato il suo intervento scagliandosi contro le mancette, gli interventi localistici o cose di questo tipo.

fra i tantissimi emendamenti localistici e le mancette per gli amici, ce n'era una che mi aveva sinceramente fatto inquietare, che erano gli 1,3 milioni dati alla Badia di Pattano dal senatore Castiello, che mi dispiace non vedere in Aula. È bastato fare una piccola ricerca per scoprire che era un'abitazione privata. Sarà stata di grandissimo pregio architettonico, non ne dubito, però è un'abitazione privata dei signori Giuliani e De Luca, non si sa per quale motivo sono stati gratificati di 1,3 milioni dello Stato da parte del senatore Castiello. Quindi, io starei un attimo attento a scagliarmi contro il Governo dicendo queste cose, perché qui, negli interventi localistici della maggioranza, che difendo con orgoglio, ho visto scuole, ho visto caserme, ho visto strade *(Applausi)*, che magari sono sfuggite all'attenzione dei Governi precedenti e quindi è giusto che i senatori e i deputati, quando hanno la possibilità, possano anche dire la loro, magari stanziando cifre piccole, ma importanti per i territori. Questo lo rivendico con forza: dare dei soldi a una casa privata di qualcuno forse un po' meno. Vediamo di rimettere le cose a posto. Altra cosa che

Ci sono due categorie di persone che vanno a prendere i soldi dove ci sono contro il consenso degli interessati.

Non capisco perché si chieda a questo Parlamento di fare dei furti nei confronti della gente. Uno può anche dire che per questioni politiche si possono dare più incentivi a uno e meno incentivi all'altro, ma di fronte alla ripetizione ossessiva che non siamo andati a prendere i soldi dove ci sono, dico ma menomale che non siamo andati a prendere i soldi dove ci sono ci sono perché evidentemente qualcuno li aveva guadagnati con qualche merito. In tutti gli anni passati invece, a furia di tasse e balzelli, spesso e volentieri gli italiani si sono ricordati che andavano a prendere i soldi dove c'erano e anche dove non c'erano. Ci siamo difesi

Per il resto vorrei sottolineare una cosa: perché secondo voi l'opposizione si concentra su queste due cose che sono oggettivamente fumo negli occhi?

e i contratti di lavoro degli italiani. Questo è, basta guardare i numeri. La voce più grande è data dalla conferma del taglio del cuneo fiscale, che significa che si conferma quell'aumento in busta paga che tutti gli italiani hanno visto l'anno scorso.

Ci sono 3 miliardi che vanno in sanità e la stragrande maggioranza va nel rinnovo dei contratti dei medici che avranno finalmente un meritato ritocco al loro stipendio. Non basta; le le voci sono quelle, il resto balla pochissimo. Ci sono 12 miliardi di cuneo fiscale e quindi aumento degli stipendi, 3 miliardi di abbattimento delle aliquote e quindi aumenti di stipendio, 5 miliardi di aumenti contrattuali e 3 miliardi per la sanità. Rimane poco altro. Ciò significa che tutto quello che c'era è probabilmente poco, ma tutto quello che si poteva trovare date le circostanze è stato messo sugli stipendi. Questa è stata una scelta politica. Perché sugli stipendi e non su altro? Semplice perché gli stipendi sono quelli più danneggiati dall'inflazione, perché tante famiglie, specialmente quelle dell'ex ceto medio, che non avevano mai avuto problemi, si sono trovate oggettivamente in difficoltà. È ovvio; se in un anno c'è un aumento del costo della vita dell'8 per cento, l'anno dopo del 5,30, come accaduto in questi due anni, significa che in assenza di rinnovo di contratti, di aumenti contrattuali e di taglio del cuneo fiscale, la capacità di spesa di queste famiglie diminuisce di quasi il 15 per cento. È una cosa pesantissima. È per questo che noi abbiamo concentrato tutte le risorse, per poche che fossero, sugli stipendi. Questo serve anche a far capire accade in certi casi alle categorie che certi partiti hanno costantemente tutelato. Si pensi, per esempio, alla Lega.

di stagnazione economica noi abbiamo sempre cercato, per quel poco che era nel nostro potere, di indirizzare quante più risorse possibile verso queste categorie e ci aggiungo anche i pensionati. mi rendo conto e ci siamo tutti resi conto che ci sono dei momenti in cui alcune categorie vanno più in difficoltà di altre. In questi casi, delle categorie suppostamente difese dalla sinistra - quando invece sappiamo benissimo che erano i primi ad

Però la direzione politica deve saper parlare alla gente e saper capire quantomeno che lo Stato cerca di essere, per quanto possibile, stanti gli enormi vincoli a cui le nostre finanze e la nostra capacità di intervento economico sono sottoposte, al fianco di queste persone. Penso pertanto che la difficoltà della sinistra è di dover ammettere che noi stiamo cercando di aiutare le categorie che loro difendono a parole, mentre noi lo facciamo con i fatti; è una cosa che la sinistra ha qualche problema ad ammettere *(Applausi)*, mentre invece noi lo facciamo.

le pensioni sono sostanzialmente bloccate nella loro rivalutazione dai tempi della cosiddetta legge Fornero, perché la prima cosa che fece la Fornero fu un taglio di tre anni di tutte le rivalutazioni. Nel nostro caso, sia quest'anno che l'anno scorso - se ne stanno accorgendo tutti i pensionati che ricevono il loro cedolino -, i pensionati trovano un aumento in certi casi consistente. È la prima volta che, pur essendo delle cifre importanti che pesano tantissimo sul bilancio dello Stato, questo Governo ha deciso di riconoscerle fino a livelli importanti di pensione: fino a cinque volte la pensione minima la rivalutazione è piena; ciò significa che fino a cinque volte il minimo della pensione l'anno scorso è stato firmato per tutti un aumento costante, mese per mese, *ab aeterno*, dell'8,3 per cento e quest'anno del 5,5 È una cosa di cui tutti si sono accorti. È per questo che non c'è indignazione nel Paese, perché tutti sanno e vedono nei cedolini delle pensioni che l'aumento c'è e che non c'era mai stato anche quando l'inflazione era più bassa e quindi sarebbe bastato mettere delle cifre molto più esigue nelle tasche dei pensionati. Invece in questo caso le cifre sono importanti, impattano molto sul bilancio e noi le abbiamo versate tutte. Anche chi ha una pensione molto alta - in certi casi sappiamo che non tutte sono coperte dai contributi - ha avuto una parte

ma ci sono tanti miliardi in più per i pensionati: non serve neanche argomentarlo a voce, perché semplicemente la verità è data dai cedolini; basta porli uno di fianco all'altro e ci sono aumenti anche importanti. Questa è una delle cose positive. Di solito la vita del parlamentare di maggioranza non è che sia rose e fiori, perché non si fa mai abbastanza, ma devo dire che in ogni caso il ringraziamento di tanti pensionati è una cosa che oggettivamente mi rincuora.

quello che non passa da una parte passa dall'altra, ma passa peggio. Pertanto, chiudiamo questo esperimento. Ci abbiamo provato. L'intento era sicuramente buono. L'intento era quello di sveltire le procedure, di fare un provvedimento veloce, in modo tale da poter presentare internazionalmente una immagine di velocità e di serietà. Ma c'è un motivo per cui questo è il Parlamento. Il Parlamento è la sede del potere legislativo e non deve essere la sede del potere approvativo. L'ho detto tante volte.

In ogni caso, anche il potere approvativo sarebbe un potere importante e ringrazio i colleghi del MoVimento 5 Stelle che, insieme con noi, oggi hanno approvato il parere sempre parlando di opposizioni unite. È stato un gesto che riconosco. È stato anche un momento importante per il nostro Stato

i vincoli di finanza, che sappiamo benissimo essere quelli che piacciono tantissimo al Partito Democratico, che ne vorrebbe di più: vorrebbe più vincoli, più gente che ragiona per noi invece della democrazia. riesce, in ogni caso, per quel poco che ci rimane, a indirizzare le risorse dove servono di più. Quindi, io sono orgoglioso di questa legge di bilancio. Sono orgoglioso di come è stata portata avanti e orgoglioso anche degli emendamenti localistici, perché, in certi casi, servono anche quelli. Al momento

mesi dal giuramento. Per suo tramite, signor Presidente, mi rivolgo subito al Governo, alla maggioranza, ai colleghi di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, con due semplici domande. Quando concentrerete le vostre energie nel valutare l'azione del vostro Governo, l'impatto delle misure che avete adottato sulla vita reale, sulle famiglie e sulle imprese, i risultati raggiunti, l'efficacia delle vostre misure? Lo dico con chiarezza. Voi avete una responsabilità di fronte agli italiani, che è quella di governare e garantire un futuro a questo Paese.

tra un po' il Paese non vi seguirà e l'Italia si sveglierà nel buio totale, senza misure per il futuro, senza misure per la crescita, con più disuguaglianza e con meno giustizia sociale. tutti i colleghi del Gruppo Partito Democratico che sono intervenuti, i colleghi della Commissione bilancio, che ringrazio per il lavoro impegnativo svolto, hanno argomentato molto bene, non solo le critiche, ma soprattutto le proposte, cioè l'idea di società e di Paese alternativa alla vostra. Vi dico nell'interesse del Paese, colleghi della maggioranza, che state dedicando troppo tempo a valutare il passato. Così facendo, dimenticate il presente e con questa legge di bilancio dimostrate che siete senza futuro. Voi avete costruito questa legge di bilancio dove il futuro non esiste. Ecco le ragioni per le quali la vostra manovra è senza respiro, espansiva tecnicamente solo per effetto della proroga di un solo anno del cuneo fiscale contributivo. Ma diciamocelo con chiarezza: non un euro in più per i redditi dei lavoratori fino a 35.000 euro nel 2024 rispetto al 2023, pur di fronte a un'inflazione insostenibile che ancora pesa drammaticamente in maniera disuguale sui redditi delle famiglie, a maggior ragione su quelli più bassi. Una manovra per due terzi in *deficit*, senza misure per la crescita, una manovra solo capace di sovrastimare la crescita e di sovrastimare anche il contributo dell'1 per per me è insostenibile. Rischiate di dover privatizzare gli assi portanti dello sviluppo di questo Paese. Rischiate, cioè, di togliere dalla mano pubblica gli assi più importanti per la programmazione di un nuovo sviluppo economico. una manovra dunque senza futuro, che - peggio ancora - guarda al 2024, ma rischia di lasciare tra la metà e la fine del 2024 il nostro Paese a un bivio pericoloso, senza alcuna indicazione su dove andare. quattordici mesi di comizi, tutti finalizzati a rafforzare la *leadership* della Presidente del Consiglio. Ma è evidente che in questo contesto cominciano a emergere grandi contraddizioni, divisioni interne alla maggioranza, veti e contrappesi e grandi difficoltà nell'affrontare le riforme necessarie per rimuovere i problemi strutturali del Paese. *(Applausi)*. Ci sono nodi strutturali ancora più evidenti dopo una pandemia globale. Guardiamo innanzitutto il versante europeo: siamo primo importante fallimento proprio sull'asse portante delle politiche dello sviluppo economico che riguardano le famiglie e le imprese. Non sono stati sufficienti, Presidente, i tanti incontri bilaterali, i tanti viaggi, le tante foto e le tante immagini di relazioni tra il vostro Governo e gli altri Governi in sede europea. Era Era evidente, era tutto prevedibile e la ragione di fondo è che a voi mancano le radici dei valori europeisti, quelle necessarie per definire le alleanze in Europa, per costruire una nuova Europa. Voi non avete nulla a che vedere sul piano culturale con l'Europa di De Gasperi, di Spinelli, di Kohl, di Mitterand, di Monnet. *(Applausi)*. Le vostre radici sono diametralmente opposte al bisogno di un'Europa coraggiosa

Abbiamo bisogno di un'Europa coraggiosa sulla strada delle transizioni ambientali, digitali e sociali, che sappiamo bene essere l'ambito necessario e ottimale. Dobbiamo progettare insieme il futuro delle nostre produzioni industriali. Ma, se questa maggioranza, per regolare i consensi interni, utilizza l'Europa per alzare i conflitti, per rivendicare un presunto orgoglio nazionale, in contrapposizione sempre con l'interesse nazionale, con le vostre azioni e le vostre iniziative, invece, rischiate di rendere l'Italia più debole, più sola, più isolata, meno centrale nelle dinamiche dello sviluppo economico e sociale di un nuovo piano di crescita. Il fallimento dell'iniziativa del Governo sul Patto di stabilità e l'accordo che avete subito è solo in sintonia con un vostro obiettivo, purtroppo pericoloso per le famiglie e le imprese italiane, che io definisco "il tirare a campare". Ecco alcune deroghe che emergono Ecco alcune deroghe che emergono fino al 2027, che rischiano di non garantire un futuro chiaro, un programma strategico, un piano di sviluppo economico-sociale, in particolare sugli investimenti. Sono deroghe alla contabilizzazione degli interessi sul debito, sono deroghe al rientro sul *deficit*. Non è un successo: è un "tirare a campare" di fronte a una mediazione al ribasso che non siete stati in grado di costruire, perché non avevate né le alleanze, né le idee. Avete criticato l'accordo proposto dalla Commissione europea. Avete attaccato anche direttamente il commissario Gentiloni. Ma poi avete venduto al ribasso un accordo che ha peggiorato la proposta della Commissione europea e che rischia di pesare anche sulla crescita del nostro Paese. Portare l'industria e il lavoro nella transizione ambientale dovrebbe essere un obiettivo, il cuore portante delle politiche economiche del Governo. Formare le risorse umane e garantire ai nostri giovani percorsi di formazione importanti aggiuntivi per abbracciare la sfida della transizione devono rappresentare l'ossessione del Governo. Invece nulla, nessuna idea sullo sviluppo, nessuno progetto sulla crescita, nessuna idea sullo sviluppo economico e strategico del nostro Paese. l'Aiuto alla crescita economica (ACE), l'unica misura che avrebbe consentito alle piccole e medie imprese di aumentare i propri capitali non a debito e di rientrare maggiormente nella filiera possibile del credito per realizzare investimenti nell'innovazione e nello sviluppo. L'unica misura che c'era l'avete cancellata senza indicare una prospettiva diversa allo sviluppo economico del nostro Paese. Colleghi, il difficile sentiero per la gestione del nostro debito pubblico passa da una maggiore crescita, che per noi deve essere inclusiva, orientata a ridurre le disuguaglianze, più giusta. Per noi, rimuovere la precarietà, alzare i salari, rafforzare la contrattazione collettiva, definire il salario minimo, sono provvedimenti indispensabili per una nuova competitività economica del nostro Paese. Dovete concentrarvi sui numeri reali. Occorre capirli: se in Italia gli stipendi non aumentano dal 1991 e negli ultimi trent'anni abbiamo avuto una crescita misera del più 1 per cento,

Dovreste pensare alla scuola, alla formazione, all'università, alla salute come un investimento, uscendo dalla logica di spesa e di costo. Questa doveva essere la sfida dell'Italia in Europa, anche chiedendo a Eurostat una riclassificazione della spesa come un investimento. Come abbiamo fatto per la ricerca doveva essere fatto per la salute, per la formazione, perché sono investimenti soprattutto al crescere dello sviluppo della ricerca. La sanità ha bisogno di essere ripensata come un investimento strategico, non come un luogo di menzogne, non come il luogo dove giochiamo sui numeri.

a pagamento per chi ha i soldi. *(Applausi)*. State cominciando a rompere il profilo dell'universalità. È di questo che siamo preoccupati, perché in questa rottura non si produce più sviluppo economico, si producono solo più disuguaglianze e si rischiano nuovi conflitti.

Vi abbiamo proposto iniziative per calmierare il costo degli affitti per gli studenti, e non ci avete dato risposte. Ci avete lasciato senza risposte, non siete pervenuti. Il Ministro non si è presentato a discutere della necessità che il Paese ha di garantire agli studenti affitti accessibili, perché l'esigenza che abbiamo di formare i nostri giovani al futuro è strategica, decisiva e non potete abbandonarli. Vi abbiamo proposto un patto e una nuova proposta sulla sanità per sbloccare il tetto delle assunzioni, per risolvere il problema delle liste d'attesa, configurando perfino un'idea e una disponibilità a sedersi a un tavolo sulle riforme. Nulla: si risponde con la provocazione e la mistificazione dei numeri. Vi abbiamo proposto il salario minimo e ci rispondete con una delega geneticamente modificata. Colleghi, aiutare i lavoratori, quelli più fragili, garantire una maggiore sicurezza del lavoro dovrebbero essere non una questione dell'opposizione, ma un'esigenza del Governo *(Applausi)*, per garantire competitività economica e maggiore giustizia, tornando a restituire centralità e dignità alla parola lavoro. Il Ministro del lavoro? Non pervenuto: nessun parere su nessun emendamento è stato mai valutato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, vi abbiamo proposto una misura che abbiamo ritenuto molto importante, quella di evitare i tagli lineari sulle Regioni, sugli enti locali e sulle Province, perché nel frattempo state ripristinando anche la stagione dei tagli lineari: nessuna risposta.

se non investiamo nella formazione delle risorse umane nelle scuole, rischia di lasciare una società sempre più in conflitto, sempre più rancorosa e sempre più violenta. Abbiamo fatto una proposta abbiamo avuto gli applausi da parte della maggioranza. Non abbiamo avuto, però, quello che chiedevamo, signor Presidente, ossia la disponibilità della maggioranza a convergere con noi su un'unica misura, per le poche risorse a disposizione del Parlamento, che poteva servire al Paese. La maggioranza ci risponde con l'apertura - come ha detto il collega Borghi - della nuova stagione delle mance 2.0: avete perso un'occasione. Ora, proprio per queste ragioni, cominciamo a pensare che siate senza futuro: cominciate a cambiare strada, cambiate politica riprendete il sentiero delle riforme, quelle che servono al Paese, non quelle che servono a distrarre il Parlamento e l'Italia dalle priorità vere. Signor Presidente, gentili colleghe, cari colleghi, discutiamo oggi una legge di bilancio frutto di un lavoro complesso, che si è posto un obiettivo essenziale: la ripresa economica e quindi il rilancio del sistema Italia, Italia, fatto di lavoratori che hanno voglia di produrre e di famiglie che vanno sostenute, perché sono una fonte insostituibile e preziosa di ispirazione e di esempio per le generazioni future e svolgono un servizio essenziale per il bene comune. Non è stato facile, con una disponibilità di risorse tanto limitata. Ma, se il compito, l'onere e l'onore, direi, della politica è fare una sintesi delle esigenze e delle necessità, vi assicuro che abbiamo lavorato e fatto ogni sforzo per la migliore possibile. *(Applausi)*. Ringrazio i colleghi di Commissione, di maggioranza e di opposizione, i relatori Liris, Testor e Damiani in special modo il presidente Calandrini per il lavoro svolto. Come ho detto, abbiamo posto la massima attenzione alla ripresa economica, ma con serietà e rispetto per la solidità dei conti pubblici. Abbiamo riservato il dovuto sostegno di risorse alle fasce deboli: mi riferisco, per esempio, alla conferma per l'anno 2024 del taglio contributivo, con un aumento in busta paga che corrisponde mediamente a circa 100 euro al mese. L'effetto di questa misura non si esaurisce certo nel beneficio economico concreto per il lavoratore, ma si estende a tutto il sistema imprenditoriale, per il quale - com'è noto - l'elevato costo del lavoro costituisce indubbiamente un freno alla nuova occupazione, con ciò che ne consegue anche in termini di perdita di competitività. Anche la delocalizzazione è perdita di competitività, oltre che di occupazione: le imprese italiane devono poter restare a produrre in questo Paese. Con la misura del *reshoring* abbiamo introdotto un abbattimento del 50 per cento delle imposte per le aziende che rientrano dall'estero con i propri impianti di produzione e restano qui, in Italia. È importante anche l'attenzione che abbiamo riservato alle aree del nostro Paese con maggiore criticità: 1,8 miliardi di euro a sostegno degli investimenti privati sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese ubicate nel Mezzogiorno, con una ZES unica. Il nostro Sud deve diventare attrattivo per aziende e investimenti. Serve coraggio per abbandonare alcune dinamiche e comportamenti al netto di ogni logica assistenzialista, che ha dimostrato tutti i suoi limiti, se non i danni. E da meridionale vi posso garantire che questo coraggio c'è. *(Applausi)*. La gente del Sud vuole il cambiamento tanto quanto tutti gli altri. Ed è determinata più che mai a consegnare al tempo andato il luogo comune per eccellenza, ovvero il malcostume sedimentato di quei territori, convinta più che mai che le virtù e le capacità dei singoli e delle comunità possano e debbano fare la differenza rispetto al passato. Per il comparto primario, invece, abbiamo cercato di rifinanziare quelle misure che si sono rivelate particolarmente utili, in modo da concentrare le risorse dove effettivamente servono. Tutti comprendiamo l'importanza di questo settore, a cui - lasciatemelo dire - dobbiamo tanto, visto che ci dà cibo e quindi anche vita, ma al quale chiediamo anche tanto. Gli agricoltori e gli allevatori sono chiamati a sforzi straordinari: produrre nel rispetto dell'ambiente, con sistemi a basso impatto ambientale, ma anche ad elevato costo; un ambiente che tuttavia è sempre più ostile, con fenomeni climatici che quasi sempre sfiorano la catastrofe. Non c'è un settore nel quale gli effetti del cambiamento climatico in atto siano più devastanti e questo ovviamente è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo già detto che gli agricoltori, lungi dall'inquinare il nostro pianeta, stanno invece dando un contributo essenziale al suo risanamento. Stiamo incentivando le pratiche agricole e forestali che sequestrano carbonio, con l'obiettivo però di garantire un'elevata qualità degli assorbimenti ed evitare ogni ecologismo di facciata. Chiediamo di testare in campo le nuove tecniche genomiche, perché costituiscono un'innovazione che il mondo agricolo non può non cogliere. Abbiamo stanziato ulteriori risorse (25 milioni per il 2024 sul Fondo innovazione) per sostenere le aziende nella transizione digitale, necessaria a realizzare sistemi di produzione che consentano di risparmiare gli *input* produttivi, compresi i fertilizzanti e i pesticidi, nonché un uso più razionale della risorsa acqua. Abbiamo istituito il Fondo per le emergenze, con una dotazione di 270 milioni nel triennio, che possa sostenere le aziende agricole della pesca e dell'acquacoltura non solo di calamità, ma anche di crisi di mercato. Interveniamo nel settore ortofrutticolo, particolarmente sofferente non solo per gli effetti del clima, ma anche per l'aumento dei costi di produzione. esempio ai territori che sono stati colpiti dall'alluvione, con dei prestiti cambiali erogati a condizioni particolarmente vantaggiose da Ismea. Abbiamo anche incrementato l'organico di Agea, perché i controlli sono indispensabili per l'attuazione del piano strategico della PAC. incrementato l'indennità spettante al personale dell'Ispettorato per la qualità e repressione frodi, in considerazione della delicatezza dei compiti e delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, che vengono svolti. Abbiamo finanziato la legge n. 499, per sostenere la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo. Per il settore della pesca abbiamo rifinanziato l'indennità per il fermo pesca temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ed esteso alle imprese della pesca e dell'acquacoltura gli interventi compensativi previsti in favore delle imprese agricole che subiscono danni da calamità. Si tratta di un intervento particolarmente atteso dal settore, che include la possibilità di beneficiare degli sgravi contributivi. È previsto anche il rifinanziamento della nuova Sabatini per il sostegno agli investimenti produttivi, con un incremento di 100 milioni di euro per il 2024. È una manovra - come dicevamo in precedenza - che punta al rilancio produttivo del Paese, ma che al contempo è vicina ai più bisognosi. Tra le misure ricordo la priorità dell'accesso al Fondo di garanzia sui mutui per l'acquisto e ristrutturazione della prima casa, a favore delle famiglie numerose con almeno tre figli *(Applausi)*, e la riconferma delle agevolazioni per le giovani coppie. coppie. L'Italia deve fronteggiare un inverno demografico importante. Gli ultimi aggiornamenti Istat relativi a natalità e fecondità nel nostro Paese per l'anno 2022 fotografano indicatori e dati al ribasso: dati a dir poco sconfortanti. È una tematica che vogliamo porre al centro delle nostre politiche, con interventi concreti. Come ha affermato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società e, quindi, lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali. Vogliamo smontare la narrativa per cui la natalità è un disincentivo al lavoro. Vogliamo incentivare chi mette al mondo dei figli e ha voglia di lavorare. Mi avvio alle conclusioni, Presidente. Ci accingiamo a votare una legge di bilancio che è in linea con le priorità di crescita di tutto il sistema Paese. Abbiamo lavorato con diligenza, responsabilità e dedizione per garantire che ogni intervento fosse calibrato rispetto alla necessità, nella convinzione che l'unica vera manovra in grado di rilanciare il nostro Paese debba prescindere - come dicevo in precedenza - da qualsiasi logica assistenzialista, da qualsiasi tentazione di disperdere le risorse in tanti interventi, senza un reale impatto strutturale e duraturo, quindi senza cambiamento. Misure per spingere la crescita e incentivare la produzione, riducendo le tasse e incentivando le assunzioni, si sommano a interventi per sostenere concretamente le famiglie e bisognosi. Tutto ciò che facciamo guarda al futuro del nostro Paese, che abbiamo ereditato dai precedenti Governi e che è nostro compito migliorare e far prosperare. Questa è la destra e questo siamo noi.

che ieri ho cercato di spiegare in quale contesto è stata fatta questa manovra di bilancio e le scelte che il Governo ha voluto fare. Ma da alcuni interventi da parte dei colleghi

sono state iniettate molte risorse e introdotte molte misure di sostegno. Questo è vero, ma le regole forse erano un po' diverse. Ricordiamo che nel periodo pandemico è stata tolta la clausola sul Patto di stabilità

la misura che ha rimesso in moto il mercato edile. Ma questa misura ha un costo: stiamo parlando di 100 miliardi, per i quali noi ogni anno paghiamo una rata di 20 miliardi per rientrare come debito. Oltre a questo, è intervenuto l'aumento dei tassi voluti dalla BCE: stiamo parlando di 13 miliardi. Quindi, se la matematica non è un'opinione, 20 miliardi più 13 miliardi sono risorse maggiori rispetto a questa manovra. È evidente che, se avessimo avuto maggiori risorse, questa manovra avrebbe sicuramente contenuto ulteriori misure per incentivare e soprattutto essere più espansiva. Come dicevo prima, però, si tratta di scelte. Si è scelto di incentrare la manovra a sostegno di famiglie e lavoratori, anche se nei vari interventi sembra che questo non sia stato recepito da parte dei colleghi, nonostante la maggior parte delle risorse vada proprio in questa direzione. È una scelta che abbiamo preso perché riteniamo che aiutare le famiglie e i lavoratori con redditi più bassi aiuti a dare

l'affermazione che certamente ha giocato un ruolo anche la vitalità osservata nel mercato del lavoro, oltre alla scelta di voler lasciare nel reddito dei lavoratori maggiori risorse. Sono scelte. Il Governo ha deciso di impegnare queste risorse verso tali scelte. Sono scelte anche le vostre, come quella di aver fatto un emendamento comune sulla violenza contro contro le donne: una scelta nobile che condivido, perché obiettivamente sono una donna anch'io, sono sensibile al tema, ho una figlia, faccio parte della Commissione d'inchiesta contro il femminicidio. contro il femminicidio. I vostri emendamenti che magari andavano a sostenere altre categorie di fragili sono stati messi da parte. E questa è stata una scelta che chiaramente non può ricadere poi sulle spalle della maggioranza. Come è stato scelto da noi di di non erogare più il reddito di cittadinanza. Per quale motivo? Noi vogliamo investire sul lavoro e, quindi, non è questione di fare una misura per essere contro un partito, ma perché obiettivamente la nostra economia è stata fermata dalla mancanza dei lavoratori. Non si può pensare di produrre se non si hanno i lavoratori.

Aula la discussione generale con 53 interventi (compresi anche quelli di ieri sera). Questo a dimostrazione di una partecipazione oggi di tutte le forze politiche e soprattutto anche delle forze economiche e sociali del nostro Paese, che hanno dato il loro contributo anche critico, perché governare non è mai semplice. Voglio soltanto sottolineare alcuni aspetti, non per difendere la manovra finanziaria; lo abbiamo fatto già negli interventi e la difendiamo anche perché è una manovra che guarda alla situazione attuale del Paese

a causa di una congiuntura economica difficile a livello internazionale (che non è una scusa, ma una fotografia reale della situazione internazionale che ha ricadute sul nostro Paese e su tutta l'Europa), alcune stime sicuramente riviste non abbiamo sovrastimato, come qualcuno ha detto poc'anzi in quest'Aula, delle stime; le abbiamo invece rese reali. Quindi è una manovra prudente, come più volte ha sottolineato anche il ministro dell'economia e delle finanze

situazioni che vengono dal passato, ma noi non aggiriamo l'ostacolo: il problema lo conosciamo, lo affrontiamo e oggi, anche in questa manovra economica, continuiamo a mettere risorse come non mai sulla sanità,

la nostra parte. Però nella manovra finanziaria oggi ci sono risorse in più per il Servizio sanitario nazionale. Che serva una riforma organica e importante oggi, alla luce delle delle stesse evoluzioni della sanità, questo è vero e necessario. Però credo che in un anno di Governo si sia fatto molto e noi siamo interessati oggi ad affrontare questo problema. di Governo ha dimostrato anche sulla manovra finanziaria unità di intenti e questo voglio evidenziarlo e sottolinearlo. Abbiamo trovato le sintesi giuste per poter rimarcare le politiche che

Questo è oggi il sunto del dibattito avvenuto in quest'Aula.

forse fuorviato o troppo condizionato da quello che è stata la mia attività precedente di assessore regionale, quindi di persona che teneva i bilanci in mano.

Si consideri che meno 33 è il dato di partenza, cioè 33 miliardi sono il dato non disponibile per la manovra libera. Quando parliamo di manovra libera, parliamo di tutte le spese e le imputazioni di spesa non vincolate, cioè quelle che uno Stato può utilizzare per disegnare la programmazione di un Paese. Quando a questi 25 miliardi non posso sommare i 33 che devo togliere per i 20 del superbonus e i 13 dei tassi BCE, di fatto io sto mortificando una manovra

la disabilità e tutti i contesti che sono stati enfatizzati, tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza. Questo dato deve essere ben fissato nella mente. Vedo in Aula il sottosegretario Freni, che, da questo punto di vista, vista, è l'esponente del MEF che ha seguito, insieme agli altri, l'ambito del bilancio e dei saldi di bilancio. Trentatré miliardi in meno sono un grosso ostacolo da gestire, soprattutto quando si vanno a chiudere i bilanci e i saldi non tornano. Pertanto, i complimenti al Ministero e al Governo, qui rappresentato dal ministro Ciriani, che ringrazio per l'attività di collante, e dai Sottosegretari,

progetta un futuro, e che sono, appunto, il lavoro e la sanità. Sul lavoro, il messaggio che va enfatizzato, e non è stato fatto abbastanza, è nel cambio di paradigma che c'è stato rispetto a Governi precedenti. Io non condanno Io non condanno scelte politiche. Io dico che si è orgogliosamente diversi, che orgogliosamente si è rappresentati in Parlamento in maniera diversa e che orgogliosamente sono gli italiani che scelgono chi deve gestire la cosa pubblica. In questo caso, la scelta degli italiani è andata a italiani è andata a responsabilizzare delle forze che non scelgono un sistema assistenziale, quindi di tutelare coloro che hanno deciso di essere assistiti dallo Stato, ma

Questo non significa, chiaramente, che chi non è in condizioni di lavorare viene dimenticato. Al netto di coloro che sono in condizioni

alla novità delle polizze assicurative sulle catastrofi naturali. Io ritengo questa una novità eccezionale, una grandissima intuizione di questo Governo perché ormai abbiamo capito che il nostro Paese è molto fragile, il ricorso delle polizze assicurative può essere un giusto modo per garantire lo Stato, garantire la ricostruzione, ma garantire anche i saldi di bilancio delle casse dello Stato. Pertanto, sono novità importanti di una di una legge di bilancio matura, consapevole, sobria, responsabilizzante e responsabile nei confronti del Paese e dell'Europa, ma soprattutto di un Governo che sa chi siamo, sa che Paese stiamo vivendo, sa qual è il contesto in cui questo Paese vive oggi, ma soprattutto sa dove questo Paese vuole andare.

in sede di replica, tuttavia il Governo tiene a fare una breve replica, direi più una replica di metodo che di merito alla discussione generale di questa legge di bilancio. Una discussione generale, almeno rispetto alle ultime che ho avuto modo di seguire, modo di seguire, insolitamente e felicemente ampia e affollata. Inizierei con una frase che credo mi sentirete dire pochissime volte in quest'Aula, ma ha ragione la senatrice Paita: questa è la nostra legge di bilancio. Questa è una legge di bilancio orgogliosamente politica e una legge di bilancio cui questo Paese da troppo tempo forse non era abituato, una legge di bilancio che dopo tanti anni è espressione di un indirizzo politico ed è ovvio che, a fronte dell'espressione di un indirizzo politico, si possa non essere legittimamente d'accordo. Forse eravamo tutti un po' anestetizzati, camminavamo in quello che Brock chiamava lo stato di sonnambulismo che derivava dalla assuefazione che derivava dalla assuefazione a tanti anni di Governi tecnici e non siamo più abituati, oggi, a dire con orgoglio che questa è una legge di bilancio politica una legge di bilancio politica *(Applausi)* frutto di un indirizzo politico che questo Governo rivendica con grande orgoglio. A quanti ci dicono - penso al senatore Manca - che ci sono nodi

proprio perché ha gli strumenti nella propria cassetta degli attrezzi per affrontarli finalmente con una visione chiara, univoca e unitaria, che in una parola mi permetterei di definire politica. Questa stessa nota politica ci consente di dire, come peraltro la Commissione europea ha avuto più volte modo di rilevare, che non conta soltanto quanto *deficit* si fa, ma come lo si usa. E non è un caso che gli apprezzamenti della Commissione europea rispetto a questa legge di bilancio siano stati tutti lusinghieri, non così per altri Paesi europei. Gran parte di questa legge di bilancio è stata fatta in *deficit*, ma è una legge di bilancio che non solo ha trovato il consenso dell'Europa sul quanto di *deficit*, ma anche sul metodo di utilizzo di questo *deficit*

Siamo orgogliosi di aver fatto questa scelta. In molti

volutamente prudente, che volutamente guarda alla congiuntura macroeconomica in modo razionale. È una legge di bilancio che non promette nulla che non possa realizzare, perché il tratto distintivo che abbiamo scelto è quello di non fare promesse irrealizzabili o o che si traducono in norme *boomerang* per il bilancio dello Stato, ma di fare soltanto promesse che potremo realizzare. In conclusione,

ma che è razionalmente il futuro che tutti noi vogliamo dare ai nostri figli e di cui orgogliosamente questo Governo fa parte. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Passiamo dunque all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli da 90 a 109). Ai sensi dell'articolo 129, comma 5, del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, e quindi i relatori e il rappresentante del Governo, per esprimere il rispettivo parere. Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che include le modifiche approvate dalla Commissione in sede referente, con una correzione di un riferimento interno e due specificazioni di natura tecnica, che non alterano la portata normativa sostanziale delle disposizioni a cui si riferiscono: l'articolo 1, commi 274, 291 e 525. Su tale emendamento, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, il Governo intende porre la questione di fiducia. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento.

1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», nel testo ritenuto ammissibile dalla Presidenza. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge, presentato dal Governo, e, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, che fin d'ora è autorizzata a convocarsi. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno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

siamo veramente molto preoccupati per quello che sta succedendo in un clima di incertezza che tutti gli operatori stanno affrontando. C'era tutto il tempo per raccogliere il lavoro che era stato fatto nel disegno e si potevano mettere a terra delle norme corrette. I decreti attuativi potevano andare in questa direzione e garantire sviluppo e innovazione al nostro territorio e alla nostra offerta turistica e dare la possibilità al nostro Paese di diventare competitivo e migliorare la propria offerta. Purtroppo, il tempo sta scadendo, il Governo Meloni ha avuto molto tempo per poter operare in questa direzione, ma soprattutto ha raggiunto un obiettivo, un obiettivo gravissimo, quello della dell'infrazione europea, che arriverà fra dieci giorni, con una serie di contenziosi e di ricorsi. Un regime di cristallizzazione dinastico che si è creato in questi anni anche per colpa delle proroghe e dell'incertezza che avevano i Comuni. Questa incertezza si è rivoltata contro

quelli che hanno i soldi, potranno tranquillamente intervenire, prendere le concessioni e portarle via dai piccoli balneari. Ecco, questo è il Governo. Questo è il tipo di Governo con cui abbiamo a che fare. che per anni racconta di difendere i piccoli imprenditori, mentre invece stava creando porte aperte per i grandi imprenditori che verranno facilmente a investire sui nostri territorio. Questo tempo schiacciato è stato tutto costruito costruito ad arte dal Governo. Noi abbiamo denunciato continuamente e siamo arrivati alla fine dell'anno. Questa è una delle ultime sedute, mancano dieci giorni per vedere se usciranno questi decreti attuativi, che sicuramente non ci saranno. Si apriranno delle grosse problematiche per gli imprenditori e, dall'altra parte, verrà fatto un bellissimo regalo di fine anno del Governo a tutti i cittadini italiani che dovranno pagare tutti l'infrazione cui ci ha portato questo Governo. Questo è il buon anno che ci lascia il Governo di incapaci, inadatti e pericolosi.